"Il link apre una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Gentile Presidente, informo la Signoria Vostra che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, adottato su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto l988, n. 400, della delega di funzioni conferite dal Ministro dell'economia e delle finanze, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il medesimo Dicastero on. Laura CASTELLI La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi giovedì 22 aprile, ha stabilito che nella seduta di domani avrà luogo la discussione congiunta delle mozioni nn. 341, 342 e 343 di sfiducia individuale nei confronti del Ministro della salute, a prima firma rispettivamente dei senatori Ciriani, Paragone e Crucioli. Per l'illustrazione di ogni singola mozione sono previsti cinque minuti. Ciascun Gruppo avrà a disposizione minuti per la discussione congiunta e dieci minuti per le dichiarazioni di voto. Per la votazione delle mozioni saranno indette tre chiame. Comunico, inoltre, che nella seduta di *question time* di giovedì 29 aprile, alle ore 15, è prevista la presenza dei Ministri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali. Restano confermati gli altri argomenti già previsti dal calendario della settimana corrente. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, professor Draghi.

Signor Presidente, onorevoli senatori,

Signor Presidente, onorevoli senatori, sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano nazionale di ripresa e resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, un insieme di numeri, di obiettivi, di scadenze. Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo: metteteci dentro le vite degli italiani, le nostre ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini che verranno, le attese di chi più ha sofferto gli effetti devastanti della pandemia, le aspirazioni delle famiglie preoccupate per l'educazione e il futuro dei propri figli, le giuste rivendicazioni di chi un lavoro non ce l'ha o lo ha perso, le preoccupazioni di chi ha dovuto chiudere la propria attività per permettere a noi tutti di frenare il contagio, l'ansia dei territori svantaggiati di affrancarsi da disagi e povertà, la consapevolezza di ogni comunità che l'ambiente va tutelato e protetto. Nell'insieme dei programmi che oggi presento alla vostra attenzione c'è però anche e soprattutto il destino del Paese, la misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità internazionale, la sua credibilità e la sua reputazione come fondatore dell'Unione europea e protagonista del mondo occidentale. Non è dunque solo una questione di reddito, lavoro, benessere ma anche di valori civili, di sentimenti della nostra comunità nazionale che nessun numero, nessuna tabella potranno mai rappresentare. Dico questo perché sia chiaro che, nel realizzare i progetti, ritardi, inefficienze e miopi visioni di parte anteposte al bene comune peseranno direttamente sulle nostre vite (soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e dei nostri figli e nipoti) e forse non vi sarà più tempo per porvi rimedio. Nel presentare questo documento al quale è strettamente legato il nostro futuro, vorrei riprendere, specie all'indomani della celebrazione dell'anniversario della liberazione d'Italia, la testimonianza di uno dei Padri della nostra Repubblica. Scriveva Alcide De Gasperi nel 1943: «vero è che il funzionamento della democrazia economica esige disinteresse, come quello della democrazia politica suppone la virtù del carattere. L'opera di rinnovamento fallirà se in tutte le categorie e in tutti i centri non sorgeranno degli uomini» - diremmo oggi delle persone - «disinteressati, pronti a faticare e sacrificarsi per il bene comune». «A noi l'onere e l'onore di preparare nel modo migliore l'Italia di domani». Prima di concentrarmi sulla descrizione del Piano, vorrei ringraziarvi per il prezioso lavoro di interlocuzione con istituzioni e parti sociali svolto dal Parlamento. La buona riuscita del Piano richiede uno sforzo corale delle diverse Istituzioni coinvolte e un dialogo aperto e costruttivo. Il Parlamento ha effettuato con rapidità - ne sono consapevole - un ingente lavoro di sintesi delle osservazioni e istanze di numerosi enti istituzionali, associazioni di categoria ed esperti, che ha contribuito alla fase finale di definizione del Piano. Tale lavoro di sintesi si è affiancato all'intensa collaborazione tra i diversi Ministeri a vario titolo coinvolti nella predisposizione del Piano. Si tratta di un lavoro che ha beneficiato grandemente dell'azione già svolta dal precedente Governo. Ringrazio anche le Regioni, le Province e i Comuni, il cui ruolo - come sappiamo e vedremo - va ben oltre le consultazioni. Gli enti territoriali sono determinanti per l'attuazione e la riuscita del Piano. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha tre obiettivi principali. Il primo, con un orizzonte temporale ravvicinato, risiede nel riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica. La pandemia ci ha colpito più dei nostri vicini europei: abbiamo raggiunto il numero di quasi 120.000 morti per il Covid-19, a cui si aggiungono i tanti mai registrati;

I giovani e le donne hanno sofferto un calo di occupazione molto superiore alla media, particolarmente nel caso dei giovani facenti parte della Le misure di sostegno all'occupazione e ai redditi dei lavoratori hanno notevolmente attutito l'impatto sociale della pandemia, che tuttavia si è sentito soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione. Tra il 2005 e il 2019 (quindi fino al momento della pandemia) il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta è salito dal 3,3 al 7,7 quindi da una storia di crescente povertà assoluta) ed è poi aumentato fino a quasi il 9,5 per cento nel 2020. Ancora una volta, ad essere colpiti sono stati donne e giovani e, ancora una volta, soprattutto nel Mezzogiorno. Con una prospettiva più di medio e lungo termine, il Piano affronta alcune debolezze che affliggono la nostra economia e la nostra società da decenni: i perduranti divari territoriali, le disparità di genere, la debole crescita della produttività e il basso investimento in capitale umano e fisico. Infine, le risorse del Piano contribuiscono a dare impulso a una compiuta transizione ecologica. Il Piano è articolato in progetti di investimento e riforme. L'accento sulle riforme è fondamentale. Queste, non solo consentono di dare efficacia e rapida attuazione gli stessi investimenti (senza queste riforme, dispero di spendere tutti questi soldi: insomma, è difficilissimo già ora), ma anche di superare le debolezze strutturali che hanno, per lungo tempo, rallentato la crescita e determinato livelli occupazionali insoddisfacenti, soprattutto per giovani e donne. Le riforme e gli investimenti sono corredati da obiettivi quantitativi e traguardi intermedi e sono organizzati in sei missioni. I progetti di ciascuna missione mirano ad affrontare tre nodi strutturali del nostro Paese, che costituiscono gli obiettivi orizzontali dell'intero Piano. Si tratta di colmare le disparità regionali tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord, le disuguaglianze di genere e i divari generazionali. Le risorse fornite attraverso il dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea sono pari a 191 miliardi e mezzo. Il Governo ha deciso di stanziare ulteriori 30,6 miliardi per il finanziamento di un Piano nazionale complementare da affiancare al dispositivo europeo. Questo Piano complementare finanzia progetti coerenti con le strategie del PNRR, che tuttavia eccedevano il tetto di risorse ottenibili con dispositivo europeo. PNRR e Piano nazionale complementare sono stati disegnati in modo integrato. Anche i progetti del secondo, cioè del Piano complementare, avranno gli stessi strumenti attuativi. Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche. Queste includono la linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, che diventerà una vera alta velocità: quindi, non più lenta di quella esistente. Inoltre, vi sarà l'attraversamento di Vicenza, relativo alla linea ad alta velocità Milano-Venezia. È poi previsto il reintegro delle risorse del Fondo sviluppo e coesione utilizzate nell'ambito del dispositivo europeo per il potenziamento dei progetti ivi previsti per 15 miliardi e mezzo. Nel complesso, insomma, potremo disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si aggiungono poi quelle rese disponibili dal programma React-EU, che, come previsto dalla normativa dell'Unione europea, vengono spese negli anni 2021-2023. Si tratta di altri fondi per ulteriori 13 miliardi. Se si tiene conto solo del Piano di resilienza e del fondo complementare, la quota dei progetti verdi è pari al 40 per cento quella dei progetti digitali è pari al 27 per cento. Il Piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno, su 206 miliardi, per una quota dunque del 40 per C'è una forte attenzione all'inclusione di genere e al sostegno per i giovani. Questo Piano, se attuato bene, ha effetti significativi su tutte le principali variabili economiche. Nel 2026 il prodotto interno lordo sarà di circa 3,6 punti percentuali superiore rispetto a uno scenario di riferimento che non tiene conto dell'attuazione del Piano. Ne beneficia anche l'occupazione, che sarà più elevata di 3,2 punti percentuali rispetto allo scenario di base nel triennio 2024-2026. Queste stime ipotizzano un'elevata efficienza degli investimenti pubblici effettuati, ma non quantificano l'ulteriore impulso che potrà derivare dalle riforme previste dal Piano e, per quanto riguarda l'occupazione femminile e giovanile, non tiene conto della clausola di condizionalità trasversale a tutto il Piano. L'accelerazione della crescita può essere superiore a quanto riportato nel PNRR se riusciamo ad attuare riforme efficaci e mirate a migliorare la competitività della nostra economia. Il governo del Piano è strutturato su diversi livelli. L'attuazione delle iniziative e delle riforme, nonché la gestione delle risorse finanziarie, sono responsabilità dei Ministeri e delle autorità locali, che sono chiamati a uno straordinario impegno in termini di organizzazione, programmazione e gestione. Le funzioni di monitoraggio, controllo, rendicontazione e i contatti con la Commissione europea sono affidati al Ministero dell'economia e delle finanze. È anche prevista una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio con il compito, tra l'altro, di interloquire con le amministrazioni responsabili in caso di riscontrate criticità nell'attuazione del Piano. Voglio sottolineare l'importante ruolo svolto da Regioni ed enti locali nell'ambito di attuazione del Piano. Sono, infatti, responsabili della realizzazione di quasi 90 miliardi di investimento, per cento del totale, in particolare con riguardo alla transizione ecologica, all'inclusione, alla coesione sociale e alla salute. La prima missione riguarda il tema della digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Nel complesso, le risorse destinate a questa missione sono quasi 50 miliardi, di cui 41 finanziati con il dispositivo europeo e 8,5 con il Piano complementare nazionale, pari al 27 per cento delle risorse totali del Piano. L'obiettivo principale è promuovere e sostenere la trasformazione digitale e l'innovazione del sistema produttivo del Paese. Abbiamo scelto di investire nella crescita dimensionale delle nostre imprese e in filiere ad alta tecnologia. Una particolare attenzione va poi al turismo e alla cultura, ma facciamo un attimo un passo indietro rispetto a questi numeri e riflettiamo che è facile, quando si parla di digitale, parlare di fibra, di *cloud*, di 5G, di identità digitale, di telemedicina e delle molte altre tecnologie sulle quali proponiamo di investire. In realtà, dobbiamo chiederci per cosa la trasformazione digitale è essenziale per il nostro Paese. Noi vogliamo che dal 2027 le nostre ragazze e ragazzi possano avere accesso alle migliori esperienze educative, ovunque esse siano in Italia. Vogliamo che i nostri imprenditori, piccoli e grandi, possano lanciare e far crescere le loro attività rapidamente ed efficientemente. Vogliamo permettere alle donne imprenditrici di realizzare i loro progetti; vogliamo che i lavoratori e le lavoratrici continuino ad acquisire le competenze per le professioni di oggi e di domani. Vogliamo che le persone più sole e vulnerabili possano essere assistite da operatori sanitari, dai volontari e dai loro familiari nel migliore e più tempestivo modo possibile. Vogliamo che le pubbliche amministrazioni e i loro servizi siano accessibili senza ostacoli, senza costi e senza inutile spreco di tempo. Vogliamo, insomma, accelerare l'adozione della tecnologia nel pubblico, nel privato e nelle famiglie per dare alla fine del quinquennio 2021-2026 eque opportunità a tutti, in particolare a giovani e donne e, soprattutto, a chi vive nei territori meno connessi. *(Applausi)*. Per il rilancio della cultura e del turismo, due settori chiave per l'Italia anche per il loro significato identitario, una prima linea di azione riguarda interventi di valorizzazione di siti storici e culturali, volti a migliorare la capacità attrattiva, la sicurezza e l'accessibilità dei luoghi. Gli interventi sono dedicati non solo ai cosiddetti grandi attrattori, ma anche alla tutela e alla valorizzazione dei siti minori. Si aggiungono misure per una riqualificazione ambientalmente sostenibile delle strutture e dei servizi turistici, che fanno leva anche sulle nuove tecnologie. Il Piano non trascura il fatto che il rafforzamento della digitalizzazione e la spinta all'innovazione devono essere realizzati in maniera sinergica tra settori e aree di intervento. Molte misure di cui dirò più avanti relativamente ad altre missioni, ad esempio relativamente a istruzione e ricerca o sanità, completano la strategia del Governo in questa area. La seconda missione, denominata rivoluzione verde e transizione ecologica, si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento. Essa è particolarmente importante per l'Italia perché - in parte per l'orografia, in parte per la delicatezza dei siti ambientali ma anche per gli abusi a cui è stata sottoposta - è maggiormente esposta a rischi climatici rispetto ad altri Paesi. La missione migliora la sostenibilità del sistema economico e assicura una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero. La dotazione complessiva di questa missione è la più cospicua tra le sei proposte (quasi 70 miliardi, di cui 60 finanziati con il dispositivo europeo). Vi sono inoltre investimenti a supporto della transizione ecologica anche in altre missioni. Questa prevede misure per migliorare la gestione dei rifiuti e per l'economia circolare; rafforza le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammoderna o sviluppa nuovi impianti di trattamento rifiuti. Per raggiungere la progressiva decarbonizzazione sono previsti interventi per incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per il rafforzamento delle reti e una mobilità più sostenibile. Vi è uno sforzo significativo per promuovere l'efficientamento energetico di edifici pubblici e privati. Per il superbonus al 110 sono previsti, tra PNRR e Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal precedente Governo. Non c'è alcun taglio. La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le case popolari. È un provvedimento importante per il settore delle costruzioni e per l'ambiente. Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione quest'anno, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici. Inoltre, nella missione non sono stati trascurati i temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici, della salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, e quelli relativi all'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno e alla disponibilità di risorse idriche. La missione 3 dispone una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa. questa finalità sono allocati oltre 31 miliardi di euro. Gran parte delle risorse è destinata all'ammodernamento e al potenziamento della rete ferroviaria. Si prevede il completamento dei principali assi ferroviari ad alta velocità e ad alta capacità, per una spesa stimata in 13,2 miliardi di euro, l'integrazione tra questi e la rete ferroviaria regionale e la messa in sicurezza dell'intera rete. Vi sono poi interventi per la digitalizzazione del sistema della logistica, per migliorare la sicurezza di ponti e viadotti e misure per innalzare competitività, capacità e produttività dei porti italiani. La missione 4, "Istruzione e ricerca", incide su fattori indispensabili per un'economia basata sulla conoscenza. Oltre ai loro risvolti benefici sulla crescita, tali fattori sono determinanti anche per l'inclusione e l'equità. I progetti proposti intendono rafforzare il sistema educativo lungo tutto il percorso di istruzione, sostenere la ricerca e favorire la sua integrazione con il sistema produttivo. Gli interventi principali riguardano il miglioramento qualitativo e l'ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione, a partire dal rafforzamento dell'offerta di asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, lo sviluppo e il rafforzamento dell'istruzione professionalizzante, i processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti, il potenziamento e l'ammodernamento delle infrastrutture scolastiche, ad esempio con il cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici, la riforma e l'ampliamento dei dottorati, il rafforzamento della ricerca e la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata, condotta in sinergia tra università e imprese, il sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico. A questa missione sono destinati quasi 32 miliardi di euro, di cui 1 finanziato con risorse nazionali, tramite il fondo complementare, e 31 con il dispositivo europeo. La quinta missione è destinata alle politiche attive del lavoro e della formazione, all'inclusione sociale e alla coesione territoriale. I fondi destinati a questi obiettivi superano nel complesso i 22 miliardi di euro e ulteriori 7,3 miliardi di euro di interventi beneficeranno delle risorse del Fondo React-EU. Sono previsti investimenti in attività di formazione e riqualificazione dei lavoratori, si prevedono l'introduzione di una riforma organica integrata in materia di politiche attive e formazione, nonché misure specifiche per favorire l'occupazione giovanile. Sono introdotte misure a sostegno dell'imprenditorialità femminile e un sistema di certificazione della parità di genere, che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il *gap* di genere. Si è scelto poi di destinare importanti risorse alle infrastrutture sociali funzionali alla realizzazione di politiche a sostegno delle famiglie, dei minori, delle persone con gravi disabilità e degli anziani non autosufficienti. *(Applausi)*. A queste si affiancano misure per la riqualificazione dei tessuti urbani più vulnerabili, in particolare le periferie e le aree interne del Paese, e interventi di potenziamento dell'edilizia residenziale pubblica e di *housing* temporaneo e sociale. Mi scuso di nuovo, ma sono le parole che sono entrate nei vari programmi. La missione 6 riguarda la salute, un settore critico, che ha affrontato sfide di portata storica nell'ultimo anno. La pandemia da Covid-19 ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macroeconomica dei servizi sanitari pubblici. Le riforme e gli investimenti proposti con il Piano in quest'area hanno due obiettivi principali: rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio e modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, al fine di garantire un equo accesso a cure efficaci. La dotazione per questa missione è complessivamente di 18,5 miliardi, di cui 15,6 relativamente a finanziamenti del dispositivo europeo e 2,9 di risorse nazionali. Particolare attenzione è stata dedicata in questa missione all'assistenza domiciliare. Il volume delle prestazioni in assistenza domiciliare aumenterà significativamente, fino a prendere in carico, entro il 2026, il 10 per cento di coloro che hanno un'età sopra i sessantacinque anni, in particolare con patologie croniche o non autosufficienti. Il miglioramento delle prestazioni erogate sul territorio è perseguito attraverso il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali (come le case della comunità e gli ospedali di comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. A queste misure si affiancano progetti per il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti; per il completamento e la diffusione del fascicolo sanitario elettronico; per una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Rilevanti risorse sono destinate, inoltre, alla ricerca scientifica, a favorire il trasferimento tecnologico, a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio sanitario nazionale. Nel più generale ambito socio-sanitario, si introduce un'importante riforma per la non autosufficienza, con l'obiettivo primario di offrire risposte ai problemi degli anziani. Questa misura affronta in maniera coordinata i diversi bisogni che scaturiscono dalle conseguenze dell'invecchiamento. Vogliamo che i nostri anziani possano essere messi in condizione di mantenere o riguadagnare la massima autonomia possibile, in un contesto il più possibile deistituzionalizzato. Dopo le sofferenze e le paure di questi mesi di pandemia, credo sia il minimo che possiamo fare. Vediamo ora l'impatto del Piano su donne, giovani e Sud. Eliminare gli ostacoli che limitano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è fondamentale per la ripresa del nostro Paese. Il Piano interviene sulle molteplici dimensioni del divario di genere e si inserisce nel percorso di riforma avviato con il Family Act (questo il nome della legge). Il Governo Il Governo intende lanciare entro il primo semestre 2021 la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026. Il PNRR sviluppa le priorità di questa Strategia nazionale e le articola in un ampio programma: 4,6 miliardi sono destinati a costruire nuovi asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia; quasi un miliardo va a finanziare l'estensione del tempo pieno nelle scuole primarie per permettere alle famiglie - e alle madri, in particolare - di conciliare meglio la loro vita professionale e lavorativa. Il Piano prevede 400 milioni per favorire l'imprenditorialità femminile, e stanzia oltre un miliardo per la promozione delle competenze in ambito tecnico-scientifico, soprattutto per le studentesse. Infine, grazie all'azione di questo Parlamento, l'assegno unico diventerà lo strumento centrale e onnicomprensivo per il sostegno alle famiglie con figli, in sostituzione delle misure frammentarie fino ad oggi vigenti. È una riforma che rappresenta un cambio di paradigma nelle politiche per la famiglia e a sostegno della natalità. Un Piano che guarda alle prossime generazioni deve infatti riconoscere la nostra realtà demografica. Siamo uno dei Paesi con la più bassa fecondità in Europa, meno di 1,3 figli per ciascuna donna contro quasi 1,6 della media europea. Per mettere i nostri giovani nella condizione di formare una famiglia dobbiamo rispondere a tre loro richieste: un *welfare* adeguato, una casa e un lavoro sicuro.

Oltre al piano degli asili nido, di cui ho già parlato, i giovani beneficiano delle misure per le infrastrutture sociali e le case popolari. In un prossimo decreto-legge sono previste altre risorse per aiutare i giovani a contrarre un mutuo per acquistare una casa e in particolare, oltre ad agevolazioni fiscali significative, per ridurre l'anticipo grazie all'introduzione di una garanzia dello Stato. Poco meno di 2 miliardi di euro (1,8 miliardi) vanno ad accrescere la competitività delle imprese turistiche, di cui una parte importante è destinata ad incentivare la creazione di nuove imprese per chi ha meno di Potenziamo il servizio civile universale per i giovani tra i diciotto e i ventotto anni, a cui destiniamo 650 milioni per il periodo 2021-2023. Si tratta di una forma di cittadinanza attiva che, allo stesso tempo, è uno strumento di formazione e un motore di inclusione e coesione sociale. I giovani possono orientarsi rispetto allo sviluppo della propria vita professionale e, allo stesso tempo, rendere un servizio nobile alla propria comunità e all'Italia. Sempre per i giovani investiamo 600 milioni per rafforzare il sistema duale e rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea col mercato del lavoro. Questo intervento agevola l'occupazione giovanile e, allo stesso tempo, viene incontro alle esigenze delle imprese in termini di competenze. Tra le altre misure legate all'istruzione, ribadiamo la centralità dello sport nel percorso formativo dei ragazzi e delle ragazze.

la invito a stare seduto. Non le ho dato la parola, stia seduto. Non si permetta. L'Aula la dirigo io. Per cortesia, l'Aula la dirigo io. Basta. Prego, presidente

Il Piano dedica 1 miliardo alle strutture sportive per i giovani, in parte dedicato a nuove palestre e attrezzature sportive nelle scuole, in parte a rafforzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale e di contrasto alla marginalizzazione. Più in generale, i giovani saranno tra i principali beneficiari di tutto il piano. Gli investimenti e le riforme sulla transizione ecologica creeranno principalmente occupazione giovanile. La creazione di opportunità per i giovani nel mondo del lavoro sarà anche l'effetto naturale degli interventi della digitalizzazione, che tra l'altro, come dicevo prima, consentiranno di completare la connettività tra le scuole. Il Piano prevede inoltre una specifica attenzione per le persone con disabilità, nell'ambito degli interventi per ridurre i divari territoriali nella scuola secondaria di secondo grado. Gli interventi per la mobilità, il trasporto pubblico locale e le linee ferroviarie favoriscono il miglioramento e l'accessibilità di infrastrutture e servizi per tutti i cittadini. È previsto un investimento straordinario sulle infrastrutture sociali nonché sui servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari. Il miglioramento di questi servizi sanitari sul territorio favorisce un accesso realmente universale alla sanità pubblica. Si prevede, infine, di introdurre la legge quadro sulle disabilità per semplificare l'accesso ai servizi e i meccanismi di accertamento. Nel corso dell'attuazione del Piano, l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità monitorerà che le riforme proposte siano adeguatamente inclusive. La crescita del Mezzogiorno rappresenta l'altro aspetto prioritario trasversale al Piano. Il potenziale del Sud in termini di sviluppo, competitività e occupazione è tanto ampio quanto è grande il suo divario dal resto del Paese. Non è una questione di campanili: se cresce il Sud, cresce l'Italia. per cento del totale degli investimenti in infrastrutture - soprattutto l'Alta velocità ferroviaria e il sistema portuale - è diretto al Sud. Gli interventi su economia circolare, transizione ecologica, mobilità sostenibile e tutela del territorio e della risorsa idrica destinano al Mezzogiorno 23 miliardi. A questi investimenti si accompagnano la riforma delle Zone economiche speciali e un robusto finanziamento della loro dotazione infrastrutturale, pari ad oltre 600 milioni.

L'obiettivo è rendere il Mezzogiorno un luogo di attrazione di capitali privati e di imprese innovative. Come dicevo, il PNRR non è soltanto un piano di investimenti, ma anche e soprattutto di riforme. La riforma della giustizia affronta i nodi strutturali del processo civile e penale. Nonostante i progressi degli ultimi anni, permangono ritardi eccessivi. In media sono necessari oltre 500 giorni per concludere un procedimento civile in primo grado, a fronte dei circa 200 in Germania. Il Piano rivede l'organizzazione degli uffici giudiziari e crea l'ufficio del processo, una struttura a supporto del magistrato nella fase "conoscitiva" della causa. Nel campo della giustizia civile si semplifica il rito processuale in primo grado e in appello e si dà definitiva attuazione al processo telematico, come richiesto nei mesi scorsi dal Senato. Il Governo intende ridurre l'inaccettabile arretrato presente nelle aule dei tribunali e creare i presupposti per evitare che se ne formi di nuovo. Questo è uno degli impegni più importanti ed espliciti che abbiamo preso verso l'Unione europea. L'obiettivo finale che ci proponiamo è ambizioso: ridurre i tempi dei processi del 40 per cento per il settore civile e almeno del 25 per vogliamo un sistema giudiziario strutturalmente più efficiente. Tutti noi vogliamo elevare la qualità della risposta del sistema. La seconda riforma di sistema riguarda la pubblica amministrazione, sulla cui capacità di rispondere in modo efficiente ed efficace incidono diversi fattori. Tra questi: la stratificazione normativa, la limitata e diseguale digitalizzazione, lo scarso investimento nel capitale umano dei dipendenti, l'assenza di ricambio generazionale e di aggiornamento delle competenze. La riforma interviene su quattro ambiti principali: assunzioni e concorsi, mediante una razionalizzazione delle procedure di assunzione e una programmazione degli organici mirata a fornire servizi efficienti a imprese e cittadini; buona amministrazione, grazie a una semplificazione del quadro normativo e procedurale; rafforzamento delle competenze, tramite una revisione dei percorsi di carriera, la formazione continua del personale e lo sviluppo professionale; la digitalizzazione, con investimenti in tecnologia, la creazione di unità dedicate alla semplificazione dei processi e la riorganizzazione degli uffici. Inoltre, entro maggio, presenteremo un decreto che interviene con misure di carattere prevalentemente strutturale volte a favorire l'attuazione del PNRR e del Piano complementare. Oltre a importanti semplificazioni negli *iter* di attuazione e di valutazione degli investimenti in infrastrutture, si procede a una semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni. Il Piano vuole anche impegnare Governo e Parlamento a una continuativa e sistematica opera di abrogazione e modifica delle norme che frenano la concorrenza, creano rendite di posizione e incidono negativamente sul benessere dei cittadini. Questi principi sono essenziali per la buona riuscita del Piano. Dobbiamo impedire che i fondi che ci accingiamo a investire finiscano soltanto ai monopolisti. A questo fine assume un ruolo cruciale la legge annuale sulla concorrenza, prevista nell'ordinamento nazionale dal 2009, ma realizzata solo una volta, nel 2017. Intendiamo varare norme volte ad agevolare l'attività di imprese in settori strategici, come le reti digitali e l'energia. Alcune di queste norme sono già individuate nel Piano, ad esempio il completamento degli obblighi di gara per i regimi concessori oppure la semplificazione delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Il Governo si impegna a mitigare gli effetti negativi che alcune di queste misure potrebbero produrre, rafforzando i meccanismi di regolamentazione e la protezione sociale. devo ringraziare questo Parlamento per l'impulso politico che anima tutto il Piano: l'attenzione a ambiente, giovani, donne, Mezzogiorno che informa ogni intervento è prima di tutto frutto della vostra azione. Sono certo che riusciremo ad attuare questo Piano. Sono certo che l'onestà, l'intelligenza, il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, la stupidità e gli interessi costituiti. Questa certezza non è sconsiderato ottimismo, ma fiducia negli italiani, nel mio popolo, nella nostra capacità di lavorare insieme quando l'emergenza ci chiama alla solidarietà, alla responsabilità. È con la fiducia che questo appello allo spirito repubblicano verrà ascoltato e si tradurrà nella costruzione del nostro futuro che presento oggi questo Piano.

sono otto anni che partecipo ai lavori di questo Parlamento e mai come oggi mi trovo e ci troviamo a partecipare al voto su un provvedimento di così enorme rilievo per il futuro di questo Paese.

una relazione che il Senato era prossimo a licenziare all'indirizzo del Governo da lei presieduto perché ne facesse tesoro in vista del testo che oggi ci presenta. In quell'intervento affrontai principalmente tre temi, relativi alle politiche della ricerca, apprezzando alcune iniziative e avvertendo il suo Governo della forte criticità di altre. Voglio qui ripercorrere quei punti e quelle criticità alla luce del nuovo testo, perché quest'Assemblea possa continuare a tracciare un confronto aperto e pubblico. Il primo aspetto sul quale voglio richiamare la sua attenzione riguarda le risorse per la ricerca. So bene che studiosi e ricercatori fuori di qui avrebbero desiderato vedere allocare molti più fondi alla ricerca e veder riconosciuto il necessario investimento soprattutto nella ricerca di base, quella libera dei tanti piccoli gruppi di ricerca e laboratori, degli studiosi ossessionati da una domanda, guidati da una visione, spinti dalla perseveranza, che vengono lasciati lavorare sulla loro capacità di trasformare la curiosità per un fatto in pezzi di conoscenza per tutti. Guardate che il nostro sviluppo nasce così, in questi piccoli laboratori e gruppi di cui è disseminato il Paese, nasce in quegli studiosi ossessionati. In poche parole nasce dalla ricerca di base, umanistica e scientifica, senza la quale nessuna nuova tecnologia può essere sviluppata e quindi nessun trasferimento tecnologico può essere possibile. Da persona che ha sempre fatto del metodo scientifico la sua bussola, talvolta risulta difficile accettare che le decisioni che si prendono in queste Aule siano frutto di molti compromessi, invece di essere chiare, nette e univoche. È bene quindi ribadire che quelli previsti dal PNRR sono importanti piani di investimento in ricerca, ma straordinari. Io mi aspetto che il Paese che si prepara - usando le parole del presidente Draghi - ad un ammodernamento riconosca la necessità di avere come voce strutturale del bilancio dello Stato fondi specifici per la ricerca di base, per gli studi in tutti gli ambiti umanistici, artistici, scientifici *(Applausi)*; una voce di bilancio di un ordine di grandezza mai visto in passato, allocata solo ed esclusivamente in maniera competitiva e trasparente, con importi e tempistiche certe. Chiediamo l'ordinario oltre allo straordinario. Oggi le risorse che si è scelto di investire non sono in grado di compensare la deprivazione sofferta nell'ultimo ventennio dal settore, ma rappresentano senza dubbio una base importante del rilancio della ricerca italiana e attraverso la ricerca, attività per definizione più orientata al futuro, del rilancio economico, sociale e culturale del Paese, a partire dalle aree storicamente più svantaggiate.

L'auspicio è che si inverta la tendenza degli ultimi vent'anni in cui il sottofinanziamento sistematico della ricerca pubblica ha fortemente limitato le potenzialità delle università, in particolare di quelle situate in territori svantaggiati del Paese, di esercitare il ruolo (che sarebbe loro proprio) di motore di sviluppo e di ascensore sociale. In quei territori il numero di studenti è diminuito in misura maggiore rispetto alla media nazionale e certamente questa diminuzione non è avvenuta in maniera uniforme tra le classi sociali. Per questo al secondo punto del mio intervento si trovano le misure per i giovani. Ho apprezzato l'enfasi che il Piano pone sul dottorato di ricerca, un percorso che deve essere pieno di ricerca e studio. Con l'aumento di 3.600 dottorati arriva il segnale atteso da anni che si è compreso come una nuova e numericamente consistente generazione di giovani, uscita da questo percorso di alta formazione, possa fecondare, con la mentalità e l'approccio del ricercatore, tutti i settori della società. Servirà però una semplificazione rispetto agli attuali settori scientifico-disciplinari, che molto spesso diventano gabbie obsolete e inutili rispetto a una formazione interdisciplinare ormai indispensabile, dove però per interdisciplinarietà non si deve intendere nessuna rinuncia all'approfondimento delle materie affrontate. Ho dubbi, invece, sulla misura che introduce ingenti risorse per i cosiddetti 5.000 dottorati innovativi che rispondono a fabbisogni delle imprese. Credo infatti semplicemente che queste non debbano essere conteggiate come risorse per la ricerca, in quanto esulano dall'ambito proprio della ricerca. L'Europa ci chiede di investire sui giovani oltre ai dottorati, un investimento, almeno della stessa portata, dovrebbe essere rivolto a quell'importante Programma per i giovani ricercatori, previsto dal Piano, per il quale le risorse andrebbero almeno raddoppiate. Quelli per i giovani ricercatori sono infatti fondi per accendere nuovi laboratori di ricerca, nuovi gruppi guidati da giovani studiosi, che si saranno conquistati le risorse per studiare e ricercare almeno per i prossimi cinque anni. Liberi, autonomi, indipendenti.

Sarebbe un fallimento drammatico se questo programma venisse piegato ad ingrossare le file di qualche cordata accademica o non accademica egemone. Sarebbe però bellissimo - e ne approfitto per la presenza anche della Ministra per il Sud e la coesione territoriale - vedere qui, sul Programma per i giovani ricercatori, un rafforzamento e un ampliamento dello stesso, frutto dell'impegno in sede governativa anche della Ministra per prevedere due misure - che definirei speciali - di coesione e inclusione, dedicate ad aree svantaggiate. In particolare, azioni *top-up* che permettano un sostanziale incremento del finanziamento vinto dal giovane studioso, anche fino al 30-50 per cento, se il progetto viene realizzato in enti al Sud o in aree interne. Questo per incentivare i processi virtuosi di contrasto alle disuguaglianze geografiche, ma anche misure speciali di parità di genere e sostegno alla famiglia per consentire alla studiosa o allo studioso, che usufruisca di un congedo di genitorialità, di nominare un sostituto di fiducia che ne faccia le veci manageriali per l'intero periodo di assenza, garantendo continuità ai progetti. Vengo ora al terzo e ultimo punto. Nel mio intervento dello scorso 31 marzo evidenziavo il rischio che i proposti sette centri di ricerca e i probabili 20 campioni territoriali di ricerca e sviluppo menzionati nella bozza del Piano, alcuni già individuati con nome e cognome, diventassero delle cattedrali nel deserto, nuovi feudi dorati, presumibilmente finanziati a cascata, senza valutazione, né misura del merito, come succede per alcuni enti anche ora, slegati dai territori e dal resto del mondo della ricerca.

e lo si è fatto nel miglior modo possibile e lo si è fatto - lo voglio riconoscere - fino all'ultimo correggendo versioni preparatorie che raccontavano ben altro e di ben peggio. Si è affermato cioè un solido principio, presidente Draghi, che le chiedo veramente di difendere in ogni sede, e poi lo si è declinato: la pietra angolare su cui edificare le misure di promozione della ricerca è l'aver individuato per tutte le misure promosse procedure di selezione su base competitiva. Nel piano definitivo si parla ancora di centri di ricerca, campioni territoriali, ecosistemi dell'innovazione, ma è comunque esplicitato e ribadito in più occasioni un richiamo a quelle selezioni aperte e competitive per stabilire quali progetti potranno meglio valorizzare e far emergere le eccellenze della ricerca già esistenti in tutta Italia, spesso solamente sconosciute alla politica e ai cittadini. Inoltre, per il coordinamento delle misure del MUR è prevista la creazione di un apposito *supervisory board.* Dalla bontà e dall'efficacia del lavoro di quest'organo dipende l'efficacia e l'effettività di tanta parte delle misure di cui oggi leggiamo. Sono fiduciosa che nell'implementare queste soluzioni si seguirà anche quanto più volte ribadito dalla ministra Messa, ovvero non mattoni, ma investire sulla messa a bando di grandi progetti di coordinamento, sui temi stabiliti o da stabilire, a cui in tanti concorreranno, realizzando cordate in competizione tra loro, con messa in rete di strutture, talenti, professionalità, conoscenze e competenze già presenti e diffuse in tutto il Paese. Penso all'intero ecosistema della ricerca, che annovera oltre 135 enti che già si occupano di ricerca nei vari settori. Ebbene, il PNRR che oggi ci presenta - mi è chiaro - non fa eccezione al necessario compromesso politico tra esigenze diverse e risorse che, pur in una disponibilità mai vista prima, sono scarse quando confrontate con le più disparate aspettative. In questo senso, il vincolo esterno, il rapportarsi con un soggetto erogatore come la Commissione europea, che ha preteso e pretenderà specifici oneri di finalizzazione e competizione, trasparenza e rendicontazione degli interventi, è salutare. La fiducia degli studiosi nelle politiche italiane per la scienza, presidente Draghi, è stata persa negli anni passati, dopo anni di assegnazioni di fondi senza competizioni, in nome di eccellenze mai verificate a progetti, a ricerche, a centri nati e imposti *ope legis*, senza nemmeno studiare e capire se fossero necessari, se quello fosse il miglior modo di studiare e di far ricerca. La fiducia, però, si può riconquistare proprio con il coinvolgimento di tutti, con procedure quanto più possibile aperte e trasparenti; seguirle, rispettarle e implementarle dove necessario sarebbe tanto semplice quanto rivoluzionario e porterebbe un effetto virtuoso di credibilità esterna nei confronti dell'Europa che investe sul nostro rilancio, oltre che interna da parte degli studiosi verso una politica che per anni non li ha ascoltati e ne ha ignorato le esigenze.

questo Piano nazionale di ripresa e resilienza ci mette nelle condizioni di farcela, ci offre strumenti per superare le difficoltà sanitarie ed economiche e per andare oltre, affinché la crisi provocata dal Covid possa diventare quell'opportunità di cui il Paese ha bisogno da tempo, un'occasione per creare un futuro di sviluppo e progresso e per superare tanti nodi irrisolti, dalla burocrazia alla scarsa produttività, dalla disoccupazione giovanile al dislivello tra Nord e Sud del Paese. Adesso ce la si può fare, perché grazie all'Europa disponiamo di ingenti risorse. Italia Viva abbiamo fortemente voluto un cambio di passo rispetto all'Esecutivo precedente, perché ci rendevamo conto che stavamo andando troppo a rilento e che il Governo non riusciva a mettere in campo risposte adeguate né rispetto alla gravità della pandemia, né sul piano di spesa per gli anni a venire, dunque un piano che nella versione attuale segna invece una svolta. È di buon auspicio il fatto che la sua presentazione coincida con le prime riaperture di questi giorni. Si tratta di un testo che non è più il copia-incolla di progetti datati, ma è una vera e propria visione strategica per il Paese, che ci mette nelle condizioni di essere all'altezza delle sfide del futuro. Il nuovo testo è in sintonia con le richieste che Italia Viva sta portando avanti da tempo. Innanzitutto la parte dedicata al piano infrastrutturale: sono oltre 25 i miliardi di euro previsti per potenziare l'Alta velocità, soprattutto al Sud, e per costruire reti intermodali di collegamento che coinvolgano anche le aree periferiche. Siamo convinti che massicci investimenti in infrastrutture pubbliche siano una boccata d'ossigeno a favore della ripresa economica. Connettere le aree rurali a quelle urbane, collegare più velocemente alcune zone ancora troppo isolate non è solo un atto di equità, ma è anche un modo pratico per spingere l'economia, anche grazie ad un forte intervento di digitalizzazione sulle reti ferroviarie, sulla catena logistica di trasferimento delle merci e sui sistemi portuali, tutte scelte molto opportune, perché non possiamo accettare che il futuro di tanti nostri territori venga impedito dal numero di rotaie che ancora oggi mancano. Anche perché trasferire il traffico dai mezzi su gomma a quelli su rotaia ha un'ulteriore implicazione, ossia limitare in modo consistente le emissioni di gas serra. Ciò, peraltro, vuol dire perseguire un altro degli importanti obiettivi che intendiamo raggiungere, ossia l'abbattimento del riscaldamento climatico. Apprezziamo anche tutto il pacchetto relativo alla conciliazione tra vita familiare e carriera professionale e al sostegno alle pari opportunità e alla genitorialità. È positivo prevedere la creazione di oltre 220.000 nuovi posti di asilo nido e oltre 1.000 mense per scuole a tempo pieno, perché rappresentano una spinta all'occupazione femminile. Il lavoro femminile, se fosse pari a quello maschile, farebbe crescere il nostro prodotto interno lordo di 88 miliardi di euro.

Act* e dalla necessità di creare *chance* per i propri giovani. Ciò è positivo perché il compito della politica oggi non può essere stanziare risorse per l'assistenzialismo, invece intervenire sulla formazione facendo sì che diventi sempre più d'eccellenza e che vi siano sufficienti posti di lavoro capaci di garantire la realizzazione personale dei giovani all'interno del proprio Paese, senza che siano costretti a dover andare altrove. Bisogna poi cercare di far fare passi da gigante al nostro Paese in materia di connettività, nel tentativo di recuperare i ritardi accumulati e riuscire a non perdere la sfida di quell'economia dell'innovazione, destinata a segnare la ripresa *post* pandemia. Per questo, sono strategici gli investimenti dedicati al mondo del sapere, alla digitalizzazione, alla formazione e alla ricerca. Puntare oltre il 20 per cento delle risorse complessive su questi ambiti vuol dire favorire la crescita economica del Paese, anzitutto attraverso la modernizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di renderla più competente, semplice, connessa, al servizio dei cittadini e in grado di evolvere al meglio. Allo stesso tempo, significa anche prevedere uno stanziamento ambizioso attraverso il quale modernizzare le industrie produttive e il mondo del turismo e della cultura. Strategici sono anche gli investimenti nel campo della ricerca, a partire dall'ambito medico-sanitario. L'emergenza Covid ci ha dimostrato quanto sia urgente e proficuo investire in enti di ricerca, telemedicina e modernizzazione delle strutture ospedaliere. La pandemia ci ha soprattutto insegnato che stanziare risorse per la sanità non è un costo, ma un investimento di cui beneficia la stessa economia del Paese. Sarebbe pertanto senz'altro utile fare il possibile per aumentare ulteriormente il *budget* per la sanità e la ricerca. Intanto salutiamo con favore l'aumento del numero di borse di studio per dottorandi e specializzandi, come pure il potenziamento della formazione duale e continua, perché sono tutte misure che mirano ad ampliare le competenze del capitale umano, del capitale umano, che rappresenta la risorsa più importante nella civiltà della conoscenza. Siamo orgogliosi che questo PNRR sia una vera rivoluzione verde, anzitutto decine di miliardi di euro per interventi contro il dissesto idrogeologico e per la tutela e la valorizzazione del territorio: tutti interventi che fanno sì che la svolta ecologica diventi uno straordinario motore di crescita e benessere. In sostanza, si tratta di una serie di misure che puntano al progresso economico e sociale del Paese. Semplice, inclusiva e *green:* questa è l'Italia del futuro che possiamo realizzare con le risorse di questo Piano nazionale di ripresa e resilienza, il quale crea le basi per il domani e aiuta il Paese a risollevarsi e a costruire un'Italia dinamica che, con un colpo di reni, ci porti in un futuro digitale, ecologico e prospero; un'Italia, signor Presidente, in cui tutti possano avere di nuovo un'opportunità.

Noi di Fratelli d'Italia riteniamo che la collaborazione tra Governo e Parlamento sia fondamentale, ma, alla stregua del Governo precedente, non si rispetta lo spazio che spetterebbe alle forze politiche. Pertanto, si dovrebbe tornare al più presto ad un equilibrio democratico, dando voce al popolo. Siamo stati autorizzati dall'Europa, ma i rappresentanti del popolo non hanno avuto neanche il tempo per discuterne i contenuti appieno. Nessuno è a conoscenza delle ripercussioni che questo programma potrà avere sulle generazioni future. Non si può più sbagliare. I fondi destinati al Sud devono essere investiti con cognizione di causa. Al Sud dobbiamo ridare dignità alle persone, ai docenti, alle famiglie, alla natalità che è sempre stata un punto di forza ma che negli anni, a causa della recessione economica, è andata via via peggiorando, soprattutto per le fasce più deboli. Assistiamo all'implementazione di alcuni provvedimenti, per i quali, al contrario, per i quali, al contrario, si parte dall'arrivo anziché dall'inizio. Mi riferisco, in questo caso, alla scuola e al piano di reclutamento dei docenti. Questo è un momento unico per poter realizzare quello che da anni si dice all'interno della scuola: trasformare le cattedre di diritto in cattedre di fatto; le cattedre di fatto in cattedre di diritto; le cattedre in deroga in cattedre di diritto. Ma veniamo al punto che riguarda *in primis* le donne, le nostre insegnanti, il mondo della scuola. Dove sono le pari opportunità tanto decantate dal PNRR e dal Governo di unità nazionale? In questo modo, tutta una serie di diritti garantiti oltre che a livello nazionale anche a quello europeo (come i diritti ad avere una famiglia, una equa retribuzione, una stabile dimora, nonché il diritto ad una integrità fisica), sono tutti posti a repentaglio nel perdurare di anni di servizio fuori sede; anni d'obbligo previsti per legge. In realtà, il servizio da loro prestato è stato ampiamente duplicato, triplicato, quadruplicato. Se si continuerà su questa scia, dove andremo a finire? Forse si ritiene più utile assicurare la temerarietà della lite? Chi ne potrebbe trarre vantaggio? Oppure siamo già in campagna elettorale, per cui 10.000-12.000 docenti sono meno appetibili di 68.000 o di 500.000? Dal 2008 ad oggi, assistiamo ad un progressivo ridimensionamento dei diritti del lavoratore dipendente fuori sede e la situazione di pandemia ne ha aggravato gli effetti. Si deve agire ora, non domani. Presidente Draghi, signori Ministri (mi rivolgevo ai ministri Orlando, Bianchi e Brunetta, ma nessuno dei tre è presente), gentili colleghi, si tratta di semplificare. Ulteriori ed evidenti criticità avrebbero sede nei metodi di lavorazione delle pratiche di pensionamento del personale docente. Il flusso di informazioni, che dovrebbe avvenire tra SIDI (il sistema informatizzato del MIUR) e l'Inps secondo un ordine di priorità e tenendo conto dell'effettiva disponibilità dei posti destinati alla mobilità, avviene non rispettando una cronologia logica e conseguenziale, tanto che l'Inps dovrebbe riuscire a comunicare al MIUR i dati riferiti ai pensionamenti del personale docente in anticipo rispetto alla scadenza della presentazione delle domande di mobilità e, conseguentemente, prima che il SIDI venga chiuso. Ciò permetterebbe ai docenti di venire a conoscenza in tempo utile dei posti realmente disponibili ai fini della mobilità. Ciò non avviene, in quanto le pratiche dei pensionamenti vanno lavorate successivamente alla presentazione delle domande in mobilità. Dovremo ancora semplificare, ma questo Governo preferisce non occuparsi Come si potrà porre in essere questa riforma di importanza epocale se non vi è la minima attenzione a queste problematiche? Pertanto sembrerebbe che, rispetto al Governo Conte, nulla sia cambiato. A tale scopo, sempre per garantire e assicurare le pari opportunità, non è stata presa in considerazione la costruzione delle mense scolastiche al Sud. A fornire un servizio alla famiglia, non sono solo gli asili nido. Le mense scolastiche permetterebbero tempo pieno a scuola, studio assistito, doposcuola didattico personalizzato, aumento dell'occupazione femminile, migliore organizzazione dei tempi lavoro famiglia. Per quanto riguarda le infrastrutture, il ponte sullo Stretto è stato assolutamente dimenticato. Suggerirei un nome: Penelope. Penelope tesseva e disfaceva la tela, così come è stato per il ponte sullo Stretto. La tela tessuta era di 3.300 metri, metri, ma il Governo Monti ha provveduto a disfare la tela. Adesso si potrebbe rimediare e si potrebbe nuovamente permettere questa tessitura definitiva. Quindi, il ponte sullo Stretto Penelope "s'ha da fare". Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, Governo, colleghe e colleghi, qualcuno diceva che l'ottimo è nemico del bene ed è ciò che continuo a ripetermi da qualche ora dopo aver letto l'ultima bozza del PNRR. non c'è campanilismo, né interesse di parte o sguardo viziato in quanto mi accingo a dire. Il mio giudizio, infatti, nasce a valle di un confronto impegnativo, irrobustito dalle considerazioni emerse con l'audizione di oltre 300 soggetti che diversamente operano nel Paese. Ho voluto audire fortemente tali soggetti in Commissione nelle diverse fasi che hanno accompagnano la redazione di questo PNRR, considerato come un'opportunità, forse l'unica, per avviare un percorso di ripartenza che ci consenta di superare antiche fragilità che la pandemia ha messo in evidenza, ma anche nuove debolezze. Ciò premesso, sono consapevole che sia un punto di caduta significativo leggere nero su bianco alla pagina 11 di questo documento che il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili del Piano sono destinate al Mezzogiorno, "scollinando" così la percentuale del 34 per cento legata alla mera popolazione residente. Tuttavia, non credo basti perché i parametri adottati dall'UE per assegnarci il 25 per cento della dotazione complessiva, come è noto a tutti, erano e restano tre: popolazione residente, PIL *pro capite* e tasso di occupazione. Su questi tre parametri il Sud, con le sue storiche criticità, purtroppo ha trainato in negativo il saldo della valutazione, facendoci assegnare questa quota così importante. cento non è, quindi, una vittoria, tantomeno un traguardo; è semmai l'*incipit* - per questo ringrazio sinceramente il ministro Carfagna - di una nuova e ritrovata consapevolezza nel dover procedere a una vera e propria inversione di rotta

problema lo riscontro nella difficoltà o, quasi, nell'impossibilità di veder declinato quell'impegno anche nelle successive 300 pagine, a partire proprio dalla missione che territorialmente è la più significativa, ossia quella delle infrastrutture. in questa missione all'Alta velocità per il Sud viene assegnata una dotazione finanziaria pari alla metà dei fondi destinati al Nord, con l'esclusione radicale, tra l'altro, della dorsale adriatica da questo acceleratore della crescita. Sapevo fin dall'inizio - e l'ho detto in tutte le salse in quest'Aula - che il concetto di cantierabilità stringente che l'Unione europea ci introduceva rischiava di tradursi per il Mezzogiorno in una sorta di beffa, ma evidentemente non è bastato. Così come non basta, signor Presidente, che l'*upgrade* da PNRR per l'Alta velocità nel Mezzogiorno si traduca nei previsti 100 chilometri all'ora per la Palermo-Catania o, ancora, nelle tre ore necessarie per percorrere i 300 chilometri

oggettivi e fanno emergere in maniera evidente come la dicitura relativa all'investimento 1.2, ossia - cito testualmente - «Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa», sottolinei una distanza siderale e per questo forse incolmabile rispetto al Sud. Le cifre per la prima indicano uno stanziamento di 8,57 miliardi, mentre per il Sud di 4,64. Numeri, laddove è stato possibile rilevarli, che non possono non destare le preoccupazioni di un intero Mezzogiorno che guarda a questo passaggio come un'occasione storica: 550 sindaci ci hanno sottoposto un appello. Se, poi, a queste cifre aggiungiamo alcune piegature - mi passi il termine - allora la preoccupazione di essere all'altezza di questa responsabilità e delle aspettative rischia di cadere nella rassegnazione. Mi riferisco nello specifico all'investimento 1.6 a favore delle linee ferroviarie regionali, in particolare nel Mezzogiorno, salvo poi andare a pagina 212 e leggere, a valere sulla stessa dotazione, il finanziamento della linea canavesana, della ferrovia Torino-Ceres, della Sansepolcro-Terni: tratte che nessuno potrà mai convincermi appartengano a quel Sud Italia che continua a patire più di altri ritardi e *deficit* di infrastrutture e servizi. Allo stesso modo, nessuno potrà mai convincermi della bontà di una scelta anche questa politica - confermata in questo Piano, come nel precedente, che nel quadro dei porti consegna solo a Genova e Trieste la centralità di investimenti robusti strategici, discriminando il sistema portuale del Sud Italia, che invece dovrebbe vederci tutti insieme nell'investimento geostrategico che la piattaforma del triangolo Napoli-Taranto-Gioia Tauro naturalmente ci consegna, e consegna al Paese, non al Mezzogiorno. E allora, sia ben chiaro, Presidente - e lo voglio ripetere ancora -: le mie non sono rivendicazioni di campanile, ma il richiamo a un dovere politico a cui tutti ci dobbiamo sentire impegnati, se vogliamo davvero "ricucire" un Paese piegato a metà. a metà. Per stare a un altro esempio evidente, credo personalmente che l'alta velocità debba essere un diritto universale, al Sud come al Nord; che raggiungere Roma da Lecce debba avere lo stesso valore, quindi la stessa accessibilità, che farlo da Firenze o da Milano. Non è più tollerabile avere due Paesi in uno. *(Applausi).* Per questo, Presidente, in questo luogo, con la responsabilità che sento nel continuare a sostenere questo Governo in passaggi significativi, ho il dovere di chiederle senza filtri un impegno chiaro ad aprire sin da ora un set di paracadute per il nostro Mezzogiorno. Lo ripeterò fino a rischiare di sembrare ossessivo: il requisito della cantierabilità non può essere l'alibi per tradire un impegno che anche l'Europa ci ha chiesto. *(Applausi)*. Un'altra grande preoccupazione mi assale: se l'individuazione degli investimenti per le infrastrutture è stata fortemente condizionata dal criterio dell'immediata cantierabilità, per cui i primi continueranno a essere primi, non vorrei che, in una logica perversa di premio a chi è più pronto, a chi è più attrezzato, a chi ha più organizzazione, anche le risorse destinate alle altre missioni e agli altri obiettivi strategici vengano assorbite - diciamo così - con maggiore rapidità e consistenza dalle amministrazioni più grandi e più attrezzate. Qui c'è tutto un tema che investe, ad esempio, le città intermedie, che sono un pezzo importante del Paese, che non possono restare in una sorta di limbo, strette tra le città metropolitane e le aree interne. La prova del nove l'avremo con il bando sugli asili nido: scade il 21 maggio senza che in esso sia stata indicata alcuna quota riservata al Sud, dove c'è la maggiore deficienza, presentando, anzi, modalità che, a mio avviso, favoriranno chi è più avanti, chi ha un'organizzazione amministrativa più strutturata. Ecco perché, allora, Presidente, le chiedo alcuni impegni, e vado a concludere. è quello di riprogrammare da subito le risorse rivenienti dalla sostituzione del finanziamento delle opere infrastrutturali con i fondi di cui al PNRR secondo il rispetto del vincolo territoriale originario

Le chiedo ancora, signor Presidente, di inserire entro i prossimi tre mesi i progetti espunti dal Piano in ragione dei criteri di tempo e di cantierabilità, come l'estensione dell'Alta velocità lungo tutta la dorsale adriatica, nella programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione e nelle relative linee di finanziamento, nonché di rivedere nell'immediato il contratto di programma con RFI per la parte investimenti, per portare

ma non smetterò mai di combattere questa battaglia. Lo devo alla mia terra e lo devo anche un po' ai miei figli. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, se dovessi elencare i motivi per i quali apprezzo pienamente il PNRR da lei presentato, i quattro minuti a mia disposizione non basterebbero. Parlerò allora non del corpo del Piano, ma della sua anima, le riforme, su cui ha detto parole importanti. Qualche giorno fa, con un piccolo gruppo di quindicenni, parlavo del PNRR e spiegavo loro che questo è un piano che l'Europa e l'Italia stanno facendo per loro.

primo luogo, le riforme sono quelle riparazioni al motore dell'economia e della società italiane, necessarie per trasformare i soldi europei in crescita, in lavoro e in riduzione delle inequità e degli squilibri. secondo luogo, se quelle riparazioni non saranno fatte, i soldi europei non arriveranno proprio. In terzo luogo, anche senza i soldi europei, in realtà quelle riforme andrebbero fatte, se vogliamo andare avanti come Paese. Le riforme in Italia devono farle gli italiani e non c'è scorciatoia: il Governo, il Parlamento, i cittadini e le imprese. Ogni riforma però è scomoda, costa sacrifici a qualcuno, soprattutto quelle legate alla concorrenza e costa voti. Ci vuole una spinta. Non basta credere, se ci si crede, che il futuro sarà migliore per tutti - più crescita e più equità - una volta fatte le riforme, ma ci vuole una spinta. Essa può venire dall'interno, ovvero dalla lenta evoluzione della mentalità e della cultura politica, economica e civile o può venire dall'esterno, in particolare dall'Europa e dai mercati. L'Italia, se guardiamo indietro, di solito ha fatto riforme in connessione con l'Europa: nel 1996-1997 con un grosso miraggio, ovvero l'ingresso nell'euro, nel 2011-2012 con una grossa pressione dell'Europa e dei mercati. Da qualche anno, mi riferisco comunque a prima della pandemia, l'Europa ha tenuto un atteggiamento accomodante nei controlli sulle finanze pubbliche dei Paesi e nella politica monetaria. In Europa, non solo in Italia, da qualche anno le riforme sono ferme, non si sono più fatte e sono iniziate le controriforme. Anche in quest'Aula, negli anni scorsi, ne siamo stati testimoni. Cioè rispetto a una moderna economia sociale di mercato si sono fatti passi indietro e oggi, anche sotto l'impatto della pandemia - ho quasi concluso, signora Presidente - ci si sta sempre di più

Mi permetterei però di raccomandarle, visto che in questo momento dobbiamo evitare arretramenti nella mentalità e nella cultura e, se possibile, andare avanti...

il Piano nazionale di ripresa e resilienza è solo una parte, certamente molto importante, di una più ampia e ambiziosa strategia per l'ammodernamento del nostro Paese, che sarà completo, se noi sapremo coniugare capacità progettuale e concretezza con l'immaginazione e la creatività. Io aggiungo che sarà completo, se sapremo anche restituire con generosità e senso di appartenenza alla comunità italiana quanto abbiamo tolto indebitamente a chi non aveva colpa, se non di essere nato in un periodo sfortunato. Dovremmo in qualche modo favorire, senza una competizione forte che non aiuta, l'ibridazione tra Nord e Sud - sono due culture nettamente differenti tra aree urbane e aree interne, tra competenze scientifiche e competenze artistiche e letterarie, tra giovani e meno giovani e - io dico anche - tra chi ha più meriti, perché con fatica e sacrifici è riuscito a conquistare competenze, magari non così specialistiche, e chi ha più competenze verticali e specialistiche, ma meno meriti, perché si è trovato in una condizione più favorevole ai nastri

storia di riscatto con grande orgoglio, quell'orgoglio italiano che ha fatto grande il nostro Paese, soprattutto se pensiamo al ventennio della grande crescita economica, quella dagli anni Cinquanta al 1973. Dico questo perché dobbiamo dare a molti

sulle misure volte a eliminare le restrizioni alla concorrenza per favorire la crescita economica e l'equità. Tutto quello che favorisce il gioco competitivo non può che essere accolto favorevolmente. Cosa ben diversa, però, presidente Draghi, è la declinazione di queste misure su altri settori, quelli che io considero un po' meno strategici, anche se sono molto importanti per il PIL del nostro Paese. Sono strategici i porti, la logistica, l'energia, le reti digitali - questo sì - e non bisogna assolutamente impedire misure che favoriscano

e, come lei dice, anche l'impostazione di filiere. Mi è piaciuto molto questo termine in luogo di quello di imprese, perché solo attraverso la creazione di filiere e quel cuscinetto che costituisce

Pochi minuti di intervento, gentile presidente Draghi, che per me sono un onore e una possibilità più unica che rara. La seguo da sempre perché chi, come lei, ha ricoperto ruoli istituzionali di grande importanza per meriti e fatiche personali ha una visione sicuramente più più profonda e scevra dagli impoverimenti della semplice logica politica. Citerò quattro sue dichiarazioni che sembrerebbero rilasciate recentemente, tanto sono attuali rispetto al contesto che stiamo purtroppo vivendo che invece sono di dieci anni fa e testimoniano dolorosamente l'immobilismo che avvolge il Paese Italia. La prima dichiarazione è in un'intervista al «The Wall Street Journal» del 2012 nella quale dichiara che nel nostro impianto istituzionale i livelli di rapporto debito-PIL sono eccessivi. Non ci sono alternative al consolidamento fiscale, che non dobbiamo negare avere un effetto recessivo nel breve termine, ma in futuro, attraverso il cosiddetto canale della fiducia, la crescita economica verrà riattivata». Una *austerity* buona è quando si riducono le tasse, e la spesa pubblica la si concentra sulle infrastrutture e sugli altri investimenti. La seconda riguarda una lettera della BCE al Governo italiano nel 2011: «È necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali». La terza dichiarazione è tra le Considerazioni finali da Governatore della Banca d'Italia «L'Italia è indietro nella dotazione di infrastrutture rispetto agli altri principali Paesi europei, pur con una spesa pubblica che dagli anni Ottanta è stata maggiore in rapporto al PIL». è contenuta nelle Considerazioni finali da Governatore della Banca d'Italia: «La scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro è un fattore cruciale di debolezza del sistema». «Il tempo di cura della casa e della famiglia a carico delle donne resta in Italia molto maggiore che negli altri Paesi». se hanno chiesto il suo autorevole aiuto per riuscire a tenere la barra dritta - come si suol dire dalle mie parti - di un'Italia alla deriva, mi sembra ora più che evidente. Questa Italia, signor Presidente, è ferma da tempo e necessita di tutto e di più; e lo strumento del PNRR può essere riconosciuto come un volano di ripresa e non solo di ulteriore indebitamento. Ma è bene ricordarci, in merito alle riforme ormai indispensabili per attivare il complesso sistema del PNRR, che il gioco della camera di compensazione delle diatribe politiche non deve assolutamente riaccendersi. Le riforme e cito quelle che sono maggiormente attenzionate, ossia pubblica amministrazione, fisco, giustizia, procedura semplificata per i lavori pubblici - non devono trovarsi sui tavoli infiniti delle Commissioni, con plichi di emendamenti prioritari, ammissibili, supersegnalati, senza relazione tecnica, testo 2, testo 3, testo 4 e via dicendo.

introdurre anche un approccio di metodologia legislativa più innovativa, più semplice e snella. Fare riforme con le stesse tempistiche a cui siamo abituati da decenni è ormai impensabile. Lo scatto di orgoglio, di autentica e convinta ripresa, a cui gli italiani vogliono credere fermamente, deve trovare in questo Parlamento e in questo Governo un alleato principe, un pilastro su cui poggiare con sicurezza le scelte che verranno operate. In difetto, si fermerebbe il processo di trasformazione richiestoci da più parti e da sempre rimandato. Un Paese come il nostro, allo stremo, non reggerebbe più. Le sue parole all'Europa di pochi giorni fa - garantisco io - risuonano nella mente di tutti noi: ci sta tutta la sua autorevole fermezza, ma anche la sua preoccupazione, a cui umilmente associo la mia personale

privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza. Questa è la vera sfida che non dobbiamo perdere. Abbiamo la forza, abbiamo gli strumenti, abbiamo il coraggio e quella straordinaria capacità di reinventarci anche dopo essere caduti; facciamo buon uso di queste preziose capacità e di questa occasione. Grazie per la sua attenzione. Grazie

un Piano - quello di cui discutiamo oggi - frutto anche dell'impegno del precedente governo Conte, grazie al quale l'Italia è la prima a beneficiare in valore assoluto - dobbiamo ricordarlo - dei fondi del programma Next Generation EU. Oggi, grazie a lei, dobbiamo concretizzare i nostri progetti per rilanciare l'Italia. Il PNRR deve essere lo strumento attraverso il quale si riducono le disuguaglianze, la povertà e l'esclusione sociale, tutti fattori, purtroppo, che sono endemici nella nostra società. Deve essere lo strumento che permetterà al Paese di essere accompagnato in quel piano di riforme strutturali che aspettiamo da tempo. Più diritti ai giovani a chi vive nei territori più svantaggiati del Paese. A proposito del tema Sud, la percentuale del 40 per cento di risorse nel PNRR, che equivale a circa 83 miliardi destinati al Sud, è certamente un primo passo. il fatto che da questa cifra sia stato escluso, come lei ha detto, il React EU, uno strumento autonomo che assegna al Sud 8,4 miliardi, così come il Fondo sviluppo e coesione, che insieme non contribuiscono a determinare quel 40 per cento. Ma occorre fare di più. Oggi 500 sindaci del Sud hanno richiesto perequazione. Desidero, da donna del Sud, un Sud connesso con il resto del Paese, che attragga investimenti, che valorizzi le bellezze del nostro territorio e dei nostri mari, prevedendo impianti di depurazione delle acque reflue. Vorrei un'intensificazione dei trasporti. Il Sud ha una serie di potenzialità: sfruttiamole e cogliamo questa opportunità, superiamo le differenze, coinvolgiamo tutti gli attori della società e provvediamo a questo rilancio. Confido nella sua sensibilità per quanto riguarda la particolare attenzione rivolta alle donne e all'imprenditoria femminile, garantendo maggiori investimenti, ma anche maggiori servizi, proprio perché la donna non deve trovarsi di fronte alla scelta lavoro o famiglia. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, abbiamo sempre sentito parlare di svecchiamento della pubblica amministrazione.

si parla ancora di preselezioni per titoli ed esperienza, ma questi giovani avranno la possibilità di lavorare? Riserviamo i titoli e l'esperienza a quei concorsi in cui siano richieste determinate competenze. parliamo di giustizia e della necessità di accelerare i processi, proprio perché l'Italia diventi più competitiva anche da un punto di vista economico e possa attrarre investitori europei.

la magistratura ordinaria, proprio perché senza le risorse umane non si va da nessuna parte. Mi auguro che ci siano la digitalizzazione e l'innovazione attese, attese, che, nella maniera più semplice, potranno essere realizzate dai giovani, che in questo modo riusciranno a rendere anche più semplice la vita ai cittadini.

a tutti i settori, alle ASL e agli ospedali, in modo che la tutela della salute di ciascun individuo non sia soltanto qualcosa di aleatorio, ma possa diventare una questione cui, in qualsiasi momento, utilizzando il fascicolo elettronico, si possa comprendere la situazione del paziente. Sono anche molto contenta che abbia parlato di

però, al di là di errori formali (che io condivido), bisogna pure che gli amministratori del Sud imparino a usare le risorse. *(Applausi)*. Basta leggere la relazione della Corte dei conti del 2019.

e chi, invece, come me, pensa che le riforme sarebbero necessarie anche senza soldi, anche se non ci fossero, e da tanto, tanto tempo.

ancora un minuto. Walter De Benedetto è affetto da artrite reumatoide; l'unica cosa che gli dà sollievo sono i cannabinoidi, che sono legali nel nostro Paese. Lui ha una ricetta, ma se ne può fare carta straccia, perché i cannabinoidi non ci sono. Noi ne produciamo troppo pochi e li importiamo dall'Olanda con il contagocce, quindi sottoponiamo "i Walter" del nostro Paese una tortura inutile e inumana. Oggi è stato prosciolto, ma il suo amico che lo aiutava a coltivare è stato invece incolpato. Capisce la mobilitazione della polizia, giudici, avvocati, tutto l'ambaradan possibile e immaginabile per un processo grottesco.

presidente del Consiglio Draghi, Ministri, colleghi, il tema di cui oggi discutiamo ha una rilevanza talmente tanto grande da rendere superfluo il sottolinearla; d'altra parte, però, probabilmente non sarà mai abbastanza, alla luce dello sforzo che nei prossimi anni si chiederà agli italiani per ripagare il debito. Consiglio ha ragione quando dice che questo Piano contiene le vite degli italiani, le nostre ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini che verranno; vi sono dentro i sentimenti della nostra comunità nazionale, che nessun numero o tabella potranno mai rappresentare. Purtroppo il nostro Paese era in sofferenza già da prima dell'epidemia, come emerge dai dati citati anche dal Presidente del Consiglio. Ora è il momento di riconoscere le potenzialità, di cogliere le opportunità legate alle evoluzioni nei diversi settori, soprattutto riguardo al mondo del digitale. ha affermato che la tecnologia è un modo per garantire a tutti eque opportunità ed è fondamentale adottarla sfruttandola al meglio ad ogni livello.

Il pilastro dell'inclusione sociale deve essere una vera e propria missione, dove impiegare tutte le nostre energie, volontà e visione politica. Ripartiamo, signor Presidente del Consiglio, ma con ben chiaro un concetto fondamentale: se vince il Sud, vince l'Italia intera. È un limite continuare a pensare alle Regioni del Mezzogiorno come a un problema da gestire. Il Sud è agricoltura, patrimonio storico-culturale, turismo, sostenibilità ambientale. Il Sud è negli occhi che trasmettono tenacia e nelle spalle larghe e forti delle tante donne e dei tanti uomini che non si arrendono. Il Sud, signor Presidente del Consiglio, è una risorsa da valorizzare e promuovere al meglio delle nostre capacità ed è questo il paradigma che dovremmo adottare. Dobbiamo invertire il *trend* per cui bisogna lasciare le Regioni del Mezzogiorno per trovare opportunità lavorative. Il momento per cambiare paradigma d'azione è ora. Bisogna cercare di trattenere i giovani creando sviluppo. Occorre quindi investire in infrastrutture, collegamenti per persone e scambi di merci. A tal riguardo sono opere strategiche il completamento dell'autostrada A2 e l'estensione dell'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria - già citata dai miei colleghi primi lotti sono inclusi nel PNRR. I cittadini si aspettano l'Alta velocità su tutta la linea Salerno-Reggio Calabria. Auspico quindi un'accelerazione sull'intera progettualità,

Garantendo una velocizzazione dei trasporti, si renderebbe più semplice potenziare i comparti strategici, tra cui l'agricoltura. Dobbiamo mettere in campo azioni concrete, comprendere che la ripresa e la resilienza sono legate al denaro europeo. Al fine di concretizzare la ripartenza è fondamentale difendere e tutelare i nostri comparti strategici. Penso al *made in Italy,* seriamente minacciato da sistemi come il *nutri-score.* Il PNRR è solo una delle tante opportunità che arriveranno nel prossimo futuro. Attenzione però: non abbiamo tempo, e ricordiamo che oggi, con le procedure vigenti, le opere infrastrutturali con un costo superiore a 100 milioni hanno un tempo di realizzazione di circa sedici anni; così facendo riusciremo a spendere solo il 48 per cento delle risorse del PNRR. Alla luce di ciò le chiedo un percorso di sburocratizzazione, un vero e proprio snellimento. Signor Presidente, onorevoli colleghi e Governo, il Piano di ripresa e resilienza, pensato per guarire le profonde ferite inferte dallo tsunami pandemico, è un programma integrato di interventi per migliorare il quadro socio-economico attuale, investendo in riforme strutturali e in un chiaro e puntuale progetto per il futuro. Ora occorrerà dargli un cuore vibrante, iniettare linfa vitale nei nodi nevralgici: salute, ambiente, cultura, solidarietà, sicurezza del territorio, giovani, donne e Sud. Ora dobbiamo attuarlo, valorizzando tutte le competenze scientifiche, tecniche e professionali del nostro Paese. È anche il momento epocale di ripensare con coraggio allo sviluppo economico, transitando da obsoleti modelli dominati da un distorto concetto di PIL ad un futuro ecosostenibile. Bob Kennedy oltre mezzo secolo fa disse che «il PIL misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta». Penso sia giunto il momento di attuare un cambio di paradigma socio-economico e avviarci sulla strada del progresso autentico, garantendo ad ogni singolo italiano che gli investimenti per la ripresa e la resilienza, che ci accingiamo a realizzare, tenderanno alla qualità della vita, all'equità sociale intergenerazionale e all'ecosostenibilità. Penso alla necessità di ridare speranza ai giovani, ulteriormente ridotta con la pandemia; agevolare il lavoro femminile, falcidiato dalla crisi pandemica; garantire il diritto di tutti - sono compresi anche i nostri fratelli non ancora esistenti - a fruire di un ambiente bello e vivibile. Nel Piano in esame, per ciò che concerne la tutela del territorio, sottolineo il recepimento delle osservazioni fatte dal Senato al precedente sia sulla necessità di creare un'efficiente *governance* per la transizione ecologica, sia sul sistema della conoscenza e tutela ambientale. Molto pregevoli i nuovi investimenti previsti per il monitoraggio e la previsione degli effetti del cambiamento climatico, la rinaturalizzazione di aree del Po, la bonifica dei siti inquinati orfani, ripristino e la tutela dei fondali e degli *habitat* marini, la digitalizzazione dei parchi naturali. Devo però constatare che il parere del Senato sulla necessità di aumentare i finanziamenti per la prevenzione dei rischi naturali è stato disatteso; anzi, per il contrasto al dissesto idrogeologico c'è una decurtazione: saranno investiti solo 2,5 miliardi, l'equivalente dei danni attesi in un solo anno. Così facendo accumuleremo debito ambientale e tragedie. Ridurre, mitigare e prevenire gli elevati rischi naturali di un Paese geologicamente fragile non è un inutile fardello; 22 milioni di italiani vivono in aree ad elevato rischio sismico e 8 milioni sono esposti al rischio idrogeologico. Le ultime tre ricostruzioni post-sisma sono costate 40 miliardi, l'equivalente dell'adeguamento sismico di tutti gli edifici pubblici italiani. La ricostruzione costa dieci volte di più della prevenzione, oltre alle calamità sociali. Il dissesto idrogeologico causa in media danni per 2 miliardi e mezzo l'anno; prevenirlo costa cinque volte di meno ed evita catastrofi. Auspico che in un futuro molto prossimo si possa sciogliere il nodo gordiano della sicurezza del territorio, fondamento per la tranquillità di un popolo e per lo sviluppo ecosostenibile e duraturo della Nazione. Penso, che oramai occorra superare perfino il concetto di salvaguardia, tutela e custodia dell'ambiente. Dobbiamo volare verso il futuro, bonificando, rinaturalizzando e migliorando l'ambiente e il paesaggio. Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza dobbiamo spalancare le porte al futuro, rendendo la vita veramente degna di essere vissuta.

scritta da qualcun altro, perché si parte dicendo che la pandemia ha colto il nostro Paese in una fase di fragilità economica e sociale, con un calo degli investimenti che ormai durava da decenni, come se le letterine arrivate da Bruxelles non fossero state firmate dal presidente Draghi e scritte dall'attuale ministro Franco; come se la cura Monti non ci fosse stata prescritta, perché non è stata voluta. È per questo che il nostro Paese è arrivato in una fase di così grave fragilità ad affrontare la pandemia. Ma l'anima di questo Piano dovrebbe essere proprio la riforma fiscale, che è quella chiave. Voi scrivete che è quella su cui poggia il rilancio del nostro Paese, sono dedicate soltanto alcune righe nel testo, perché di fatto non potete fare nulla e lo stesso presidente Draghi lo ha detto alla Camera: ci vorrebbe una forte volontà politica. Eppure, avrei voluto sapere se il disegno di legge delega partirà dalle intenzioni dell'espertissimo Brunetta o del competente Garavaglia, che avevano coperture per 270 miliardi per la *flat tax* o con la massimizzazione della progressività richiesta da lei. Sarebbe interessante che il Parlamento sapesse dove volete andare a tagliare, se le imposte dirette

Un'altra questione che voglio affrontare è quella del Sud, perché lei gongolante ha detto che avete destinato il 40 per cento delle risorse al Sud. Ebbene, sono poche e il Governo dei migliori avrebbe dovuto osservare i criteri dell'Unione europea, che dicono ben altro, ossia che, se fossero stati osservati quei criteri soltanto

che percorriate la Jonica e ancora ci volete rifilare la Napoli-Bari, che era già interamente finanziata, tra fondi nazionali e fondi europei. Vorrei capire se state sostituendo i fondi ancora una volta per il Sud, perché di questo si sta parlando. Avete già iniziato con l'agricoltura, scippando una parte di quote dei fondi europei. Vorrei anche parlarvi dell'audacia che dovrebbe avere questo Governo, perché la grande opportunità dei fondi europei potrebbe risolvere la grande questione dell'ex Ilva. Abbiamo il grande Ministero della transizione ecologica, ma abbiamo un Ministro della sanità che non si occupa della salute di quel territorio; abbiamo un Ministro che già parla di compromessi. Voglio sapere quanti morti sono il rischio ragionato per mantenere ancora l'acciaieria; quanti malati oncologici pediatrici ancora sono il rischio ragionato per Taranto, che si trova a muoversi ancora in una bolla con l'impunità penale. Queste sono le risposte che al Paese dovreste finalmente dare e non le lezioncine con l'*excursus* storico*,* che va dal 1950 al 1973, dimenticando che dopo sono arrivati i Berlusconi, i Craxi, i D'Alema e i Prodi e nella classe dirigente, caro presidente Draghi, di quegli anni in cui si sono diminuiti gli investimenti, c'era proprio

Signor Presidente, vedo che in buona sostanza questo Paese rimane sempre lo stesso, non fa quel passo in avanti che dovrebbe fare ed è ancora

e rassicurare l'Europa sulle cosiddette riforme orizzontali o di contesto, di cui la giustizia è un punto centrale. Non a caso, siamo stati fermi tutti questi anni perché sulla giustizia non abbiamo potuto

Dico questo perché la questione giustizia è diventata centrale in quanto siamo un Paese che spende più di tutti gli altri per il mantenimento dell'accusa

presente il Ministro della giustizia, che tra l'altro ringrazio anche per il bellissimo discorso che ha fatto domenica nella sua intervista

che vivrà non solo di porto, ma anche della capacità di essere connessa con il resto d'Europa. I Paesi di Visegrád si stanno unificando nell'Alta velocità, mentre noi resteremo fuori. Attenti a questo...

oggi è un giorno importantissimo per l'Italia perché discutiamo del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di uno strumento che potrà consentire al nostro Paese di uscire dalle secche di una crisi economica senza precedenti conseguente alla pandemia e potrà consentirci di ovviare a storture e lacune del nostro sistema che ci trasciniamo dietro da decenni. Si tratta di un giorno importante e ci sarebbe molto piaciuto che a illustrare il PNRR fosse stato Giuseppe Conte, perché la nascita del Piano nazionale è ascrivibile a lui e alla maggioranza che lo ha sostenuto per tutto il 2020 e in cui ebbe un ruolo decisivo il MoVimento 5 Stelle. Tutto nacque dalla lettera scritta da Conte il 25 marzo 2020, capace di riunire attorno a sé e all'Italia i Governi di altri 8 Paesi e di produrre uno sconvolgimento nelle politiche europee di *austerity*, che lei ben conosce, presidente Draghi.

o BEI. Colleghi, mi viene davvero da sorridere per non piangere ripensando a chi, in quest'Aula, spacciava per salvifico uno strumento miope e di fatto condannato come inefficace dalla storia delle recenti crisi finanziarie. Conte e gli altri otto *leader* europei chiedevano più risorse finanziate da debito comune europeo. Da quel 25 marzo, si è innescato in Europa un dibattito che, a fine luglio 2020, ha finalmente portato alla nascita del *recovery fund* da 750 miliardi. Il Piano nazionale, quindi, è un risultato conseguito dal Governo Conte 2, confermato dall'attuale Esecutivo al 100 per cento nelle sue missioni e nella sua struttura. Altro che discontinuità; tra l'altro, non avrebbe potuto essere diversamente. Il Piano e lo sforzo compiuto dal Governo Conte 2 per farlo digerire ai Paesi cosiddetti frugali andranno anche apprezzati per la loro eredità politica, culturale ed economica, perché non c'è dubbio che, ancora oggi, il cammino per il cambiamento dell'Unione europea sia tutt'altro che compiuto. È, però, parimenti indiscutibile che qualcosa di epocale e di irreversibile sia avvenuto: l'emissione di titoli di debito comune, la sospensione del Patto di stabilità, gli stimoli monetari espansivi della BCE sono una vera e propria rivoluzione. Intorno a questi cambiamenti si sta sviluppando in Europa un dibattito che, giustamente, chiede di ampliare la carica di cambiamento che la pandemia si è portata dietro. proprio in questi giorni tornano a chiedere lo smantellamento di parametri anacronistici e senza alcuna base scientifica, come il 3 per cento del rapporto *deficit*-PIL o il 60 del rapporto debito-Pil, se tutto questo sta avvenendo, vuol dire che noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo reso fertile il terreno del cambiamento e i suoi frutti germoglieranno e cresceranno sempre di più, perché queste idee cammineranno sulle nostre gambe. Ci sarebbe molto piaciuto discutere e analizzare il Piano nazionale in tempi più congrui, pur rendendoci conto della vastità e della complessità dell'operazione. Per questo motivo, abbiamo chiesto e pretenderemo di essere costantemente informati dello stato di avanzamento dei progetti e del conseguimento degli obiettivi. La responsabilità di questi tempi ristretti è ascrivibile alle spregiudicate operazioni politiche messe in essere dal mandatario Matteo Renzi e dalla crisi governativa da lui innescata. Diceva di voler a tutti i costi il MES e ora non serve più; diceva di voler più tempo per esaminare e scrivere il Piano nazionale e, invece, ha ottenuto il risultato contrario: davvero complimenti! Io aggiungo che in questo Piano nazionale di ripresa e resilienza, il 40 assegnato al Sud e questo è soltanto il primo passo di un cambio di paradigma davvero necessario. Quindi, noi ci auguriamo che questo 40 per cento quanto prima possa aumentare proprio per colmare quel *gap* che esiste tra Nord e Sud. Se riparte il Sud, riparte tutta l'Italia.

Presidente, lei ha detto che la missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, è particolarmente importante, perché l'Italia è maggiormente esposta ai rischi climatici rispetto ad altri Paesi. Ha ragione, perché l'Italia è una penisola con 8500 chilometri di coste estremamente fragili e ha la più alta biodiversità europea, purtroppo compromessa, oltre ad un avanzato dissesto idrogeologico a causa di un ambiente naturale altamente antropizzato. La risoluzione approvata dal Senato sulla precedente versione del Piano conteneva una serie di proposte a favore della biodiversità terrestre e marina, con un impegno stimato di circa 4 miliardi di euro, ovvero meno del 2 per cento del *budget* del *recovery*. Eppure, il Governo ha disatteso gli impegni assunti. Ce lo ricorda oggi anche la Lipu, che ha avviato un'interlocuzione con la Commissione europea per la parziale revisione del Piano, affinché si inserisca ciò che ha chiesto il Parlamento. La nostra è una transizione non ecologica, ma piuttosto energetica o, meglio, il rafforzamento di uno *status* di *lobby* che fanno fatica a cambiare paradigma, come ci ha ricordato oggi ENI in audizione. Inoltre, il Piano finanzia la produzione di energia bruciando rifiuti agricoli e scarti alimentari, che sono risorse. Non si parla di agroecologia per la conservazione dei servizi ecosistemici del suolo agricolo o di sostenibilità della zootecnia. Al contrario, si sostiene lo sviluppo del biometano ottenuto da recupero energetico dei residui organici con un importo di 2 miliardi di euro: un debito che sarà spalmato sulle prossime generazioni insieme all'aumento della temperatura. Si finanzia la realizzazione di imponenti opere infrastrutturali, di comunicazione e trasporti, di energia, anche rinnovabile (sia in mare che a terra), senza una pianificazione, ma con un decreto semplificazione che ambientale (VIA). Noi vogliamo il progresso, ma non vogliamo più investire il futuro dei nostri figli su un uso indiscriminato del territorio e su fonti energetiche che utilizzano ancora la combustione. Nell'ultima versione del *recovery* c'è un'importante novità e di questa sono contenta. Il mare ha ora un suo spazio nel Piano con un investimento di 400 milioni di euro a favore della biodiversità marina, del ripristino degli ecosistemi degradati e della loro tutela su larga scala, preordinato - si spera - alla creazione anche di aree marine protette. Serve invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi, potenziandone la resilienza ai cambiamenti climatici e favorendone il mantenimento e la sostenibilità di attività fondamentali non solo per le aree costiere, ma anche per le altre filiere produttive marine. Sono contenta che si intenda, inoltre, potenziare il sistema della ricerca italiana sul mare, la dotazione di navi oceanografiche gestite dallo Stato attraverso un'Agenzia nazionale, ma in generale questo Piano disattende...

fino a qualche mese fa ho temuto che l'opportunità rappresentata dal *recovery* andasse sprecata perché gestita con una visione di Paese che non condividevo, incentrata sull'assistenzialismo e sullo statalismo, che molti danni avrebbero potuto recare alla nostra economia.

ci siamo confrontati negli ultimi mesi di lavoro parlamentare. Abbiamo sempre creduto nella necessità di avviare una grande stagione di riforme per far ripartire il Paese. Semplificare le procedure per la realizzazione delle infrastrutture, svecchiare la pubblica amministrazione, dotarsi di un sistema della giustizia più veloce e giusto, riformare il fisco alleggerendo il carico su famiglie, lavoratori e imprese saranno il presupposto essenziale per godere a pieno dell'opportunità che ci offre l'Europa. Tanti sono gli obiettivi del Piano, ma ve ne è uno che mi sta particolarmente a cuore, ovvero il rilancio del Sud. Gli investimenti messi in campo dovranno servire ad affermare un principio semplice, ma sacrosanto: ogni cittadino italiano deve avere le medesime possibilità, poter rivendicare gli stessi diritti e usufruire degli stessi servizi da Pantelleria a Bolzano. Complessivamente il Sud potrà contare su una mole di risorse senza precedenti. Presidente, come ha detto anche lei, si porterà avanti un lavoro corale. Per cui, il confronto con le amministrazioni locali dovrà essere costante. Nel Meridione c'è davvero tanto da fare. Chi conosce a fondo le problematiche del territorio è fonte preziosa di suggerimenti. Ascoltare in modo attento le singole realtà potrà fare davvero la differenza. Sarà importante impegnarsi, inoltre, affinché le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possano finalmente trovare utilizzo tempestivo ed efficace. Solo in questo modo, infatti, la generica autorizzazione di spesa di somme ingenti a valere su questo fondo uscirà dalle secche dell'immobilismo e le risorse saranno immesse per davvero nell'economia. Fino ad allora questo Fondo sarà virtuale e non reale. Per il Sud possiamo - per esempio - da subito recuperare tanti progetti validi che sono stati accantonati e avere più coraggio e ambizione. Abbiamo anche chiesto a gran voce che nel Piano rientrasse il ponte sullo Stretto. *(Applausi)*. C'è stato detto che non era possibile inserirlo tra le opere realizzabili entro il 2026. Ne abbiamo preso atto, ma siamo convinti del contrario, anche perché il progetto è pronto da tempo e potrebbe partire immediatamente. Per questo temiamo che, in realtà, manchi la volontà di portarlo avanti. Lo consideriamo un errore perché abbiamo competenze, capacità e risorse per farlo. Pertanto, confidiamo che il progetto possa essere realizzato con il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il ponte sullo Stretto è un'opera strategica per l'Italia e per l'Europa, oltre al fatto che darebbe una risposta alla crisi di una Regione che rappresenta il Sud nel Sud. Presidente, mi riferisco alla Sicilia,

nel frattempo, serve agire subito per salvare tanti lavoratori onesti che, con il loro sacrificio, hanno contribuito a limitare la diffusione dei contagi. Il virus non si propagherà più velocemente se i ristoranti chiuderanno un'ora più tardi; non sarà quell'ora a cambiare le cose. La nostra economia va sostenuta da...

Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, Ministri, colleghe e colleghi, ho votato convintamente la fiducia a questo Governo e lei, signor Presidente, finora non ha tradito le aspettative, anche nella politica estera. Oggi si gioca una partita vitale attorno alla suddivisione delle risorse del PNRR. È verissimo che non si tratta di una questione di campanile, come ha detto lei: se si riprende il Sud, cresce tutto il Paese; è molto vero. Ma l'Europa ha stabilito alcuni criteri di riparto tra le varie Nazioni (PIL *pro capite*, popolazione e disoccupazione). Il Mezzogiorno, in base a quei criteri, ha fatto elevare notevolmente la quota dei fondi europei destinati all'Italia. Eppure, come lamentano le comunità che rappresentiamo, i criteri di ripartizione delle risorse adottati dall'Unione europea non corrispondono a quelli recepiti dall'Italia. In tal modo, il nostro Paese rischia di non colmare quel divario infrastrutturale e socio-economico che va avanti da troppo tempo. Anche nel Dopoguerra quasi tutti gli aiuti del Piano Marshall finirono nel triangolo industriale del Piemonte, della Lombardia e della Liguria, congelando ogni possibilità di sviluppo del Mezzogiorno, come evidenziato anche dall'illustre meridionalista Pasquale Saraceno. Ciò che è accaduto con il Piano Marshall rischia di accadere di nuovo oggi con il PNRR. Dopo decenni di interventi, il ritardo nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord, in termini di PIL *pro capite*, è oggi maggiore rispetto agli anni Le diseguaglianze e l'incidenza della povertà sono ampie, la dotazione infrastrutturale e la qualità dei servizi necessari pubblici sono insoddisfacenti. Basterebbe solo pensare alle ferrovie dello Stato e alla quantificazione economica dei costi netti del sistema per lo Stato e, per converso, alla condizione dei trasporti nazionali e locali del Sud. A Matera, città dalla quale provengo, capitale europea della cultura, i treni viaggiano ancora a scartamento ridotto; non c'è la ferrovia dello Stato, ma in compenso abbiamo la stazione. Le risorse del *recovery* *plan* sono dunque l'ultima occasione per il Mezzogiorno, per vedere rimossi quei blocchi che il Paese si porta dietro da oltre un secolo e mezzo. Non è un caso che una rete di sindaci - riuniti nella sigla *recovery* Sud - ritiene che il Piano non sia rispettoso delle indicazioni comunitarie. Sulla base di questi criteri, la cifra che dovrebbe spettare al Mezzogiorno non è del 40 per cento, ma si aggira tra il 66 e il 68 per cento. Che non si tratti di calcoli avventati lo rileva anche la dichiarazione che ha fatto il ministro Carfagna. La verità è che i vincoli territoriali suggeriti dalle commissioni, soprattutto sull'effetto di interdipendenza economica, non sono stati rispettati. È noto, infatti, che, per ogni 100 euro investiti al Sud, oltre 40 rimbalzano in termini di forniture nel resto del Paese: Paese: se dei 209 miliardi fossero destinati al Sud oltre 145 e 63 al Nord, attraverso l'effetto di interdipendenza economica, nel Mezzogiorno resterebbero 89 miliardi: il 42 sarebbe una percentuale...

finestra") *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente del Consiglio, desideravo da tempo poter interloquire con lei, e l'occasione odierna è quanto mai propizia. L'Italia sta decidendo importanti investimenti per il suo futuro, ma d'altra parte è legittimo porsi le seguenti domande: per chi stiamo facendo tutto questo? Chi beneficerà di queste opere e di queste riforme? Per chi ci stiamo indebitando? È notizia di questi giorni che, nel saldo tra nati e morti, abbiamo perso circa 400.000 abitanti: una città grande come Firenze. Come che sia, la tragica realtà dell'inverno demografico rischia di cancellare irreversibilmente il futuro del nostro Paese. A chi lasceremo tutto questo? A Paesi vicini, come ad esempio la Turchia, che vanta tassi di natalità più che doppi dei nostri? Parafrasando la famosa frase attribuita a Massimo D'Azeglio, dopo aver rifatto l'Italia, rischiamo di non avere più italiani a cui lasciarla. Signor Presidente, mi perdoni se dico un'apparente banalità, ma la vita umana, a cui tutti teniamo e che è necessario

Ecco che, per aggredire seriamente il declino demografico e con esso il declino economico e sociale dell'Italia, è quanto mai necessario tornare a investire sulla famiglia. "investire" e non "spendere", perché ogni euro investito nella famiglia rende infinitamente, sia sul piano economico che su quello della crescita umana e sociale del Paese. L'assegno unico è un primo passo, ma non basta.

È necessario mettere coraggiosamente mano a riforme strutturali che garantiscano un *humus* in cui gli oltre 20 milioni di famiglie italiane e i quasi 10 milioni di giovani possano prosperare. Le politiche familiari - come insegna il professor Pierpaolo Donati - devono essere soprattutto specifiche, distinte dalle pur utili politiche sociali e dalla lotta alla povertà, e mirate a promuovere il nucleo familiare e non i suoi singoli componenti. In questo senso, vanno bene le politiche di investimento, di cui alla missione 6 del PNRR, che testé ci ha illustrato, sia con riguardo alla maternità, sia con riguardo alla conciliazione dei tempi casa-lavoro, facendo attenzione tuttavia a non dimenticare che è necessario promuovere anche la paternità e garantire ai bambini una relazione equilibrata e corretta sia con la mamma, sia col papà.

perché così molte giovani coppie potranno coronare il loro sogno, radicandosi sul territorio e frenando la tentazione al nomadismo. C'è però un altro aspetto che sottoponiamo alla sua attenzione: l'equità fiscale. di privilegi, signor Presidente, ma di semplice equità, perché è assurdo e contrario all'articolo 53 della Costituzione pagare tasse su redditi e spese destinate all'adempimento del dovere, costituzionalmente imposto ai genitori, di mantenere, istruire ed educare la prole. È auspicabile che si metta mano ad un'ulteriore incentivazione per tutte quelle piccole e medie imprese familiari che, col lavoro di mamma, papà, nonni e figli, fanno grande ogni giorno il nostro Paese. Ci sono molte altre politiche familiari, signor Presidente, che vorremmo raccontarle e speriamo di poterlo fare presto, con un po' più di calma. Tuttavia, il problema della natalità non è solo una questione economica. Non è un mistero che la famiglia naturale, così come riconosciuta dalla Costituzione, sia sotto pesante attacco ideologico e sono poste all'esame leggi divisive e ideologiche, che vengono spinte ossessivamente in un momento in cui il Parlamento e il Paese avrebbero bisogno della massima unità e della massima coesione per superare questa emergenza. Modelli sociali para-familiari o, peggio, pseudo-familiari vengono proposti continuamente e in modo ossessivo alle giovani generazioni. Signor Presidente, tutto rischia di diventare famiglia e, conseguentemente, nulla più sarà famiglia. È chiaro che questo gigantesco esperimento di ingegneria sociale, molto caro ad alcune realtà italiane ed europee, è già in larga parte realizzato nei Paesi cosiddetti avanzati e i risultati sono là da vedere: l'individuo prende il posto della persona e la solitudine diventa la cifra demografica del tessuto sociale. In Svezia già oggi il 50 per cento degli abitanti vive da solo. Senza famiglia, le persone nascono, crescono, vivono e muoiono sole. Per questo, signor Presidente del Consiglio, per invertire il *trend* demografico, il *trend* sociale e, in definitiva, il *trend* culturale, è necessario restituire alle politiche familiari il posto che meritano nel bilancio pubblico, ma anche avere ben chiaro il paradigma culturale a cui vogliamo riferire la nostra azione. Non ci ha convinti, presidente Draghi. Non ci uniremo al coro che plaude all'evento epocale e storico di quest'Assemblea commissariata e dello scenario mediatico, colonizzato da corporazioni e oligarchie che limitano il dibattito e il pensiero discordante. Fuori dalla bolla non siamo soli. Domenica, in piazza del Plebiscito, a Napoli, c'era il movimento dei 500 sindaci a protestare contro l'iniqua distribuzione dei fondi e ieri, a piazza Montecitorio, c'era la Società della cura: oltre 1.400 reti nazionali, organizzazioni, movimenti e i partiti della sinistra che protestavano. Lei non rappresenta il nuovo, ma un sistema vecchio e superato dai fatti che non vuole cedere il passo. Lei rappresenta una restaurazione imposta, un modello del XVI secolo che non è adatto ad affrontare il futuro, che chiede invece giustizia sociale ed ecologica, fuori dalla crescita infinita in un mondo finito, fuori dalla competitività sfrenata e dal mito della privatizzazione dei servizi - le cui magnificenze lei celebra e rilancia ancora che hanno mostrato i nervi scoperti del fallimento sin dalla crisi del 2008, qui da noi col crollo del ponte Morandi, con i suoi morti, e in tutto il mondo con questa pandemia. Eppure, non cambia passo, ma accelera.

cultura, settore devastato dalla pandemia, con 1,1 miliardi, lo 0,6 per cento, per il patrimonio culturale e 0,16 miliardi, ossia niente, per l'industria culturale. Salta il salario minimo legale, che pure c'era. Un Piano scritto da McKinsey su mandato di Confindustria Nord, dunque. Per spianare la strada agli investimenti il Piano mette in campo le vecchie idee: liberare l'iniziativa economica dai controlli. Si limita ancora la responsabilità per danno erariale e si semplificano le verifiche antimafia fino al 2023, nonostante la bocciatura secca dell'Autorità nazionale

celebrato come una vittoria, mentre si tratta di una sottrazione di ben 60 miliardi. L'Europa ha usato precisi criteri per destinare i fondi per la disparità territoriale; ha valutato l'inverso del PIL, la disoccupazione e la popolazione, e all'Italia sono state assegnate fine di ridurre la disparità territoriale tra Nord e Sud dovuta alla cronica arretratezza economica e sociale delle otto Regioni meridionali. Non conta la sbandierata previsione di crescita attesa; il divario non verrà colmato dall'indice che al Sud si spera passi dal 22 al 24 per per una popolazione che rappresenta ben il 34... colleghi senatori, membri del Governo, signor Presidente del Consiglio, il Piano nazionale di ripresa e resilienza contiene sì numeri, scadenze e progetti, ma è una strategia del futuro, che cambierà l'Italia: è la direzione in cui si registrerà il cambiamento e non possiamo sbagliare. Quando parlo di cambiamento, intendo quello vero, ossia quello che vedrà al primo posto i deboli e i bisogni dei cittadini. Ma questo avverrà? avverrà? Dipende da noi. Avverrà quando le parole "sostenibilità", "transizione ecologica", "resilienza", "uguaglianza", "coesione territoriale", "colmare il divario fra il Nord e il Sud", non saranno degli *slogan*, ma saranno sentiti e accompagnati da azioni chiare. È una corsa contro il tempo - questo lo sappiamo - e riconosciamo il grande lavoro che è stato fatto; ricordiamo anche che è stato iniziato dal presidente Giuseppe Conte. Sì, è una corsa, ma il Parlamento vuole e deve esserci. Abbiamo lavorato sul Piano con una relazione che riportava molte osservazioni, ma devo dire con rammarico che molte proposte nel Piano non le abbiamo ritrovate, soprattutto quelle che riguardavano la tutela del nostro ecosistema, della biodiversità, della risorsa idrica. Voglio sperare che il Piano, che ha un carattere generale, in seguito abbia nei progetti delle linee chiare da poter seguire; progetti che - lo ripeto, anche come parlamentare - tuttora non abbiamo conosciuto. È un piano tecnico a cui dobbiamo aggiungere un pezzo di cuore. Anche lei, presidente Draghi, all'inizio del suo discorso ha detto che in quel piano ci sono volti e vite umane. Ma non basta l'aumento del prodotto interno lordo, non basta aumentare l'occupazione; creare benessere è un'altra cosa: un'altra cosa: significa che il tutto deve viaggiare insieme alla cura dell'ecosistema, alla diminuzione dell'inquinamento, alla salute dei cittadini. In quel piano, al primo posto deve esserci la tutela della vita del pianeta;

prevedrà una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 fino al 2040: quindi un piano di circa 10 miliardi.

come facciamo a dire che daremo veramente un futuro ai nostri figli? Concludo richiamando anche l'impegno del Governo a varare delle misure di semplificazione per il superbonus; in realtà, non servono solo misure di semplificazione: bisogna finanziarle, e l'orizzonte del 2023 deve essere chiaro per poter continuare un lavoro ben iniziato. La bellezza del nostro Paese va tutelata perché è unico al mondo, come Venezia che ha la sua fragile laguna, come gli ulivi secolari in Puglia, come le nostre splendide coste come i nostri corsi d'acqua e il patrimonio culturale. Ma poi c'è un'altra bellezza importante, che è il sorriso su ogni volto che ora è coperto da quelli che sono stati i nostri errori: il Covid-19 è infatti un errore che deriva da un modello economico sbagliato e questa transizione è necessaria per un modello che sia economico ed ecologico,

il Piano nazionale di ripresa e resilienza penalizza ancora una volta il Sud, destinandogli solo il 40 per cento delle risorse. È vero, verranno finanziate opere pubbliche importanti e ci saranno interventi che certamente porteranno beneficio e sviluppi al Mezzogiorno. Ma, nonostante i grandi passi avanti fatti dall'attuale Governo rispetto a quello precedente e l'apprezzabile lavoro del ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, il Mezzogiorno continua a essere la parte più debole del Paese. Il *recovery plan* rappresenta l'ultima vera occasione di riscatto per il Mezzogiorno, che non pretende di più, ma reclama solo ciò che gli spetta secondo i criteri di distribuzione dei fondi indicati dall'Europa. Da sindaco calabrese e da senatore della Repubblica, che porta in quest'Aula la voce degli amministratori e dei sindaci meridionali del *recovery Sud*, così come ho fatto in altre occasioni, proprio per tutelare fino in fondo i diritti di tutti i cittadini, non voterò il *recovery plan*, ma continuo ad avere fiducia, ritenendo che questa sia comunque una straordinaria opportunità data al Sud. Mi auguro che i fondi possano arrivare direttamente ai Comuni, perché i sindaci, soprattutto quelli del Sud, trovino il modo di non restituire i fondi, ma di spenderli per le loro comunità. Concludo ringraziando il Gruppo a cui appartengo per il contributo che ha dato, attraverso i suoi Ministri e i suoi Sottosegretari. Li ringrazio e in questo momento per me non esistono colori politici, se non il verde, il bianco e il rosso della bandiera italiana e della fascia tricolore che indossano tutti i giorni i sindaci. Quel tricolore che racchiude in sé ed esprime gli ideali, i valori e i principi dell'unità, simbolo indiscusso dell'Unità di Italia, che da Nord a Sud ha il dovere di garantire pari dignità umana, sociale ed economica a tutti i cittadini italiani. Signor Presidente, professor Draghi, il tema della giustizia è cruciale per la ripresa e lei ha fatto bene ad ampliare in modo significativo il relativo paragrafo nel suo Piano, rispetto alle due striminzite paginette della bozza iniziale.

Per questo le risorse dedicate alla giustizia dal *recovery fund* sono insufficienti, direi quasi irrisorie. Non c'è riforma delle regole processuali o sostanziali che possa funzionare senza risorse adeguate. Serve un forte investimento sul piano organizzativo e sul piano del personale amministrativo, ma soprattutto dell'organico dei magistrati. Solo per fare un esempio estremo, chi pensa di risolvere i problemi mediante la formula del ricorso in luogo dell'atto di citazione per introdurre il giudizio o è un illuso, o non è mai stato in un'aula di tribunale.

a far scrivere le sentenze da chi, pur membro dell'ufficio per il processo, non è un giudice. E ancora: no al giudice unico di appello; la collegialità è un valore e non possiamo dimenticarlo. per gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al processo (mediazione, negoziazione e arbitrato), ma no all'obbligatorietà; occorre salvaguardare il diritto di ogni cittadino ad un giudizio sui propri diritti.

lavorano con abnegazione e senso di sacrificio, senza alcuna tutela previdenziale e assistenziale e con un compenso a cottimo quasi ridicolo. Senza di loro la giustizia italiana collasserebbe. Bisogna riconoscere la loro grande professionalità, il loro senso dello Stato e vanno quindi stabilizzati sulla base della stessa legge che stabilizzò nel 1974 i vice pretori onorari. Sul processo penale, spesso il processo è la vera pena che colpisce indifferentemente colpevoli e innocenti.

C'è un grave problema di abuso della carcerazione preventiva, che lei e il suo Governo dovete finalmente avere il coraggio di affrontare. Pensi che solo la cosiddetta

che abolisce la prescrizione dopo la sentenza di primo grado persino per chi è stato assolto, va sospesa, professor Draghi, in attesa della riforma, invano promessa, dell'istituto, tanto annunciata ma mai attuata. No agli imputati a vita. E, ancora, sull'ergastolo ostativo (mi ascolti, professore, per cortesia), è inutile che lei vanti nella sua relazione una legislazione all'avanguardia nella lotta alla criminalità organizzata, se poi si rimettono in libertà persino i mafiosi che sciolgono i bambini nell'acido. Noi lanciamo una sfida: cambiamo la Costituzione, se è necessario, ma i criminali mafiosi devono rimanere in carcere, non devono essere messi in libertà. Mi avvio alla conclusione. Lei dice Lei dice che bisogna riformare il CSM; noi le diciamo: basta con la degenerazione correntizia e con il mercimonio delle più alte cariche della magistratura! Bisogna essere radicali, bisogna adottare il sistema del sorteggio temperato. E, ancora, no alle porte girevoli tra magistratura e politica: il magistrato che si candida, eletto o meno che sia, non deve tornare a svolgere funzioni giurisdizionali. occorre riformare la responsabilità civile dei magistrati. No a un privilegio medievale: in democrazia chi sbaglia paga. Faccia questo, professor Draghi, e avrà noi al suo fianco.

ho ascoltato con attenzione il suo discorso sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e la ringrazio, perché ha premesso all'illustrazione degli obiettivi, dei progetti e delle risorse una visione, che è il filo rosso che unisce tutto lo svolgimento del Piano. Al centro c'è l'Italia, il suo futuro; al centro ci sono le persone che l'Italia abitano e, come lei ha detto, la vita degli italiani, dei giovani, delle donne, degli anziani, di chi ha dovuto tenere chiusa la propria attività per tutelare la salute di tutti e i territori svantaggiati. Ci ha ricordato - e ne siamo tutti consapevoli i *gap* strutturali del nostro Paese, in particolare la necessità imprescindibile di riformare la giustizia e la pubblica amministrazione. Pensiamo a quanto gli uffici di progetto dello Stato siano stati essenziali per la ripartenza e la ricostruzione quindi fondamentale, per dare supporto al tutto, innestare in fretta risorse fresche e qualificate negli uffici pubblici. Ci ha ricordato le riforme. Colleghi, sulle riforme si parrà anche la nostra nobilitate, perché ci vuole lo sforzo di tutti, ma del Parlamento *in primis*, per fare le riforme necessarie, come ci ha ricordato in un intervento molto applaudito il senatore Zanda la scorsa settimana. Ruolo centrale del Parlamento, ma per farlo occorre - e qui la cito di nuovo - non avere «miopi visioni di parte anteposte al bene comune». Signor Presidente, lei ha sottolineato le direttrici trasversali che innervano il Piano: la clausola di condizionalità su giovani e donne, come lei sa fortemente richiesta dal Partito Democratico, affinché tutte tutte le misure abbiano delle ricadute su questo, e la scommessa sullo sviluppo del Sud per la crescita dell'Italia tutta. Non ci sono solo enumerazioni e statistiche nel suo discorso, ma il profilo di una comunità. è risultato chiaramente anche dagli esempi che ha fatto per parlare della trasformazione digitale, perché tutti i ragazzi e le ragazze possano scegliere le migliori opportunità formative, perché con la telemedicina non solo gli anziani, ma chiunque ne abbia bisogno possa essere meglio assistito. A questo deve poi arrivare la trasformazione digitale. È proprio dalle persone che lei è partito ed è su queste che anche io desidero concentrare alcune sottolineature. I dati che ci ha riportato sulla povertà assoluta sono allarmanti: la crescita dal 2015 al 2019 dal 3,3 al 7,7 per cento, addirittura quasi il 10 per cento nel 2020, ne abbiamo tutti contezza. Abbiamo tutti davanti agli occhi le file nelle nostre città davanti alle mense delle parrocchie o davanti alle associazioni di volontariato che danno il pacco alimentare. Gli effetti di questo impoverimento anche sul ceto medio non scompariranno a breve. Il soddisfacimento materiale è la prima risposta necessaria, ma non è sufficiente. La riduzione dei trasferimenti agli enti locali in passato aveva già indebolito le nostre reti sociali, la pandemia ha dato loro un colpo efferato. Per uscire da questa crisi, le infrastrutture sociali sono altrettanto importanti di quelle materiali (lei ne ha parlato). Occorre un sostegno progettato per non disperdere i punti nevralgici della cultura della solidarietà.

la ricostruzione della socialità, il rafforzamento del volontariato e del terzo settore renderanno più forte la nostra comunità. Un'altra sottolineatura riguarda il rafforzamento di tutto il percorso educativo. Agli asili nido sono destinati 4,6 miliardi, le stesse risorse che erano state pensate nel progetto del Governo precedente. Da alcuni anni per gli asili nido non si parla più giustamente di servizi sociali, ma di servizi educativi, perché questo sono. È una scelta importante che potrà essere implementata, non dimenticando che la carenza è soprattutto al Sud. Signor Presidente del Consiglio, abbiamo esperienze molto importanti, competenze formidabili maturate negli anni nei nostri Comuni.

comunali. Ho ancora negli occhi la straordinarietà di quei servizi, le insegnanti dei nidi e delle scuole dell'infanzia. Così, infatti, volevano essere chiamate, perché dicevano che la dicitura «scuole materne» si riferisce al fatto che i bambini sono delle mamme, invece quelle erano scuole dell'infanzia perché i bambini li fanno le mamme e i papà. Facevano esperienze straordinarie: ho visto laboratori con artisti importanti far lavorare i bambini degli asili nido, ho visto laboratori musicali dove suonavano tutti gli strumenti del mondo. A Reggio Emilia c'è stata una scuola, per quanto riguarda l'educazione all'infanzia, che ha fatto da esempio nel mondo. I genitori non desiderano solo che i loro figli siano accuditi; ci tengono alla qualità del loro tempo negli anni più importanti della vita. Pertanto, insieme alle costruzioni pensiamo a questo progetto. servizio civile è un progetto a cui io credo molto. Quando ho avuto la responsabilità del Ministero della difesa a volte venivo fermata e mi si domandava perché non ripristinavamo la leva obbligatoria; io spiegavo che è antistorica rispetto a quello che oggi devono fare le Forze armate, ma sarei stata molto d'accordo ad un servizio civile obbligatorio, per per i legami della nostra comunità e perché è un messaggio valoriale potente, fortissimo per i nostri giovani. Su questo ho presentato anche un disegno di legge. La proposta non è quella di un servizio civile obbligatorio, ma di implementare il servizio civile universale, che sarebbe già un segnale molto importante e sarà importante nella ripartenza.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

di quel protagonismo cui l'Europa l'aveva candidato. Vince l'Italia, se vince il Sud, si dice; ancora una volta non avverrà. Questo è il motivo per il quale ci sono state delle critiche prese di posizione da parte dei presidenti di Regioni del Sud e di ben 500 sindaci che si sono riuniti in piazza per evidenziare lo strappo che ancora una volta è stato compiuto a danno del Meridione. Nonostante le parole fatte giungere dal ministro Carfagna alla piazza, le perplessità restano tutte. La Ministra ha fatto riferimento alla Cassa per il Mezzogiorno, ai Fondi Voglio precisare che i fondi della vecchia Cassa per il Mezzogiorno ammontavano a 140 miliardi di euro e che i soldi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, oltre che i Fondi strutturali 2021-2027 e React-EU sono già dovuti al Sud, a prescindere. Non credo sia giusto presentare qualcosa che già è tuo di diritto come un regalo generosamente concesso. Sono sicura che la Ministra volesse evidenziare che finalmente, per una volta, i Fondi assegnati non saranno per buona parte dirottati al Centro Nord - spero - dopo più di venti anni di tale consolidata prassi, tanto regolare, quanto illegale. Voglio anche ricordare che la spesa per la Cassa corrispondeva a circa il 5 per cento del PIL, pari alla cifra annua garantita dall'Italia ai Paesi del Terzo mondo, quando al Nord, nel contempo, gli investimenti pubblici ammontavano al 35 per cento del PIL. Il vero punto della questione che ha indotto i 500 sindaci ad alzare la voce contro il piano è però che quanto si sta facendo passare per concessione straordinaria offerta al Mezzogiorno, assegnandogli il 40 per cento appena dei soldi di Next generation UE è in realtà un illegittimo dirottamento dei Fondi predisposti dall'Europa appositamente per il Sud Italia allo scopo di avvicinare le due parti del Paese. L'Italia è stata la la Nazione che ha beneficiato della fetta più cospicua dei fondi, il 28 per cento in più. Questo è avvenuto proprio a causa della difficile situazione del Mezzogiorno. Il Sud ha contribuito ad attivare ben 135 miliardi, dei 209 assegnati all'Italia dall'Unione europea. Pertanto al Sud sarebbe dovuto spettare il 65 per cento dei finanziamenti, ma così non è stato. L'Europa aveva dettato dei paletti molto precisi, che sono stati disattesi. C'è un aggravante se è vero che al Nord la pandemia ha mietuto tante più vite, al Sud ha portato tanta povertà. Pertanto, rifacendomi alla lettera scritta il 7 ottobre 2009, dove l'Europa intimava all'Italia il taglio laddove non avesse rispettato rispettato quei paletti che erano stati ben messi, ci sarebbero stati dei tagli. Mi chiedo cosa succeda ora e chiedo al presidente Draghi di porre qualche punto in più a favore del Sud.

ho cercato di sforzarmi di mettermi nei panni del cittadino comune, per capire cosa abbia recepito di questo Piano nazionale di ripresa resilienza. Ebbene, io penso che il cittadino italiano abbia capito che, innanzitutto, l'Europa c'è, l'Europa ha cambiato passo, l'Europa, finalmente, si sta dimostrando solidale ed è un processo che è stato avviato con il *quantitative easing*, di cui è stato autore proprio il presidente Draghi. Questo processo di solidarietà si sta perfezionando, purtroppo, in questa fase di pandemia, ma finalmente abbiamo l'Europa che tutti immaginiamo e sogniamo. Certamente, dobbiamo dire con molta chiarezza, signor Presidente, indietro non si torna. Non si può tornare indietro. Dobbiamo, però, dire, con altrettanta chiarezza, che tutto ciò dipende solo da noi, dalla nostra serietà e dalla nostra affidabilità. Se noi cederemo al richiamo dell'istinto naturale della ricerca del consenso, difficilmente attueremo questo piano ambizioso. Se, invece, avremo come bussola gli interessi generali del Paese, siamo convinti che si potrà portare a compimento questo Piano. L'altro elemento che rassicura il cittadino italiano è il fatto che i soldi ci sono, sotto varie forme: a fondo perduto, prestiti, fondi inimmaginabili. Tutto ciò lo rassicura, perché sa che non è più solo e, soprattutto, che può avere speranza: e senza speranza non può costruire il suo futuro. Poi, ci sono i dubbi e le preoccupazioni dei cittadini italiani, che io ho voluto sintetizzare con una domanda: ma siamo in grado di spendere tutti questi soldi? Soprattutto, siamo in grado di spenderli bene? La risposta, che purtroppo non c'è in questo Piano, si chiama riforme. Le riforme sono state rinviate. Pertanto, ci sarà la possibilità per il Parlamento di entrare nel merito di queste riforme. La vera sfida, però, saranno le riforme che attueranno il Piano nazionale. Lì si dimostrerà il coraggio di questa classe dirigente: se è una classe dirigente consapevole delle difficoltà del Paese oppure se è una classe dirigente tutta rinchiusa su se stessa. Il cittadino presidente Draghi, è consapevole della Babele normativa che lo attanaglia da troppi anni. Peraltro, a questa Babele si aggiunge la Babele narcisista di scienziati che, negli ultimi tempi, hanno messo da parte la scienza e hanno esaltato l'*influencer*. È un cittadino italiano, mi permetto di dirlo, sconfortato dalla Babele delle competenze, dei conflitti di competenze tra le Regioni e lo Stato centrale. Il nostro compito è abbattere tutte queste "Babeli". Siamo consapevoli che non ci sono più scuse, che dipende solo ed esclusivamente da noi, da questa classe dirigente. Presidente Draghi, il giorno dell'insediamento lei ha citato Schumpeter: sostituire parti vecchie con Le parti vecchie sono quelle obsolete, quelle che bloccano la libera iniziativa, quelle che non danno dignità alla persona. Noi auspichiamo, signor Presidente, che in questo Piano ci sia una vera e autentica transizione e non una associazione, perché transizione vuol dire mettere da parte le parti vecchie per costruire le parti nuove. Presidente, come lei ben sa, questo è un Governo frutto della generosità e della responsabilità di tutte le forze politiche diverse tra loro.

prima della partenza per Cleveland: sono convinto che, in uno dei momenti più angosciosi e nonostante tutti i soliti disfattisti che girano intorno a noi, l'Italia dimostrerà di essere pronta e degna fra i Paesi liberi e civili. Signor Presidente,

citando il nostro capo dipartimento, l'onorevole Bitonci, il Piano funziona solo se si affrontano le riforme, a partire dal taglio della burocrazia, per esempio.

finalmente sblocca 350 milioni di euro per il settore *tour operator*, agenzie di viaggi e fiere.

Alla proposta di qualcuno che vuole lanciare la moda di prendere il sole con la mascherina, rispondo provocatoriamente: facciamo *jogging* con la tuta da sci. A

inserire nel *recovery*, si rischia il blocco del settore. Sulla semplificazione ci giochiamo l'efficacia di questa misura. Non ci piove. La messa a terra di questa misura passa attraverso la semplificazione e ovviamente nel 2023 rischiamo il blocco degli investimenti da questo punto di vista.

Concludo perché il tempo non è molto. Il *recovery plan* evidentemente non può essere la soluzione a tutti i problemi, soprattutto se non è accompagnato dalle riforme che tutti si aspettano.

l'Europa e soprattutto lei, signor Presidente, difendeteci da quei Paesi che fanno concorrenza al nostro Continente, che queste regole non le rispettano. Fatelo e noi saremo con lei, *whatever it takes*, signor Presidente.

Signor Presidente del Consiglio, Signori Ministri, cari colleghi, il mio intervento, in considerazione del poco tempo disponibile, sarà rivolto a fornire alcuni suggerimenti tecnici e costruttivi, derivanti dall'esperienza governativa in tema di investimenti e dalla personale esperienza accademica in materia economica.

irripetibile per promuovere investimenti pubblici, introdurre riforme, sostenere lo sviluppo e realizzare la coesione sociale del Paese. Grazie al Governo Conte Il nostro Paese ha ricevuto più fondi europei per le condizioni di arretratezza socioeconomica in cui versa il Sud Italia, divenuta una delle aree più povere e sottosviluppate d'Europa.

in sede di assegnazione delle risorse ai singoli Stati membri. Altro che il 40 per cento dichiarato nel Piano: l'applicazione dei tre parametri (PIL medio *pro capite*, numero di abitanti e tasso di disoccupazione) avrebbero potuto garantire al Sud Italia il 65 per cento delle risorse stanziate. L'applicazione di questi stessi criteri alle singole Regioni del Mezzogiorno, Presidente, avrebbe prodotto un risultato di questo tipo: Abruzzo 4,2 miliardi, Molise 1,4, Campania 43, Puglia Puglia 26,7, Basilicata 2,2, Calabria 16,8, Sicilia 41,1, Sardegna 8,9. Presidente, per l'ennesima volta il Sud è sacrificato per l'interesse più generale del Paese. Questo lo possiamo solo considerare un buon punto di partenza. Per raggiungere gli obiettivi ambiziosi del Piano sono state confermate una serie di riforme: pubblica amministrazione, fisco, giustizia, semplificazione e concorrenza. Presidente, ritengo necessario che si adottino anche altre riforme, come quella del conflitto di interessi, dell'abuso d'ufficio, la riforma sul sistema bancario (soprattutto del credito cooperativo), il contrasto alla corruzione, all'infiltrazione mafiosa, alla speculazione finanziaria distruttiva dell'economia reale, quest'ultima riforma da sostenere, possibilmente, a livello europeo e internazionale. Inoltre, sono state già citate le riforme sui e aggiungo anche la riforma strutturale del debito pubblico, che definisca le modalità di rientro del debito e promuova un piano di autofinanziamento interno, Presidente, volto a favorire politiche di bilancio espansive senza ricorrere necessariamente ai mercati finanziari, ampliando il principio di trasferibilità dei crediti fiscali anche ai crediti verso la pubblica amministrazione e prevedendo un istituto speciale di investimento che dovrà canalizzare in maniera fruttifera

da oltre 100 miliardi di euro è di oltre quindici anni, contro i dieci anni di Germania e Francia.

La nuova riforma in materia di appalti pubblici dovrà dare certezza al quadro normativo, ridurre le diverse fasi degli investimenti, introdurre nuovi strumenti gestionali di monitoraggio, risolvere l'annoso problema dei ricorsi e dei contenziosi, prevedere un certificato di qualità delle imprese affidatarie, che attesti la loro sostenibilità economico-finanziaria, onde scongiurare crisi aziendali in corso d'opera, rivedere i compiti del e, inoltre, introdurre una *accountability* verso i cittadini sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Inoltre diventerebbe anche importante, per il Sud Italia, l'inserimento della cosiddetta clausola di inclusione economica.

certe di reintegro dell'anticipazione di 15,5 miliardi di euro per i fondi FSC, sulla realizzazione di centri di ricerca e stazioni di rifornimento di idrogeno anche nel Sud Italia, sul rafforzamento della spesa per l'ammodernamento delle linee ferroviarie interne al Meridione, con particolare riferimento alle infrastrutture di prossimità (in Aula sono state già citate le tratte Taranto-Bari chilometri) e sulla possibilità, anche per il Sud, di intercettare i traffici marittimi intercontinentali. Nella realizzazione della transizione energetica saranno poi importanti le decisioni sull'impianto siderurgico di Taranto, dove l'unica transizione ammissibile dovrà prevedere l'abbandono del carbone, non più sostenibile, sperimentando nuovi processi produttivi innovativi, ambientale speciale (VIAS) e anche un accordo di programma, finalizzato a gestire le linee produttive destinate alla chiusura. Signor Presidente, concludo ricordando che il successo del piano di ripresa può dipendere solo dalla crescita del Sud Italia. La pandemia ci lascia un Paese con maggiori disuguaglianze, che non possiamo ignorare. L'Europa ha condizionato l'erogazione dei fondi alla riduzione dei fondi alla riduzione di tali disuguaglianze: non possiamo rischiare di perdere tali risorse. I fondi destinati al Sud sono ritenuti insufficienti e continueremo a sostenere la necessità di rivedere tali risorse per il Sud. Allo stesso tempo, sappiamo che oggi la partita più importante da vincere è quella di spendere queste risorse nel miglior modo possibile. *(Applausi)*.

Oggi, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, non c'è solo una luce che intravediamo, ma una serie di lucine accese, che tutte insieme possono illuminare il destino del nostro Paese. lucine accese anche dal lavoro di interlocuzione che il Parlamento ha compiuto, che dovrà continuare e che lei, signor presidente Draghi, opportunamente richiama. Sono lucine accese, che devono rimanere tali, anzi essere sempre più luminose, grazie all'attuazione concreta del PNRR. La crisi è sanitaria e da lì bisogna ripartire, per illuminare il nostro cammino, La crisi è sanitaria e da lì bisogna ripartire, per illuminare il nostro cammino, per rispetto dei nostri 120.000 morti: non dimentichiamo mai che siamo in debito con le loro famiglie e con il personale socio-sanitario, che ha lavorato e che in molti casi ancora lavora in condizioni pazzesche. Le riforme che dobbiamo affrontare devono partire dai nodi strutturali non risolti del nostro sistema Paese, che forse è l'ultima occasione per sciogliere, ha ragione, presidente Draghi. Mai più ospedali intasati, malati non Covid abbandonati, ritardi nelle cure domiciliari. Mai più differenze tra Regioni persino nella scelta delle priorità tra le persone da vaccinare che abbiamo toccato il culmine - che, grazie al suo Governo, è stata definita e ordinata, vaccinando per primi gli anziani e i fragili, con il suo personale monito morale, oltre che con l'impegno del generale Figliuolo, a non scavalcare le priorità. Mai più far saltare il tracciamento del virus, non investire in ricerca, in intelligenza artificiale, in telemedicina e in cure personalizzate. Mai più le RSA come le abbiamo conosciute, pratiche burocratiche infinite e i nostri giovani medici specializzandi scoraggiati. Una sanità dunque rinnovata tecnologicamente e, nello stesso tempo, umana rappresenta il migliore fattore di protezione per l'economia e per i riflessi sull'occupazione. La sanità, con la giustizia e il lavoro, costituisce uno dei pilastri fondamentali dello Stato sociale. i 20 miliardi del PNRR da spendere per prevenzione, medicina territoriale, sanità digitale e assistenza domiciliare. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo spirito repubblicano che il Presidente del Consiglio giustamente evoca e che suscita in me commossa emozione deve annullare tutte le classi dirigenti, ma soprattutto la politica e la scienza, in un rilancio etico per il personale, per tutte le professioni, per i quadri amministrativi del nostro Paese. discorso, presidente Draghi, un destino diverso e luminoso del PNRR perché è teso a coinvolgere tutta la Nazione, per essere un tutt'uno con la cittadinanza. Una cittadinanza che tanto ha sofferto, anche prima dell'epidemia, per una sanità che non sempre è arrivata con efficacia alle porte delle persone, specialmente nei paesini più sperduti del nostro Paese. Cittadine e cittadini informati e coesi in una comunità nazionale lungimirante. Una cittadinanza che in questi quattordici mesi, per grandi numeri, ha dimostrato coraggio e sopportazione e di cui dobbiamo essere orgogliosi e del cui benessere e della cui dignità Quindi il PNRR non deve e non può essere un insieme slegato di progetti, cosa che lei ha giustamente sottolineato, ma deve avere una visione coraggiosa e fattiva, che non può più tollerare rendite di posizione: una volontà vera, dunque, per l'innovazione e la modernizzazione attraverso due percorsi, a mio avviso. Innanzitutto, la realizzazione pratica di una medicina territoriale, inserita però in un progetto e in un modello di riforma nazionale, supportata da semplificazioni burocratiche e digitalizzazione, operazioni strettamente connesse tra di loro. Dobbiamo lanciare un grande piano di formazione dei professionisti socio-sanitari e del personale della pubblica amministrazione, con una strettissima sinergia socio-sanitaria. Senza il valore umano - lo abbiamo scoperto anche durante l'epidemia - non c'è riforma che tenga. Si rilanci il senso del lavoro in *équipe*, nella condivisione di progetti ambiziosi e concreti, per un *continuum* assistenziale senza buchi tra casa e ospedale e viceversa, con strutture intermedie realmente efficienti, concependo il medico di base come un primario territoriale insieme a gruppi multiprofessionali, in modo che nessuno possa sentirsi abbandonato in caso di bisogno. luogo, gli incentivi alla ricerca sui vaccini, anticorpi monoclonali e tutta la filiera industriale della sanità siano organizzati subito, alla stessa stregua della difesa di un Paese. Bene la creazione di un centro di eccellenza per la sorveglianza continua e la prevenzione di altre epidemie. A questo proposito, raccolgo il richiamo di eccellenze del settore scientifico sul fenomeno montante della resistenza ai batteri e, quindi, dell'impegno su questo per prepararsi ad altre problematiche. Concludo con la sensazione che il PNRR è uno sguardo già vivo e concreto, ma va confrontato da subito con l'attualità. La sanità come un grande investimento per la sicurezza e la cura della cittadinanza senza discriminazioni. È molto probabile che il PNRR andrà sostenuto e protetto e avrà bisogno di ulteriori risorse. Italia Viva ha lanciato per questo un piano sanità 2030, con un grande itinerario di ascolto di operatori e territori. Usciamo da un momento drammatico. Lei, signor Presidente del Consiglio, ha citato da De Gasperi, e a me piace ricordare l'onorevole Tina Anselmi, la madre del Servizio sanitario nazionale, che ricordava come negli anni Quaranta ci fosse la convinzione che il dialogo permette a un Paese di progredire. Anche se la frase che mi è rimasta nel cuore è: le conquiste non sono mai per sempre. Interpretiamo questa fase storica, colleghe e colleghi, con immenso spirito di servizio e predisposizione a un dialogo continuo: condizioni che, esse sole, possono determinare il destino dell'Italia a partire dall'attuazione pratica del Piano nazionale. Esistono protagonisti che sono riusciti a passare alla storia perché ci hanno lasciato in eredità straordinarie conquiste. Siamo di fronte a un vero Dopoguerra e spetta a noi tutti, dal Palazzo alle piazze, riuscire a concentrare così grandi significati in fattive realizzazioni. Saremo giudicati e ricordati; meglio se avremo trasformato quello che appare come un sogno - del resto Shakespeare diceva che siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni - facendo dell'Italia, rispetto all'Europa, un modello di ricostruzione. Non un Paese indebitato, ma esempio di idee, progetti e innovazione.

Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, a me onestamente sorge qualche dubbio su questo PNRR. Soprattutto mi sorge il dubbio che sia stata una trattativa tra lei e la Commissione europea: infatti, quando sento dire «garantisco io», mi viene il dubbio che forse l'Europa non si fida dell'Italia o non si fida degli italiani. italiani. A noi sembra impossibile che si possa esautorare questo Parlamento, che è l'unico luogo dove siedono i rappresentanti del popolo, e ci si nasconda dietro la data del 30 aprile. Sappiamo tutti che quella del 30 aprile non è una data perentoria e che qualche giorno in più si sarebbe potuto prendere se si avesse avuto a cuore il luogo deputato dove siedono i rappresentanti del popolo.

molto, molto forte. C'è un altro motivo per il quale, secondo noi, lei, presidente Draghi, avrebbe dovuto avere più rispetto per il Parlamento. Parlamento. Quando doveva formarsi il suo Governo, Fratelli d'Italia chiedeva le elezioni, perché diceva: «Diamo, come è scritto nella nostra Costituzione, la parola al popolo italiano, che sicuramente anche in una fase così difficile saprà scegliere per il meglio». Ma ci veniva risposto di no: siamo una Repubblica parlamentare, quindi se il Presidente quindi se il Presidente del Consiglio incaricato trova la maggioranza in Parlamento, si rispetta la Costituzione. Ebbene, presidente Draghi, lei è proprio il frutto: è seduto su quella sedia proprio perché c'è stata un'interpretazione sulla Repubblica parlamentare. Invece vediamo che per lei il Parlamento è qualcosa di fastidioso. Capiamo, è un rito che deve fare; oggi è venuto qui e ci ha letto la sua interpretazione, la sua visione di quella che deve essere l'Italia del futuro, ma ha rifiutato di dare il tempo a tutti noi di poter approfondire. Noi abbiamo un ruolo anche più difficile, se mi consente, perché noi rappresentiamo l'opposizione in questo Parlamento, ed essere opposizione è un compito molto difficile che ci fa assumere ancora più responsabilità. Come potremmo dare il nostro voto come se firmassimo una cambiale in bianco? La realtà La realtà è che non possiamo in ventiquattro ore; per carità, qui siederanno tutte persone più perspicaci e più veloci di noi, che hanno saputo leggere molto bene e dettagliatamente tutte le pagine del suo PNRR. Per noi non è così. Però dobbiamo anche sfatare un altro mito, anche perché non bisogna dare tutte queste speranze agli italiani, dicendo che adesso arriveranno i soldi dell'Europa e del *recovery fund* e si metteranno a posto tutti gli enormi danni che ha provocato la pandemia alla nostra Nazione.

200 miliardi. Oggi noi stiamo parlando di 130 miliardi di debito, ma quei 200 miliardi sono stati spesi non male, malissimo, perché certamente non sono serviti a tenere in piedi l'economia, non sono serviti a salvaguardare i posti di lavoro e non sono serviti ad aiutare gli ultimi. Sono stati buttati nel cestino, perché voi avete speso quei 200 miliardi con una visione ideologica, che è quella di accontentare un po' tutti i partiti della maggioranza. E ci siamo trovati il *bonus* vacanze, che certo non mi sembra uno strumento per aiutare il turismo; ci siamo trovati i banchi a rotelle, che sono stati devastanti, devastanti, perché vediamo come è messa la scuola ancora oggi, e non ci sembra certo che abbia aperto in sicurezza. Avete dato delle mance; noi li abbiamo chiamati non decreti sostegno e ristoro, ma elemosina. Lei si ricorderà bene che

ci vuole un bel coraggio a chiamarlo decreto sostegni. Pertanto, il mito che si deve sfatare è proprio quello di non presentarsi agli italiani dicendo che adesso arrivano i soldi dell'Europa. Peraltro, molti di questi sono un debito che peserà sulle nostre future generazioni.

quando ci capita di leggere articoli sui giornali, molto spesso il titolo cattura la nostra attenzione. Poi, ahimè, quando andiamo a leggere il contenuto dell'articolo, vediamo che è molto distante dal titolo del giornale. Qui è un po' la stessa cosa: cosa: chi non è d'accordo sulla riforma fiscale? Tutti siamo d'accordo che è necessaria una riforma fiscale; tutti siamo d'accordo che in questo Paese le tasse sono troppo alte, ma lei per questa riforma fiscale, Presidente,

europea) - che bisognerà rivedere e rivalutare i valori catastali. Per noi questa si chiama patrimoniale mascherata con un vestito nuovo e diverso, ma sempre di aumentare le tasse si tratta.

su coloro che sono proprietari di immobili. E non parliamo di quelli ricchi, Presidente, ma parliamo della maggioranza degli italiani che, dopo una vita di sacrifici e di sudore della fronte, è riuscito a comprarsi una casa. Quindi, capisce che il titolo può essere fuorviante. Ma abbiamo un'altra preoccupazione. Abbiamo visto come la sua maggioranza si sia divisa su un'ora in più di coprifuoco, mentre lei sa che noi riteniamo che non fosse proprio nelle sue facoltà mettere il coprifuoco, perché crediamo che compito di un Governo sia quello di studiare i protocolli,

Capisco che per tutti lei è "super Mario", ma come farà a realizzare le riforme con una maggioranza che giustamente e lecitamente è contrapposta sulla visione dell'Italia e della Nazione? E allora quale sarà la sua riforma della giustizia? Quella del MoVimento 5 Stelle, che vuole tutti in galera, o quella di una parte dei partiti che sostengono la sua maggioranza, come chiediamo noi, che anche il processo si velocizzi, visto che oggi non c'è mai fine al processo? Starà con chi vuole togliere il carcere ostativo o starà con quella parte della maggioranza che vuole la certezza della pena? Sul fisco le ho già detto. Ciò che ci preoccupa è che anche lei, in questo documento, ci dice che prima bisogna fare le riforme e poi gli investimenti. Presidente, capisco che non è avvezzo alla politica, ma alla storia dovrebbe esserlo. Basterebbe che lei studiasse ciò che è successo negli ultimi anni, quando molti soldi non si sono spesi perché andavano a infrangersi contro il muro della burocrazia.

Presidente, dopo più di quattordici mesi di incubo, credo che oggi sia una buona giornata, una giornata di speranza per tutti gli italiani. Next generation EU ci fa compiere un passo verso una Unione della solidarietà e della responsabilità; un'Unione che è più forte della somma delle parti, ha detto il Presidente della Commissione europea il 28 novembre scorso, inaugurando l'anno accademico dell'università Bocconi. Solidarietà e responsabilità sono le due parole chiave attorno a cui ruota tutto questo progetto. La pandemia ha portato a un salto in avanti dell'Unione europea, inimmaginabile fino a poco tempo fa. Il Next generation EU non è solo uno strumento di portata senza precedenti; è finanziato con titoli di debito comune, verrà ripagato in parte con imposte comunitarie e viene ripartito secondo criteri di solidarietà. non era scontato che l'Italia diventasse il primo beneficiario di questo programma. *(Applausi)*. Aver ottenuto questo risultato è una grande vittoria di chi, a Roma come a Bruxelles, ha sempre lavorato per l'Europa della solidarietà e della responsabilità. una battuta d'arresto, anzi una sconfitta, di chi in Europa ha remato contro e in Italia sosteneva, anche in quest'Aula, che dall'Europa era meglio uscire; e oggi finalmente ha cambiato idea. Presidente, il Piano che oggi votiamo non è solo un atto di solidarietà; ci carica di responsabilità, perché quanto accadrà in Italia da oggi al 2026, ossia se noi saremo o meno in grado di utilizzare al meglio questa opportunità, sarà un elemento decisivo. Sarà decisivo per consolidare questa svolta politica. Sara decisivo per archiviare definitivamente la stagione dell'austerità. Sarà decisivo per rendere permanente il Next generation EU. Non dimentichiamo che con questo programma noi prendiamo in prestito denaro dalle generazioni future. È innanzitutto per questo motivo che dobbiamo mettere a terra questi soldi nel migliore dei modi. I progetti del Piano che oggi discutiamo possono cambiare il volto dell'Italia nei prossimi anni, perché i soldi per la digitalizzazione possono portare Internet ultraveloce dappertutto e questo cambierà il modo in cui funzioneranno i servizi pubblici, il modo in cui si studierà e si lavorerà. I soldi per la transizione ecologica aumenteranno la produzione di energia pulita, ci aiuteranno a migliorare la rete idrica, la gestione dei rifiuti, il trasporto pubblico locale. Il superbonus, su cui questo Piano stanzia 14 miliardi di euro, aiuterà decine di migliaia di famiglie a risparmiare energia e farà ripartire l'edilizia. È positivo che il presidente Draghi si sia impegnato a prorogarlo al 2023. I soldi per le infrastrutture porteranno finalmente l'Alta velocità anche nel Mezzogiorno e ci permetteranno di mettere in sicurezza ponti e viadotti.

Finanzieremo progetti di formazione e di riqualificazione, aiuteremo l'imprenditoria femminile e cambieremo il sistema sanitario nazionale, perché quei quasi 19 miliardi del Piano ci aiuteranno a rafforzare la presenza sul territorio e a investire massicciamente in tecnologia e in digitalizzazione. Signor Presidente del Consiglio, dietro tutti questi progetti è visibile quella nuova visione dell'economia di cui ha parlato oggi Giuliano Amato. È una visione in cui ci riconosciamo pienamente: un'economia sostenibile sul versante sociale e ambientale, in cui il capitalismo è nuovamente temperato da principi etici; un'economia in cui pubblico e privato tornano a integrarsi. Le riforme, come ha detto anche oggi, signor Presidente del Consiglio, sono una componente decisiva del Piano non solo per attuarlo, ma soprattutto per superare le debolezze strutturali che spiegano vent'anni di stagnazione del nostro Paese. Il programma di riforme e il cronoprogramma contenuti nel Piano sono sfidanti, sono molto ambiziosi (pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione, concorrenza, Fisco) credo che ne siamo tutti consapevoli. Su queste tematiche i punti di partenza tra le forze che sostengono il Governo sono lontani e in qualche caso in passato sono stati anche contrapposti. Non è però una missione impossibile realizzare quelle riforme; le faremo se avremo la capacità politica di superare veti e di costruire punti d'incontro tra forze e interessi molto diversi *(Applausi)*. Questa, infatti, è la forza del riformismo quando diventa azione politica. Faremo queste riforme se dimostreremo con i fatti che le dobbiamo fare non perché ce lo chiede l'Europa, ma perché quelle riforme convengono all'Italia e agli italiani. tuttavia tenere a mente una lezione, perché più volte in Italia abbiamo cercato di fare le riforme strutturali per modernizzare il nostro Paese. I cambiamenti non sono mai un pranzo di gala, devono essere accompagnati da misure sociali per aiutare chi perde dalle riforme. Il riformismo calato dall'alto sulla testa del popolo è sempre destinato alla sconfitta Per questo, signor presidente Draghi, serve un nuovo patto sociale, un patto per la ricostruzione tra le forze politiche, il Governo, le parti sociali. È per questo che serve un'assunzione di responsabilità politica che vincoli tutte queste forze di fronte al Paese. Il lavoro deve essere al centro di questo patto per la ricostruzione, perché l'Italia impiegherà almeno due anni per recuperare quello che abbiamo perso nel 2020, quando quasi un milione di persone hanno già perso il lavoro; precari, autonomi, giovani, donne e altri lo perderanno nei prossimi mesi. In quest'anno di pandemia le disuguaglianze sono aumentate e si sono aperte nuove fratture sociali ed è a rischio la tenuta e la coesione del Paese. Per questo nel Piano è necessario dare priorità ai progetti che creano più lavoro, a partire da quello per i giovani e per le donne, attuando concretamente la condizionalità che il Partito Democratico ha fortemente chiesto e ottenuto di inserire nel Piano. Next generation EU deve servire per migliorare i servizi per l'impiego, per rafforzare le politiche attive del lavoro, per aiutare le imprese che sceglieranno di non licenziare, per incentivare chi nei prossimi anni creerà lavoro e avvierà nuove imprese ed è cruciale mettere in campo nuove politiche industriali.

dobbiamo definire i percorsi più efficaci per coinvolgere nella fase di attuazione il Parlamento, gli enti territoriali, le parti sociali. È questo il senso della proposta di una Commissione bicamerale sul PNRR, è questo il senso della richiesta di creare i canali, affinché affinché tutto il Paese partecipi all'attuazione del piano *(Applausi)*. Signor Presidente del Consiglio,la via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà. Sono le parole di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi che concludevano il Manifesto...

anzi, meglio, con alcune incertezze che ci sono sui numeri delle risorse a disposizione. A pagina 22 del Piano c'è una tabella che riassume tutte le risorse: 191,50 miliardi del PNRR, 13 miliardi del React-EU e 30,64 miliardi del Fondo complementare, quello che viaggia nell'arco degli anni. Il totale fa 235,14.

da destinare alla realizzazione di opere specifiche. Il totale di queste risorse fa 276 miliardi. Capisco che sul PNRR dobbiamo scrivere le cose che riguardano direttamente il PNRR, però probabilmente se il Ministero dell'economia che verifichi le cifre e faccia capire tutte le risorse che sono a disposizione potrebbe sicuramente aiutarci. Il compito che attende tutte le forze politiche è quello della straordinaria opportunità economica e culturale di ridisegnare il volto dell'economia italiana, avviando una stagione di riforme strutturali e di politiche industriali, capaci quindi di costruire un ecosistema sostenibile, digitale e competitivo a livello europeo, ripensando anche il modello stesso di organizzazione territoriale attraverso la riqualificazione e la diffusione di servizi e infrastrutture, senza ovviamente dimenticare la specificità italiana. Voglio però andare nel concreto con alcuni accenni specifici. Parto dalla digitalizzazione; ritengo che sia necessario superare la logica di aree bianche e aree grigie per adottare quella del diritto universale alla connessione - ribadisco il concetto: diritto universale alla connessione coinvolgendo negli investimenti gli operatori che più guadagnano dalla diffusione capillare della Rete, dai fornitori di contenuti ai circuiti dei pagamenti digitali, ad esempio. Tra parentesi a pagina 100 del Piano, a piè pagina vi è una definizione delle aree e si fa dove c'è un minimo di confusione. Vengono citate le aree nere, che sono quelle dove noi sappiamo esistere più operatori, e sono definite a fallimento di mercato. Forse vale la pena di rileggere quella pagina perché mi sembra leggermente pasticciata. La digitalizzazione ovviamente è un passaggio fondamentale che segue logicamente il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Valorizzazione e inclusione del territorio nazionale non vuol dire solo promuovere itinerari turistici per borghi caratteristici, ma rendere quei borghi nuovamente abitabili, portando servizi, pubblica amministrazione, credito, sanità e infrastrutture materiali e immateriali, *hub* logistici, 5G, riqualificazione digitale degli uffici pubblici, stazioni di *coworking*, intercettando anche quel fenomeno che sta emergendo e che è stato definito deurbanizzazione. Inoltre la specificità tutta italiana del tessuto delle piccole medie imprese e della loro organizzazione in distretti industriali va valorizzata, creando le condizioni logistiche per la loro formazione anche nelle aree del Paese più periferiche. È un tema che riguarda il Sud, le isole, ma soprattutto e anche le aree interne. Dobbiamo investire in economia di prossimità, rendere tutto il territorio nazionale un luogo dove poter costruire il proprio futuro. Un secondo argomento che vorrei toccare velocemente è la *green* *economy*. La stessa logica di sviluppo deve essere alla base della tradizione energetica ed ecologica; bene quindi l'investimento sulla filiera dell'idrogeno e dell'economia circolare, ma attenzione al tema della mobilità elettrica, in particolare per quanto riguarda la realizzazione e lo smaltimento delle batterie al litio. C'è qui un auspicio alla realizzazione di impianti di costruzione di batterie, ma lei sa, Presidente, che in una ridente località svedese, ma anche a Torino, nelle aree ex Olivetti sono in costruzione impianti enormi; a Torino vengono investiti circa 4 miliardi,

Al di là però di questi progetti specifici, il tema non è tanto la produzione delle batterie, quanto l'approvvigionamento delle materie prime rare; litio, *in primis.* In questo senso sarebbe necessario un impulso maggiore per implementare la ricerca...

*(FIBP-UDC)*. Signor Presidente del Consiglio, il *recovery plan* rappresenta un'occasione importante, direi irripetibile per il rilancio del nostro Paese. La pandemia si è abbattuta con durezza sull'Italia colpendo soprattutto le componenti più fragili della società: donne e bambini. Il progetto di rilancio che con il PNRR stiamo delineando non poteva quindi - questo l'ho ripetuto in varie occasioni - prescindere da una particolare attenzione ai più fragili. Dobbiamo ripartire dalle famiglie e dai più piccoli, certamente il *recovery* prevede stanziamenti e risorse mai viste prima in favore di queste categorie, anche se confesso che avrei preferito un impianto un po' più organico. Mi spiego meglio: sarebbe stato bello vedere nero su bianco, fra le missioni del Piano, anche una specifica missione dedicata all'infanzia. Bambini e adolescenti sono il nostro futuro e ogni progetto per la ripresa e la rinascita dell'Italia deve necessariamente prevedere interventi in loro favore e in favore delle famiglie e delle coppie giovani. Ho apprezzato, signor Presidente, la chiarezza con la quale ha rappresentato la gravità della situazione demografica del nostro Paese: tanti morti a causa dell'epidemia, ma anche drammaticamente un crollo delle nascite. La peste bianca della denatalità ha trovato nella pandemia ulteriore linfa. È necessario rilanciare le nascite, molte coppie non fanno più figli, come lei ha ricordato, perché non riescono ad avere accesso ai mutui e quindi a comprare casa e a programmare il futuro. Come Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, ma prima ancora come donna e come mamma, ho più volte ribadito l'esigenza di un piano di investimenti per la fascia 0-6 anni. L'obiettivo che l'Italia deve porsi è che le spese per l'infanzia in generale e quelle per la famiglia siano almeno pari alla media europea. Un impegno straordinario - è innegabile - serve soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno, dove questa percentuale di offerta dei posti negli asili nido oggi appare un miraggio. È inaccettabile che ci siano bambini di serie A e di serie B solo perché nati in Regioni d'Italia diverse. Non dimentichiamo, poi, che la carenza di servizi educativi per l'infanzia, unita all'iniqua ripartizione dei carichi di lavoro familiare, condiziona negativamente l'offerta di lavoro femminile e riduce il tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro. In questa spirale, le donne madri si fanno carico di maggiori oneri e di maggiori responsabilità. Non posso, quindi, che apprezzare la scelta di proseguire nel solco tracciato, da un lato con l'istituzione dell'assegno universale per i figli e dall'altro con il finanziamento di 4,6 miliardi di euro per asili nido e scuole per l'infanzia e relativi servizi di educazione e cura. Secondo le stime, attraverso il progetto dovremmo giungere alla creazione di circa 228.000 posti. Certo, 900 milioni di euro per investimenti volti ad assicurare l'estensione del tempo pieno e delle mense sono un po' pochi, ma comunque lo voglio vedere come un punto di partenza soprattutto per il Mezzogiorno, dove, come sappiamo, non solo i nidi, ma anche il tempo pieno scarseggiano. Questa è una misura fondamentale per garantire ai genitori e in particolare alle donne la possibilità di conciliare la vita familiare e quella lavorativa. A tal proposito, giudico positivamente anche la proposta del ministro dell'istruzione Bianchi, che ha annunciato lo stanziamento di 510 milioni per tenere aperte le scuole per far recuperare la socialità ai ragazzi anche nei mesi di giugno e di luglio. Positivo è anche lo stanziamento di 3,9 miliardi per l'edilizia scolastica, risorse che devono tradursi non soltanto in importanti interventi strutturali e antisismici, ma anche in un più generale ammodernamento e in un'innovazione degli ambienti anche per superare le "classi pollaio". Le conseguenze dell'epidemia hanno messo a dura prova la salute psichica dei più giovani. So bene che il Piano ha privilegiato investimenti più concreti, ma a volte bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo e pensare anche ai beni immateriali come appunto il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti. Va valutata, quindi, prossimamente l'opportunità di prevedere nella missione istruzione e ricerca l'inserimento sistematico e strutturale dello psicologo scolastico negli istituti di ogni ordine e grado. Questo Piano parla di futuro e senza bambini non ci può essere futuro. *(Applausi)*. PRESIDENTE.

Essere in Europa, sì, ma da protagonisti, non da comparse pagatrici. Non siamo gli alunni un po' discoli da bacchettare e accontentare ogni tanto; siamo un Paese fondatore di quello che era un sogno e che vorremmo continuasse a essere tale e non già una gabbia o un vincolo da cui potersi e doversi liberare.

Tra i dimenticati ricordo i 5 milioni di italiane e italiani portatori di disabilità. Un Paese civile non può avere cittadini di serie B né a scuola, né sul lavoro. *(Applausi)*. Sono

speciali che meritano qualcosa in più e non qualcosa in meno. Mi riferisco all'abbattimento di barriere architettoniche nelle biblioteche, nei musei, nelle scuole, lungo le strade, nei palazzi, sui treni e sugli autobus, centinaia di milioni di euro investiti per offrire un lavoro vero a donne e uomini che non chiedono compassione, né elemosina e che si sentono una ricchezza per questo Paese. che la disabilità, anche in questo piano ambizioso, non sia vissuta, a pagina 385, come una postilla obbligatoria da inserire non si può fare. Abbiamo chiesto e ottenuto - la ringrazio anche per questo - un Ministero appositamente dedicato alle donne, agli uomini, ai giovani e agli anziani

non udenti e disabili fisici e psichici significa che questo è un Paese che guarda davvero avanti. Per questo la ringrazio, Presidente, e vedremo di usare bene

i cantieri durano in media, dall'inizio alla fine, 815 giorni, ossia quasi un anno in più rispetto alla media europea. Siamo penultimi in Europa, davanti solo alla Grecia, per lunghezza, burocrazia

noi invochiamo la direttiva europea sui ritardati pagamenti per dare ossigeno alle nostre imprese. E ricordiamo e invochiamo anche (e qui vedremo

l'azzeramento e la sospensione della normativa italiana sugli appalti, sostituita dalla ben più efficace ed efficiente normativa europea. *(Applausi)*. Azzeriamo il codice degli appalti italiano e utilizziamo la normativa europea. Viva l'Europa sui tempi di pagamento e sugli appalti veloci. Vediamo se dai banchi della sinistra ci sarà tutto questo euroentusiasmo anche quando si tratterà di tagliare alcuni artigli, alcune lunghezze e alcune autorizzazioni all'interno delle quali si nasconde la corruzione. Perché più lungo è il processo di un appalto, più facile è trovare un corrotto e un corruttore. Se velocizzeremo i tempi sul modello Genova, vedrete che ruberanno di meno

Noi abbiamo risposto all'appello del presidente Mattarella, mettendo prima l'Italia rispetto all'interesse di partito e se qualcuno pensa di buttarci fuori ha sbagliato a capire. Noi qua siamo e qua rimaniamo orgogliosi e convinti per aiutare il nostro Paese.

C'è stato un dibattito di giorni e di ore sulle riaperture e sul coprifuoco. La ringrazio perché chi stamattina ha potuto andare a bere un caffè seduto al bar l'ha fatto per una scelta di coraggio, per un rischio calcolato. Giustamente, nell'ultima settimana 4.000 italiani hanno lasciato i posti letto degli ospedali, 500 sono usciti dalle terapie intensive e 3 milioni di Italiani sono stati vaccinati.

la ringrazio per questo Piano ambizioso, presidente Draghi. La ringrazio anche per aver superato ritardi accumulati da qualcuno che, per mesi, evidentemente ha sonnecchiato. Quindi, siamo arrivati meglio degli altri e prima degli altri. a fidarsi di chi ha il coraggio di difendere le proprie idee, anche assumendo posizioni scomode, e di diffidare invece di chi dice sempre e solo sì, non per amor di Patria, ma per amor di poltrona. Grazie, Presidente, e viva l'Italia.

Signor Presidente, un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno lavorato su questo Piano e che continueranno a lavorare per dargli una corretta definizione e soprattutto una rapida attuazione. Abbiamo bisogno, infatti, di fare in fretta, ma soprattutto, signor Presidente, di fare bene. estremamente necessaria per il nostro Paese, per le future generazioni e per i nostri giovani. *(Applausi)*. Questo Piano, però, era una cosa impensabile fino a marzo 2020, nel senso che, per fortuna, abbiamo avuto il presidente del Consiglio Conte, che, grazie anche all'impegno di altri Stati membri, è riuscito a convincere l'Unione europea a impegnarsi e a indebitarsi per tutti i Paesi in difficoltà, come il nostro, con uno strumento comune. Questa era una cosa impensabile

ma non presenta quelli che sono i progetti esecutivi. Noi abbiamo bisogno di avere contezza delle cose precise che verranno fatte, ma soprattutto dei luoghi in cui verranno fatte cui verranno fatte e questo, purtroppo, ancora non c'è. Signor Presidente del Consiglio, su questo chiediamo un impegno del Governo a farci avere quanto prima il progetto completo con i dettagli perché qui abbiamo solo contezza delle missioni e delle componenti, ma sulle azioni singole abbiamo veramente poco. Veniamo a una cosa particolare. Noi ci siamo sempre espressi nei confronti del Governo in modo ampio tramite delle risoluzioni, degli atti che impegnano il Governo e non siamo mai riusciti a esprimerci in modo diretto con delle cose da fare in modo condizionato

Andiamo oltre perché sono sicuro che da qui all'esecuzione di questi lavori si dovrà ripassare dal Parlamento, almeno in sede di legge di bilancio. Qualcosa dovrà passare dal Parlamento perché dobbiamo avere contezza di ciò che verrà fatto e dobbiamo approvare soprattutto ciò che verrà fatto. Quindi, immagino che in un futuro non troppo lontano

perché per l'ambiente dobbiamo fare molto. Purtroppo, in Italia abbiamo inquinato tanto nei decenni precedenti. Ora abbiamo bisogno di una vera rivoluzione e purtroppo, Presidente, mi scusi, non ci sono ancora elementi sufficienti per dire che questa transizione ci sarà. *(Applausi)*. Purtroppo, è così

Ora c'è, ma le risorse non sono ancora abbastanza. Bisogna fare di più e spero - visto che ci sarà un fondo aggiuntivo - che buona parte di quelle risorse potranno essere usate per l'ambiente. Non possiamo più continuare, infatti, a piangere le morti delle persone che si sono ammalate di tumore perché vivevano in un'area inquinata. Presidente, su questo dobbiamo fare assolutamente di più. Veniamo al capitolo della non autosufficienza. Presidente, veramente cerco di fidarmi perché nel Piano precedente sulla non autosufficienza vi era una parte che che contava 3,3 miliardi. Ora sulla prima componente di quella missione siamo scesi a circa un miliardo, però c'è molto di più sulla qualità dell'abitare e sull'*housing* sociale. Ci sono circa 3 miliardi in più, però le persone che hanno bisogno veramente necessitano di servizi assistenziali, di qualcuno che li vada a trovare per farli stare bene e, quindi, non possiamo investire solo sul mattone.

Ha facoltà di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, professor Draghi.

questo Senato è stato protagonista nel disegno, attraverso le molte consultazioni fatte nei mesi scorsi, attraverso le osservazioni di cui abbiamo tenuto conto. Sarà protagonista nell'attuazione del Piano, quindi, credo che molte delle osservazioni fatte richiamino giustamente la scarsità dei tempi che c'è stata. Ho ricordato in altre occasioni che il 30 aprile non è una data mediatica; è una data per avere subito i soldi. di presentare il Piano il 10 maggio i soldi li avremmo avuti dopo, non so se a giugno o addirittura dopo l'estate. Quindi, ecco il motivo dei tempi molto stringenti. Tra l'altro, non ho mai detto «garantisco io»: non è il mio stile. Al centro del Piano c'è l'Italia, con le sue straordinarie qualità che ci rendono orgogliosi e anche le sue ormai storiche fragilità, su cui credo che tutti siamo d'accordo. Occorre trovare ora il consenso per affrontarle e risolverle. Questo piano ci dà l'occasione per farlo.

dobbiamo lavorare insieme, e quando dico insieme non intendo soltanto qui dentro, ma insieme con il Governo, con gli enti locali, con tutto il popolo italiano.

No. I cambiamenti avranno effetti certamente economici ma anche sociali importanti, e si possono attuare soltanto se c'è accordo, se c'è volontà di successo, non di sconfitta. Ciò che ci sta davanti è molto complesso: le riforme, l'impianto istituzionale, Ministeri, Regioni, Comuni, Province, e poi la vera e propria messa a terra, come si dice. Dicevo stamattina che corruzione, stupidità, interessi costituiti continueranno a essere i nostri nemici e ribadisco che sono certo che saranno battuti è l'inerzia. Mi riferisco all'inerzia istituzionale che si è radicata nei nostri comportamenti anche per la stratificazione di norme che ha accompagnato gli ultimi trent'anni. Queste riforme ci aiuteranno a superarla e per questo sono così importanti. Tornando

Ricordiamoci che le riforme saranno adottate con strumenti legislativi, disegni di legge, leggi delega, decreti-legge, nei cui procedimenti di adozione il Parlamento tutto avrà, come è ovvio, un ruolo determinante nella discussione e nella determinazione del contenuto. Quindi, ancora una volta la collaborazione tra il potere legislativo ed esecutivo è cruciale in questa prospettiva.

conto ci fa vedere che non ci sono solo le risorse del Piano, ma il Mezzogiorno dispone di un complesso di risorse, provenienti da diverse fonti di finanziamento. Il PNRR e il fondo complementare destinano al Mezzogiorno circa 82 miliardi di euro su 206 miliardi di euro totali, delle risorse ripartibili su base territoriale; il 40 per A queste risorse però si aggiungono quelle dello strumento React-EU, appositamente attivato dall'Unione europea per contrastare gli effetti della crisi pandemica. Su un totale di 13,5 miliardi di euro destinati all'Italia, al Mezzogiorno andranno 8,5 miliardi di euro, destinati in larga parte a realizzare iniziative nel settore delle politiche del lavoro e dell'inclusione sociale, della salute e della ricerca. Le aree del Mezzogiorno potranno inoltre beneficiare delle ingenti risorse stanziate dal bilancio dell'Unione europea per i fondi strutturali 2021-2027 e i fondi per lo sviluppo rurale e la pesca: unitamente alle corrispondenti risorse del cofinanziamento a carico del bilancio statale, al Mezzogiorno andranno circa 60 miliardi di euro, su 85 Queste risorse saranno destinate a realizzare interventi in molteplici settori: ricerca, innovazione, tecnologie digitali, sostegno dell'economia a basse emissioni di carbonio, gestione sostenibile delle risorse naturali, sistema delle imprese, occupazione, scuola, Le aree del Mezzogiorno potranno inoltre beneficiare, per la realizzazione dell'Alta velocità, la linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, di ulteriori risorse, pari a 9,4 miliardi di euro, su un totale di 10,4 miliardi Si tratta delle risorse reperite con lo scostamento di bilancio approvato dal Parlamento nei giorni scorsi, saranno incluse nel prossimo decreto-legge sul Fondo complementare e saranno aggiuntive al fondo stesso. Ulteriori risorse provengono dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, con questa ripartizione: nella programmazione per il 2014-2020, sono previsti 24 miliardi di euro per il Sud, su un totale di circa 30,

ricostituzione delle risorse per il 2021-2027 utilizzate nel PNRR, per 12,4 miliardi di euro al Sud, su un totale di 15,5 su scostamento di bilancio approvato dal Parlamento nei giorni scorsi, che saranno incluse nel prossimo decreto-legge sul Fondo complementare. Naturalmente sarà importante evitare che i programmi straordinari siano compensati da una riduzione della spesa ordinaria, ma detto questo, qual è la lezione che si trae? La prima lezione che si trae è che il Sud non è stato discriminato in questo afflusso di fondi. Si potrà far meglio, si potrà cercare di riparare a qualche mancanza in tutta questa congerie di di sorgenti e di fondi, ma sostanzialmente l'impressione non è quella di una discriminazione colpevole. La seconda lezione è che le risorse saranno sempre poche, se uno non le usa. Questo è il punto. Per usarle, certamente le riforme aiuteranno, ma ma c'è veramente una storica inerzia che bisogna superare, che non è colpevole, ma è un'inerzia che si vede, soprattutto nella fase di progettazione. Quindi, anche su questo bisogna impegnarsi collettivamente e il Governo ha previsto nel PNRR la costituzione di gruppi di lavoro che possono essere di aiuto, in questa fase, naturalmente se graditi.

Oltre 1,2 miliardi, pari al 44 per cento del totale territorializzato, appaiono destinati ai principali porti del Mezzogiorno per interventi portuali propriamente detti e altri interventi per la resilienza delle strutture portuali contro il cambiamento climatico. Questi sono interventi fatti con risorse nuove e non attraverso la programmazione del Fondo di coesione e sviluppo. Ci sono poi 630 milioni di interventi per le aree retroportuali e industriali comprese nelle zone economiche del Mezzogiorno, che andranno a incidere, tra l'altro, proprio sui principali nodi logistici e portuali del Sud: Napoli, Taranto e Gioia Tauro. Per Gioia Tauro è inoltre previsto nel contratto di programma il finanziamento per oltre 60 milioni di euro per il collegamento del porto alla rete regionale ferroviaria. Sull'Alta velocità, ho detto prima dei 4,640 miliardi che copriranno i primi lotti funzionali di Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina-Catania e Roma-Pescara. Altri 4,9 miliardi circa sono previsti per le connessioni diagonali, come la Battipaglia-Taranto e per il potenziamento di linee e stazioni ferroviarie meridionali. È molto rilevante sottolineare che al Fondo complementare da 30 miliardi si aggiungono ulteriori 9,4 miliardi, risorse necessarie per i successivi tre lotti della Salerno-Reggio Calabria, come ho detto prima. il bando per l'assegnazione ai Comuni dei primi 700 milioni di euro per gli asili nido è stato indetto sulla base di una norma della scorsa legge di bilancio. I criteri di riparto di queste risorse riservano il 60 per cento del totale alle aree svantaggiate, in gran parte quelle del Mezzogiorno, delle zone periferiche delle grandi città e delle aree interne. Per i prossimi bandi sarà evidentemente necessario correggere gli eventuali elementi di debolezza che riscontreremo con questo bando. L'obiettivo - ricordiamo - è dotare l'intero Paese di un'infrastruttura sociale che renda possibile il raggiungimento dell'obiettivo europeo del 33 per cento di bambini coperti da un servizio essenziale per le famiglie e per l'occupazione femminile. C'è stata poi una domanda sui criteri di assegnazione dei fondi *recovery*, la famosa cantierabilità come criterio di selezione. Sì, è vero che l'Italia ha ottenuto la quota più significativa di fondi europei proprio perché c'è un'ampiezza dei divari territoriali da colmare, ma è anche vero che l'Unione europea chiede di ridurre tali divari (territoriali, di genere, generazionali) con azioni effettive e riforme efficaci, e non con una mera ripartizione contabile delle risorse. Il nostro obiettivo con il Piano è ridurre questi divari e le stime sulla crescita e l'occupazione che ho dato prima e che il Piano produrrà testimoniano la bontà di questa visione. Il PNRR però - ricordiamolo - ha un vincolo di utilizzo di cinque anni. Non è un alibi, è un dato di fatto; deve tener conto anche delle storiche difficoltà del Sud di assorbimento dei fondi pubblici.

sono d'accordo con tutto quello che ha detto e, quindi, non ho risposte specifiche, se non rimarcare che il suo invito di procedere all'assegnazione dei fondi attraverso procedure competitive è stato pienamente accolto, anche nella costituzione dei centri di ricerca. Non ci sono più numeri; si creano soltanto se si vincono i bandi. Più fondi alla ricerca su base ordinaria: certamente, e su questo si tornerà nella prossima legge di bilancio. Quanto al secondo punto, e cioè al fatto che c'è un nesso tra riforme e politiche economiche, politiche monetarie e fiscali, sono stato spesso rimproverato, avendo inaugurato una politica monetaria più espansiva, di aver rimosso gli stimoli per i Governi a fare le riforme. Questa è un'accusa che mi è stata spesso rivolta, perché si crede che le riforme si facciano solo strozzando i Paesi con gli alti tassi di interesse. Ma questo non è vero, poiché non c'è alcuna relazione tra riforme e tassi di interesse, tanto è vero che oggi facciamo le riforme e le faremo con i tassi pari a zero. Perché questo? C'è il PNRR che inaugura una diversa stagione di politica fiscale, di politica di bilancio a livello europeo. Si tratta di una scommessa che facciamo collettivamente in tutta Europa sulla capacità di spendere - ma soprattutto di spendere bene - questo denaro. Questa scommessa vede l'Italia in prima fila come il Paese che ha tirato di più su questo Fondo (forse la Spagna qualcosa di più). Quindi noi saremo in un certo senso responsabili del successo o della perdita di tale scommessa. Una sconfitta su questo fronte è grave, prima di tutto perché i primi a pagarne il prezzo saremo noi. Ma è grave anche per il futuro dell'Europa, perché non ci sarà più possibilità di convincere gli altri europei a fare una politica fiscale comune, a mettere i soldi insieme. Voglio ricordare che mettere i soldi insieme e fare una politica fiscale comune

sono su connessione e connettività. Comincio dalla banda larga: il Governo intende stanziare 6,31 miliardi per le reti ultraveloci, la banda larga e il 5G; l'obiettivo del Governo è portare entro il 2026 reti a banda ultralarga ovunque, senza distinzioni territoriali ed economiche. - avviamo la mappatura dei piani di investimento previsti dai privati per identificare le aree del Paese che, senza interventi del Governo, resterebbero sfavorite. Per queste aree è previsto un contributo statale per assicurarci che non si creino nuovi divari digitali da qui al 2026. Vogliamo che si evitino duplicazioni di investimento, che gli operatori di mercato scelgano le tecnologie più adatte ad ogni zona, e che comunque la scelta dei cittadini e la concorrenza vengano tutelate. Grazie a questa nuova e completa infrastruttura intendiamo investire per ammodernare la nostra amministrazione, connettere tutte le scuole e gli ospedali, incentivare le imprese a investire e digitalizzarsi. La semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni è un obiettivo essenziale per la riuscita del Piano più in generale, per il rilancio del settore delle costruzioni. In merito agli appalti, intendiamo riformare la disciplina nazionale sulla base delle tre direttive dell'Unione europea 2014/24 e 2014/25, per renderla più snella rispetto a quella vigente, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri dell'Unione europea.

A prescindere dal PNRR, la semplificazione normativa e amministrativa è un obiettivo cruciale per il Governo. Il PNRR di per sé contiene molte misure per accelerare l'attuazione degli interventi. Le riforme previste nel Piano sono poi accompagnate da indicazioni sulle tempistiche: sarà approvato un altro decreto-legge a maggio con gli interventi urgenti di semplificazione, e questo lavoro proseguirà in maniera progressiva e costante fino al 2026.

hanno espresso punti di vista diversi: per il senatore Dal Mas spendiamo troppo, per il senatore Balboni spendiamo poco.

la Francia ne ha 3; eppure la Germania ne ha 7, il Regno Unito ne ha 8,6 e la Spagna ne ha 5. Anche qui è importante investire, è importante spendere ed è importante anche aumentare gli organici, ma è importante farlo bene. Quindi, la qualità del capitale umano che si accumulerà nei prossimi mesi e anni è molto importante.

Chiedo al sottosegretario Amendola di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

presidente Draghi, questo è un giorno davvero importante per l'Italia. Oggi discutiamo del progetto che può davvero consentire al Paese di sciogliere nodi e ritardi che ne hanno strozzato la crescita e la competitività per più di vent'anni tutto questo è possibile grazie all'Europa. È il più grande Piano di aiuti dai tempi del Piano Marshall, che vede l'Italia come principale beneficiaria, perché ha posto criteri che fotografano fedelmente le fragilità economiche e sociali legate alla pandemia. Si è affermata cioè l'idea che davanti a una tempesta di così vaste proporzioni gli ordinari strumenti di gestione politica e monetaria sarebbero risultati inadeguati. Occorreva un salto in avanti, un cambio di schema di gioco, mandando in soffitta le regole e i dogmi che avevano caratterizzato negativamente la gestione dell'ultima crisi economica, perlomeno fino al momento in cui, sotto la sua guida, non ci fu quel vasto intervento per salvare l'euro e le economie nazionali. il Covid bisognava intervenire nell'economia reale, sospendendo il Patto di stabilità e dando ai Paesi la possibilità di fare nuovo debito. Allo stesso tempo occorreva uno slancio di visione, quello che ritroviamo nelle missioni indicate nel *recovery plan*, in grado di trasformare questa catastrofe umana, economica e sociale in un'opportunità per costruire società più giuste ed economie più solide. Per questo, Presidente, la responsabilità è doppia. Abbiamo un debito morale nei confronti dell'Europa, per il fatto che da questo momento, attraverso il *recovery si può riaccendere il percorso per una sempre maggiore integrazione, attraverso un bilancio comune e la stabilizzazione di misure votate all'innovazione. Dobbiamo riuscirvi mettendo subito in campo quelle riforme che sono state indicate nel Piano. Servono interventi coraggiosi per spingere l'economia e far crescere i livelli occupazionali. Serve un grande patto tra tutti gli attori politici e istituzionali, le forze sociali, i corpi intermedi, gli attori economici, affinché il percorso delle riforme non sia viziato da rivendicazioni di parte, e affinché in esso tutti remino per centrare gli obiettivi. una riforma della pubblica amministrazione per innalzare qualità e capacità di spesa, attraverso l'immissione di figure che, dal giorno stesso, sappiano cosa fare, nonché attraverso un progetto per una formazione che accompagni i dipendenti pubblici in ogni fase del loro percorso lavorativo. una riforma del fisco, per stabilire un nuovo patto con i cittadini; un fisco finalmente chiaro nelle regole che, con il riordino delle varie misure, consenta davvero di alleggerire la pressione, in particolare sul costo del lavoro. una riforma della giustizia civile, che ripristini la certezza del diritto e la giusta durata dei processi, che oggi fa perdere all'Italia un punto del PIL all'anno e rappresenta il principale freno per gli investitori stranieri. Ma ci vuole anche una vera e propria campagna per l'occupazione, attraverso un sistema formativo che favorisca l'incontro tra domanda e offerta, puntando anche sugli istituti tecnici, sulle scuole professionali, su quel sistema duale che, almeno in Sudtirolo, è stato di grande importanza per i livelli di occupazione giovanile prima della pandemia *(Applausi)*, rafforzando le strutture per l'infanzia e favorendo misure di conciliazione tra famiglia e lavoro. Il livello del tasso di occupazione, in effetti, è direttamente proporzionale al benessere di una società. Signor Presidente, è una scelta giusta quella di lasciare alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali la responsabilità di quasi metà dei progetti, nel rapporto 60/40, che lei ieri e oggi ha sostenuto. È la scelta che dà maggiori garanzie di equilibrio e mette al riparo dai rischi di ingolfamento di una struttura troppo centralizzata e da quelli di sovraccarico per le amministrazioni locali. In questo quadro è molto positivo il rafforzamento delle risorse per la ricerca, le politiche attive del lavoro, l'innovazione tecnologica, nonché il forte impegno per la cultura e il turismo, per la competitività dell'intero tessuto produttivo, per le infrastrutture strategiche, con la nomina, già nelle scorse settimane, dei commissari straordinari. Apprezziamo altresì la volontà di non escludere quei progetti ritenuti indispensabili per l'ammodernamento del Paese, ma che non rientravano nella tipologia di progetti finanziabili con le risorse europee. Si tratta, Presidente, di un segnale politico importante, di chi non vuole limitarsi a sfruttare le risorse europee, ma intende inserirle in un ragionamento complessivo sul futuro del Paese. Adesso, Presidente, viene la parte più difficile, ma anche più entusiasmante. Lei lo ha detto con quel linguaggio della franchezza che la contraddistingue e noi in questo saremo con lei, per semplificare le norme, per scrivere le riforme, per fare in modo che non un solo euro vada disperso. Lo dobbiamo fare e nel frattempo dobbiamo spingere al massimo la campagna vaccinale, per fare in modo che da qui possa passare un ulteriore allentamento delle misure restrittive, anche mettendo in campo strumenti, come quello che abbiamo avviato in Sudtirolo, che ci possano avvicinare sempre più alla normalità. Oggi si scrive una pagina importante. Il Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) esprime il voto favorevole sul PNRR e le augura buon lavoro.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio dei ministri, onorevoli colleghi, è stato il Piano nazionale di ripresa e resilienza a costituire il *casus belli* che ha portato alla crisi del Governo Conte e alla nascita del Governo guidato dal presidente Draghi. L'onestà intellettuale vuole che oggi si dia una risposta alla seguente domanda: ne valeva la pena? È cambiato qualcosa? Io penso che, per chi ha letto il testo del 9 dicembre del precedente Governo e chi ha sentito l'intervento del presidente Draghi oggi, la risposta sia chiara. Molto è cambiato, ma non mi riferisco a singole aggiunte o modifiche; mi riferisco a una cosa che allora non c'era e che oggi c'è: un'anima, una direzione, una visione. Questo elemento è evidente oggi nel dibattito mondiale, nel dibattito europeo e deve diventare oggetto di discussione tra di noi. Non è un fatto legato alla stampa internazionale: è un po' provinciale guardare la stampa internazionale e pensare che essa sia la depositaria della verità. il sentimento che il futuro in Italia è tornato in buone mani è un elemento che c'è nel dibattito dei *leader* internazionali, sui mercati e nelle aspettative verso il nostro Paese. Di fronte a questo elemento, signora Presidente, c'è un dato di fatto oggettivo: il *recovery plan* non è uno, ma son due. Voi vi com'è possibile che ciò avvenga. In realtà, accanto ai 200 miliardi che vengono in qualche misura incanalati dall'Europa - il presidente Draghi nella sua replica ha dato anche una lezione tecnica, oltre che politica, sul valore per il futuro di questo investimento - c'è una cifra più o meno analoga, di cui non si parla mai, che Banca d'Italia stima essere nei depositi e nei conti correnti del risparmio degli italiani (imprese e famiglie) che hanno iniziato a risparmiare dal primo giorno della pandemia. una cifra che viaggia tra i 170 e i 200 miliardi di euro. È come se le risorse fossero doppie: da un lato i 200 miliardi europei, ma dall'altro un *recovery plan* totalmente italiano bloccato dalla paura. Recuperare parole di fiducia, signora Presidente, è dunque una priorità anche economica. Recuperare un clima di fiducia passa anche da gesti simbolici, come non litigare su un orario del coprifuoco, ma prendere atto che è fondamentale procedere con l'allargamento delle riaperture, perché questo porta a investire il denaro degli italiani ed attrarre i denari non soltanto delle aziende, ma anche dei turisti. Questo elemento è una pietra miliare nella storia del nostro Paese. lei è appena arrivato in quest'Aula e non ha potuto gustare tutti i riferimenti a quante volte abbiamo scritto la storia in questa legislatura: una volta alla settimana nel corso dei tre anni precedenti qualche Ministro ha fatto un *post* dicendo che stava scrivendo la storia. Questo è valso sia col Governo Conte 1 che con il Governo Conte 2. Bastava stare applicati ai *social* e si trovava sempre qualche Ministro: il primo è stato un ex Ministro che ha detto che scriveva la storia perché stava trasferendo le competenze dell'unità sul dissesto idrogeologico e sull'edilizia scolastica ai rispettivi Ministeri; poi qualcuno ha scritto la storia affacciandosi da un terrazzino e abolendo la povertà con il reddito di cittadinanza; poi qualcuno ha scritto la storia con i provvedimenti più disparati. Io penso che nessuno abbia scritto la storia in questi tre anni. tre anni. È certo però che pochi la storia l'hanno studiata. Gli anni Venti del secolo scorso hanno preso avvio con una terribile pandemia, la spagnola, che ha fatto più morti - si spera di quelli che farà alla fine il coronavirus, ma per la incapacità delle classi dirigenti si sono prodotti due elementi: la crisi delle traballanti democrazie dell'epoca la depressione economica culminata nel 1929, alla fine di quel decennio degli anni Venti, in una delle più grandi tragedie della storia economica contemporanea e recente. Io vorrei che noi avessimo la consapevolezza che nessuno qui può scrivere la storia semplicemente perché fa un decreto o un piano, ma che c'è la consapevolezza di dover presentarsi all'appuntamento della storia con la consapevolezza di chi ha imparato dalle lezioni del passato. In questo senso il Governo Draghi

in Unione europea negli ultimi dodici mesi. Nel 2020 ad aprile sembrava che l'Unione europea avesse colto il valore della ripartenza e che il Regno Unito con Boris Johnson, che allora era anche in un momento di difficoltà personale, non avesse capito praticamente niente. Invece cosa è accaduto dopo un anno? La campagna vaccinale ha visto il successo degli inglesi anche rispetto all'Unione europea e piange il cuore a me che sono europeista vedere come la campagna vaccinale sia diventata uno *spot* per coloro i quali sostengono la Brexit rispetto al mal funzionamento dell'Unione europea. La storia cambia velocemente, e anche quella del nostro Paese. Se prendiamo il compasso e torniamo indietro, il 27 aprile del 2016, c'era un Governo - io ne so qualcosa - che sembrava destinato ad avere consenso per anni. Nell'aprile del 2017 il presidente del Consiglio Gentiloni sembrava destinato ad essere il punto di riferimento di un equilibrio di larghe intese per anni. Nell'aprile del 2018 sembrava che si dovesse fare un Governo guidato dall'onorevole Di Maio con il PD come sostegno. Nell'aprile del 2019 sembrava che il Governo Conte 1 non potesse fare a meno della *leadership* di Salvini. Nell'aprile del 2020 nessuno poteva toccare il Governo Conte 2. Nell'aprile del 2021 credo che vi sia una guida del Governo capace di cogliere il valore strategico di un progetto di lungo periodo e non di un orizzonte che divora i personaggi politici.

che l'Italia ha un Governo che pensa alle future generazioni e non alle future elezioni, che finalmente possiamo andare sui giornali internazionali non perché abbiamo i banchi a rotelle nascosti nei magazzini che non servono o perché abbiamo o perché abbiamo i ventilatori cinesi malfunzionanti, ma garantiti degli amici degli amici. *(Applausi)*. Abbiamo finalmente l'occasione di andare sui giornali di tutto il mondo come quelli che presiedono il G20 con una visione post pandemica; come quelli che hanno qualcosa da dire sull'Unione europea che verrà, anche adesso, ma a maggior ragione dopo che Angela Merkel lascerà, e in un momento di grande tensione per la Francia, che va verso una campagna elettorale difficile. Siamo quelli che possono restituire entusiasmo e fiducia a condizione di provare, signor Presidente, a mettere in pratica le sue parole. Lei ha detto che l'onestà, l'intelligenza e il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, la stupidità e gli interessi costituiti. Siamo tutti d'accordo sull'onestà contro la corruzione; sull'intelligenza contro la stupidità, De Gaulle lo definiva vasto programma, ma è una sfida comunque affascinante e suggestiva; intelligenza artificiale o naturale che sia, siamo tutti con lei. che però - secondo me - arriva dalle parole del presidente Draghi è quella relativa al gusto del futuro contro gli interessi costituiti. Questa è la vera anima del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si dice - lo ha detto il Presidente - ai ragazzi che possono puntare a studiare nei luoghi migliori con i maestri migliori. Si dice alle imprese che non devono aver paura di sfidare il futuro, perché possono giocarsela contro la cultura della rendita. Si dice però anche alla politica che forse è arrivato il momento, per una volta, di avere un orizzonte più ampio, di pensare sul serio che il gusto del coraggio e del futuro sia più forte di chi in questi anni ha sempre pensato di poter andare avanti con la cultura della rendita e con la paura del domani.

Signor Presidente, presidente Draghi, colleghi, nonostante le sue giustificazioni, io credo che nessuno possa negare che stiamo discutendo e votando un Piano che il Parlamento il Parlamento non conosce. Lo conosce sicuramente il Governo; lo conoscono i capi delegazione dei partiti; lo conoscono sicuramente i burocrati zelanti di Bruxelles, ma non lo conosce il Parlamento della Repubblica italiana, che è costretto a votarlo a scatola chiusa secondo una procedura che credo non sia mai stata così avvilente per il suo *status*. Diciamo questo, presidente Draghi, non per amore di polemica fine a se stessa e nemmeno per difendere il ruolo dell'opposizione. Lo diciamo per difendere il ruolo della politica, il ruolo del Parlamento, paradossalmente per difendere anche i colleghi di maggioranza, di cui immagino l'imbarazzo, dovendo votare qualcosa che non conoscono, che non hanno potuto nemmeno leggere. nemmeno leggere. Qualche tempo fa si diceva che il Parlamento era una scatola di tonno da aprire. Il Parlamento è diventato un inutile soprammobile. Presidente Draghi, forse a lei interesserà poco o addirittura dispiacerà, ma il sottoscritto

che indebita i nostri figli e i figli dei nostri figli, senza averlo potuto leggere, commentare, migliorare, emendare. E diremo a futura memoria che tutto questo è avvenuto con il silenzio di tutti, tranne che del Gruppo Fratelli d'Italia.

ma anche di alterare le regole elementari del gioco democratico e che considera la presenza di una forza di opposizione coerente come un fastidio e non invece per quello che è, ovvero una garanzia di libertà e di pluralismo. Venendo al merito della discussione sul Piano nazionale di ripresa e di resilienza, certamente non vogliamo né sottovalutarlo né minimizzarlo, ne conosciamo l'ampiezza, la portata e l'importanza. La presidente Meloni, nei colloqui che abbiamo avuto, ha anche inviato dei documenti scritti e ha elencato quelle che sono per noi le priorità. Ma non possiamo non vedere - ad esempio - che mancano tutte le riforme che - lei mi insegna, presidente Draghi - devono accompagnare il Piano. Manca la riforma della giustizia, manca la riforma del fisco, manca la riforma della pubblica amministrazione e, senza delle riforme, questo Piano viaggia con il freno a mano tirato. Dirò poi una cosa che sicuramente è molto contro corrente, ma credo che dobbiamo fare un bagno di realismo e di prudenza, perché ho sentito troppi voli pindarici. è certamente una grande occasione per il nostro Paese, ma non è una bacchetta magica che in un colpo solo risolve tutti i problemi del Paese. Abbiamo a disposizione 220 miliardi, che sono diventati 250, che potremo utilizzare nell'arco di sei anni; probabilmente i primi effetti si dispiegheranno l'anno prossimo; abbiamo letto le stime di crescita che avete scritto nel DEF e le consideriamo - come tutte le stime di crescita macroeconomica scritte dai Governi - molto ottimistiche, e speriamo di sbagliare. Ma dobbiamo anche - per amore di verità ricordare che, a fronte dei 220 miliardi in sei anni del *recovery plan*, in dodici mesi ne abbiamo già spesi 180 di scostamento di bilancio e i risultati, o meglio i non risultati sono sotto gli occhi di tutti, Presidente, compreso il fatto che buona parte di quelle risorse è ancora ferma ai Ministeri perché mancano i decreti attuativi. *(Applausi)*. Prima di occuparci del *recovery plan*, allora, occupiamoci di usare le risorse che già abbiamo e che non riusciamo a spendere. Lei, Presidente, ci ha spiegato che questo Piano deve servire a rinnovare, a cambiare, a modernizzare il Paese, tutte cose che noi condividiamo e che ci auguriamo possano accadere.

Altrimenti, presidente Draghi, sul terreno di un'economia e di una società distrutte, non funzioneranno nemmeno i miliardi del *recovery plan.*

più. Siamo vicini a quel punto molto delicato e pericoloso in cui il dramma sociale e l'emergenza economica rischiano persino di travolgere l'allarme sanitario.

la cosa più straordinaria, sempre in termini di realismo e pragmatismo, è che tutta questa gente

dal più umile al più prestigioso, che si può contribuire non solo alla realizzazione di se stessi, della propria famiglia e della propria comunità, ma anche a ricostruire la speranza e la fiducia in questo Paese

di chi ha sofferto in silenzio e di chi crede ancora nel merito e nel talento; sicuramente non a beneficio di chi crede che il futuro si conquisti pescando il biglietto fortunato della lotteria degli scontrini,

ore 22 che colpisce a morte il nostro turismo? Lascio a lei la risposta, presidente Draghi. Nonostante tutto, i torti e gli errori, noi continueremo lungo la nostra strada, che è quella di un'opposizione senza sconti e pregiudizi. Noi non siamo quelli del tanto peggio, tanto meglio: siamo quelli del tricolore e continueremo sempre e comunque a tifare per l'Italia, perché almeno questa libertà di sicuro non ce la potrete togliere. Grazie, Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, ogni storia, come quella che stiamo vivendo oggi, ha un suo inizio. E, se oggi siamo qui a discutere dei 248 miliardi di euro complessivi che l'Europa mette a disposizione del nostro Paese, lo dobbiamo di sicuro al prezioso lavoro di negoziazione della nostra delegazione che il 21 luglio scorso, dopo giorni difficili di trattative, ha contribuito in modo decisivo alla nascita di questo strumento straordinario da 750 miliardi di euro per salvare i Paesi più colpiti dal Covid. uno strumento che segna un cambio di passo decisivo anche per l'Europa, diventata così davvero la casa di tutti. Il *recovery*, infatti, è una grande occasione per l'Italia, ma lo è anche per l'Europa. È un'opportunità unica che abbiamo per poter procedere davvero verso una positiva integrazione solidale, mettendo in campo una politica permanente di condivisione, che implica che i Paesi sappiano tenere il loro debito sotto controllo, rendendo però sostenibile, attraverso una crescita robusta, quello che loro sono. In questo modo, quel Patto di stabilità potrà essere trasformato in un vero patto di sostenibilità, in questo caso ambientale e sociale. Presidente Draghi, io non ho problemi a dire che l'agenda che lei ha delineato è l'agenda dei democratici, perché è un'agenda è un'agenda europeista, che mette al centro le donne, i giovani, il capitale umano, l'ambiente, l'innovazione e le riforme per modernizzare il Paese. Capisco che altre forze facciano più fatica a rivendicare questa affinità e questa visione comune. Sono, tra l'altro, quelle forze che sono state titubanti e anche molto contraddittorie

Noi, invece, non abbiamo mai cambiato idea. Siamo per l'Europa e questa è l'Europa che vogliamo. Con il PNRR si gioca la sfida del futuro e la politica che si intesta la sfida del futuro è la politica che ha il coraggio di non inseguire il consenso facile: del qui e ora e del risultato immediato. Insomma, è la politica che sa cogliere la sfida di questo tempo, che è il tempo della ricostruzione. Per rimettere in piedi il Paese e costruire opportunità, infatti, dal lavoro alla formazione, ci vuole tempo; un tempo più lungo di quello dettato dalle scadenze elettorali, che cercano, appunto, il facile consenso. La differenza tra i populisti e i riformisti è tutta qui. I populisti mettono sempre in campo una visione dominata dall'ansia di dover cavalcare una paura, di dover piantare una bandierina; i riformisti non guardano solo all'emergenza, ma mettono in campo una visione più complessiva per dare risposte al futuro. Signor Presidente, mi consenta di fare un appello alla responsabilità di tutte le forze politiche, affinché si possa parlare più di PNRR e meno delle raccolte di firme per contestare i provvedimenti approvati dal Governo di cui si fa parte. Davvero non è possibile che si facciano battaglie su questioni che sono già risolte, perché sono risolte nella modalità in cui è scritta la norma ciò che è stato detto nella cabina di regia: si deciderà insieme, sulla base dei dati, secondo quello che lei, presidente Draghi, ha chiamato - e va bene per tutti - il rischio calcolato. Allora, le misure andranno di pari passo con quello che sarà il rischio, perché noi vogliamo aprire per non chiudere più. Presidente, l'orizzonte politico delle forze di Governo che hanno la responsabilità di guidare il Paese in questa fase non può essere ridotto alle prossime ventiquattro ore o ai sondaggi settimanali. Se il PNRR è la sfida per il futuro, è chiaro che abbiamo bisogno di avere uno sguardo più lungo. Il PNRR discute dei prossimi anni. Si tratta, però, dell'inizio di un percorso, che mette al centro un metodo e una traiettoria che dovrà essere applicata, da ora in poi, a tutte le misure economiche che anche questo Governo e questo Parlamento si troveranno ad affrontare. crediamo, infatti, che il futuro passi davvero, oltre che dalle transizioni ecologiche e digitali, da quelle tre priorità che abbiamo messo al centro: giovani, donne e Mezzogiorno. Un Paese non può crescere, infatti, se non è in grado di includere e di dare opportunità a tutti. Presidente, lo dico con orgoglio: il Partito Democratico ha chiesto con forza la clausola di condizionalità su tutti i progetti per promuovere occupazione di donne e giovani. Questo indica la volontà di costruire una società più forte ed equa, dove tutti possano partecipare e contribuire alla costruzione di crescita e benessere. Nei prossimi anni dovremo dare al Paese ancora più asili nido di quelli previsti dal Piano, più tempo pieno, più misure per la natalità, in un Paese che non fa più figli e dove le donne sono costrette, troppo spesso, a scegliere tra la maternità e il lavoro e dove i giovani sono precari e senza alcun sostegno per realizzare i loro progetti. Dovremo essere capaci di investire sul capitale umano, sulla creazione di posti di lavoro e sulle politiche attive per riuscire a stare dentro i cambiamenti, che sono imposti da questa transizione. Presidente, ricordo un tema che a noi è particolarmente caro: i nostri ragazzi. Noi non sappiamo veramente cosa questa pandemia stia lasciando in loro. I dati ci dicono che hanno bisogno di sostegno, vicinanza e aiuto per prevenire un disagio psichico che si sta diffondendo. Abbiamo bisogno di intervenire presto. Anche questa è un'emergenza e il Governo

Per fare in modo che diventino una vera opportunità, queste riforme devono essere fatte bene con la centralità del Parlamento, che chiaramente sarà vigile e si intesterà questa grande fase di cambiamento. Noi faremo la nostra parte. Per il Partito Democratico la centralità e il ruolo del Parlamento in questa fase sono ancora più decisivi perché le riforme servono davvero a rimuovere gli ostacoli che hanno rallentato in questi anni la realizzazione degli investimenti. anche le riforme vanno sottratte alle pressioni politico-elettorali. Serve un cambio di passo all'altezza della sfida in atto. Noi ci saremo; riteniamo il Next Generation un successo di chi, come noi, ha sempre creduto nell'Europa e siamo contenti che chi non ci credeva oggi abbia cambiato idea. Il Governo è nato per portare l'Italia fuori dalla crisi. Ricordo bene l'applauso che questa Assemblea le ha riservato nel corso del suo discorso di insediamento quando ha detto che l'unità non era un'opzione, ma un dovere guidato da ciò che ci unisce tutti, l'amore per l'Italia. Sono trascorsi poco più di tre mesi da quel giorno, ma mi pare ci sia bisogno di ricordare a tutti noi presenti in quest'Aula l'impegno cui siamo stati chiamati, perché condividere una responsabilità non significa liberarsi le mani quando si vuole e quando fa più comodo; significa provare a superare le differenze per il bene del Paese insieme, perché nessuno si salva da solo. Lo dobbiamo ai nostri giovani. È questa la vera sfida. Annuncio pertanto il voto favorevole

signor Presidente del Consiglio, colleghi, all'inizio della pandemia ci siamo ripetuti tante volte che niente sarebbe stato come prima ci siamo anche ripetuti molte volte che niente doveva essere come prima, nel senso che la normalità

l'Italia è al centro di questo Piano con la sua bellezza e le sue fragilità. Il nostro compito fondamentale è non tornare a quella normalità che è stata la causa di molti nostri problemi, ma cercare di fare un grande salto in avanti. Credo

che sono state ripetute durante il dibattito: gli assi strategici, per me fondamentali, che si intrecciano strettamente. Sto parlando della transizione ecologica e dell'inclusione sociale, che vanno di pari passo perché intervenire sulle emergenze ambientali significa fare un grande lavoro per abbattere le disuguaglianze e lo svantaggio di tantissime persone. Su questo fronte sono state

sempre - per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è data, e quindi noi ci siamo dati, dobbiamo fare tutti insieme un grande sforzo per implementare le risorse, per raggiungere obiettivi fondamentali e centrali, per far sì che

Non c'è un Piano e poi l'ordinaria amministrazione, Presidente. Tutto il nostro lavoro deve puntare a questo scopo. Bisogna fare di più sulle rinnovabili altrimenti non ce la faremo a raggiungere quegli obiettivi. Bisogna fare di più per abbattere le emissioni. Lei ha parlato giustamente di riforma fiscale: dobbiamo usare anche la fiscalità ambientale, bisogna dirlo con forza, un altro strumento che dobbiamo mettere in campo; anche quella è una grandissima riforma.

Per non parlare del nostro capitale naturale: la bellezza che lei richiamava dell'Italia è la bellezza della nostra cultura, la bellezza dei nostri luoghi storici, la bellezza della nostra natura e biodiversità. Su questo dobbiamo investire perché da lì viene la possibilità di recuperare anche tutte le risorse naturali e l'inclusione sociale. Quindi su questo non solo bisogna avere chiare le condizionalità, che devono essere trasversali, ma dobbiamo

il Parlamento non ha alcuna intenzione di abdicare al proprio ruolo, che è quello di indirizzare, monitorare, controllare e dare il proprio contributo. Le risoluzioni che sono state approvate sono oro prezioso, perché ci servono proprio per fare questo lavoro. Non tutte sono state ovviamente riprese e recuperate nel Piano presentato oggi,

di persone qualificate. Dobbiamo fare una grande riforma per immettere giovani professionalità, perché abbiamo bisogno di una grande capacità di progettazione.

di poco più di un anno dalla tempesta sanitaria ed economica che ha travolto il nostro Paese e l'intero mondo, oggi siamo ad una svolta cruciale e determinante, per il presente e il futuro della nostra Nazione. Nazione non è un concetto astratto, ma indica la somma e la sintesi di tutte le nostre vite, di tutte le nostre comunità e le nostre attività, di tutti coloro che hanno attraversato un momento storico veramente importante, dalla Seconda guerra mondiale ad oggi. Lo hanno fatto pagando davvero in termini anche di perdita di affetti, di lavoro, di reddito e di speranze. A tutti coloro che hanno resistito con pazienta e dignità abbiamo il dovere oggi di dare risposte *(Applausi)*, di indicare l'orizzonte di serenità che meritano. come accadde quarant'anni fa dopo la Seconda guerra mondiale, oggi alla classe dirigente tocca tracciare la strada per uscire da questa crisi e dal dramma della pandemia, dramma della pandemia, e portare finalmente il Paese «a riveder le stelle», per citare il sommo poeta, padre della nostra lingua e della coscienza nazionale, nel suo settecentesimo anniversario. *(Applausi)*.

un ruolo che dobbiamo dimostrare di meritare, come rappresentanti eletti dai cittadini, per dare voce alle loro istanze e tutelare i loro interessi in questo vero e proprio appuntamento con la storia. L'anno 2020, come sappiamo tutti, ha stravolto la vita e la socialità di ognuno di noi. I dati economici sono drammatici

uno scenario di guerra, apocalittico, tant'è che anche il nostro linguaggio è cambiato in questo periodo particolare, perché tutti noi abbiamo parlato di guerra. Oggi siamo qui invece a parlare di dopoguerra e di speranze, perché quello che approviamo oggi è davvero il più grande Piano di rilancio della storia repubblicana. Qualche settimana fa, in un precedente intervento svolto sempre in quest'Aula, ho fatto un confronto tra quello che è oggi il Next generation EU, quindi il *recovery fund*, e quello che è stato negli anni passati, dopo la Seconda guerra mondiale, il Piano Marshall, ossia un grande piano di investimenti per far uscire dalla miseria della guerra - appunto l'Europa. È un raffronto tutt'oggi assolutamente importante da fare, perché negli stessi numeri e nella stessa quantità economica possiamo assolutamente affermare che il *recovery fund* oggi ha una portata di investimenti maggiore anche dello stesso Piano Marshall. Soprattutto, c'è stato un cambio di passo: finalmente un debito che hanno mutualizzato tutti i Paesi europei; è stata una svolta importante. Ecco perché oggi il documento che approviamo ha una portata storica molto, molto importante, unica e straordinaria, può rappresentare veramente il volano, lo sviluppo, la rinascita, la ripresa per il nostro Paese, se utilizzato al meglio. L'opportunità

che abbiamo fatto tutti insieme. Tra le proposte che oggi sono capisaldi dei programmi politici di Forza Italia abbiamo la riforma della pubblica amministrazione. Presidente Draghi, lei ha parlato di inerzia nel suo intervento di replica: noi oggi dobbiamo sburocratizzare il Paese *(Applausi)*, e lo dobbiamo fare con una riforma importante della pubblica amministrazione. Abbiamo poi la riforma della giustizia, che dovrà intervenire sull'eccessiva durata dei processi e puntare a ridurre il forte peso degli arretrati giudiziari. Servono inoltre degli interventi di revisione del quadro normativo e procedurale. Vi è poi la riforma del fisco: anche se non è contenuta

Grazie, presidente Draghi, perché le nostre proposte sono state accolte, come quelle di proroga del superbonus 110 per cento al 2023, che è uno strumento oggi essenziale per rilanciare l'edilizia. Grazie, presidente Draghi, per la proposta sui mutui agevolati al 100 per cento per l'acquisto della casa da parte dei giovani: anche questa è un'opportunità che noi abbiamo proposto per aiutare la famiglia e la natalità nel nostro Paese. Per quanto riguarda altre questioni, come l'IMU e gli estimi catastali, vale il principio in quest'epoca in cui i soldi si danno e non si prendono; quindi, noi siamo contrari a qualsiasi aumento della pressione fiscale. Saremo i guardiani degli immobili dei nostri italiani e non permetteremo assolutamente alcun innalzamento delle tasse sulla casa per gli italiani. Passiamo a quella che è stata una nostra battaglia, il capitolo Mezzogiorno, di cui si è tanto parlato nel dibattito in quest'Aula. Al Mezzogiorno d'Italia il Piano destina 82 miliardi su 206; oltre

alle possibilità che il Mezzogiorno ha avuto con la famosa Cassa del Mezzogiorno e con gli investimenti che tanto sono serviti - e tanto serviranno anche questi - a ridurre il *gap* non soltanto con il Nord, ma con il resto dell'Europa. Per il Mezzogiorno d'Italia è una proposta importante ed è soprattutto un momento un momento per dimostrare finalmente le grandi capacità e qualità del nostro Paese. È una sfida, quella della ripresa economica, importante. La politica oggi si gioca veramente in quest'Aula, con questo piano, la sfida per il futuro e si gioca anche tutta la sua

Per concludere, Presidente, vorrei rifarmi a uno spunto che mi viene offerto da una frase che lei ha pronunciato nel suo intervento in quest'Aula: «nell'insieme dei programmi che oggi presento alla vostra attenzione, c'è anche e soprattutto il destino del Paese».

anche quando non ne abbiamo ancora appresa la natura: il nostro futuro detta le leggi del nostro oggi». *(Applausi)*.

colleghi, oggi ci accingiamo a quello che per qualcuno potrebbe essere definito un passaggio storico, ma che essenzialmente per tutti gli italiani è un passaggio di speranza, di sicurezza, di futuro.

perché dobbiamo sempre ricordarci che ci troviamo di fronte non a una montagna di soldi da spendere, ma a una grande responsabilità nei confronti degli italiani. ha bisogno di essere accompagnata da un approccio franco e pragmatico, convinto e determinato, umile ma autorevole. Questo è fondamentale affinché i risultati siano conseguenti. Il sistema Italia - e lo sappiamo bene - non era ben messo già prima del Covid-19. allora porci delle domande: perché siamo rimasti indietro? Cosa non ha funzionato? Quali regole non hanno funzionato? Quali soluzioni occorrono?

una responsabilità e un'opportunità uniche: riformare il Paese e dare una prospettiva di sviluppo e di crescita alla prossima generazione; ma la crescita deve essere finanziata.

Con queste risorse dobbiamo creare lavoro per gli italiani, crescita e sviluppo. Solo così avremo dato alla prossima generazione non debiti da pagare, ma la certezza che, con il nostro lavoro di oggi, garantiremo loro il benessere futuro, come quello che abbiamo ricevuto dalle precedenti generazioni. Presidente Draghi, queste circostanze ci richiamano al nostro dovere di sacrificio e di impegno per il futuro e per la prossima generazione. Bisogna, però, essere molto chiari: non ci sarà un'altra occasione per riformare il Paese, per riscrivere le regole, per recuperare le distanze interne all'Italia, che negli anni di sprechi non hanno saputo colmarsi. È il momento per togliere lacci e lacciuoli e ce lo siamo detti troppe volte: questo è il momento per farlo, non ci sono scuse per giustificare il mantenimento dello *status quo*. Se ci sono regole che devono essere cambiate, Bisogna, però, stare molto attenti, come lo saremo noi (e chiediamo anche a lei di esserlo, Presidente), affinché le riforme non finiscano nelle mani di quegli apparati autoreferenziali che negli anni hanno spacciato per riforme la propria autoconservazione, producendo un corpo normativo troppo spesso asfissiante e soffocante per l'intero Paese.

ma un meccanismo che asfissia e non lascia sviluppare l'economia. Su questo deve agire in maniera determinata. Noi siamo al Governo per essere determinati in queste riforme e questo ovviamente ci aspettiamo. Bisogna rivedere delle regole, magari quelle dell'autorizzazione preventiva? Andiamo da rivederle. Bisogna rivedere le regole autorizzatorie? Andiamo a rivederle. Non ci possono essere zone franche e non ci possono essere tabù quando si parla di riforme. Signor Presidente, da qui occorre ripartire, ancora prima di parlare della quantità di risorse a disposizione. Su questo mi permetto una considerazione che rivolgo al Parlamento: in troppi interventi si è sentito parlare della quantità di risorse a disposizione e non del modo con cui le stesse devono essere spese, delle regole che devono essere alla base della spesa. infatti che c'è un nodo nella capacità di utilizzo delle risorse, che non rende le stesse efficaci a tutte le latitudini del Paese. Su questo l'impegno del Governo deve essere massimo e determinato. e resilienza occorre essere determinati e concreti nel dare corso alle riforme necessarie a recuperare il *gap*, a partire dalle attività produttive. Signor Presidente, in questi mesi gli italiani sono stati indotti ad avere fiducia rispetto al Piano: non possiamo permetterci di tradire questa fiducia. Dobbiamo dare agli italiani fiducia ed averla negli stessi, per rialzare il Paese. Le riforme necessarie le abbiamo chiamate per nome e cognome e abbiamo voluto che fossero inserite in maniera chiara e determinata anche nella proposta di risoluzione che tra poco ci accingeremo a votare: la riforma della pubblica amministrazione, volta a favorire la semplificazione e l'efficacia dell'azione amministrativa; la digitalizzazione dei servizi; gli investimenti in capitale umano e in ricambio generazionale; la riforma della giustizia, volta a garantire la riduzione dei tempi dei processi e a smaltire gli arretrati giudiziari, e la riforma del Fisco. Quest'ultima, pur non ricompresa nel PNRR, è parte integrante della strategia di Governo e vogliamo che sia attuata dalla A alla Z, per dire agli italiani che le risorse che stiamo dando loro non saranno poi costretti a restituirle con lacrime e sangue insieme alle tasse. sfruttare al massimo gli spazi di collaborazione tra il pubblico e il privato. Questo è un Paese che ha sempre sviluppato economie pubbliche, ma che fatica ad intraprendere economie di mercato; bisogna mettere in sinergia la capacità pubblica e quella privata affinché ci rialziamo tutti assieme, senza che una sia di ostacolo all'altra. È un Piano strategico per tutto il Paese. È un Piano nel quale sono scritti nero su bianco i principi di destinazione della spesa e degli investimenti, al Nord e al Sud, al termine dei quali vogliamo che finalmente possano essere colmate tutte le distanze che ancora esistono in Italia, non solo tra Nord e Sud, ma anche tra centro e periferia. Consiglio, se cresce il Sud, cresce tutta l'Italia; se non riparte il Nord, non riparte tutta l'Italia Per ottenere questo occorre il nostro massimo impegno, lo ribadisco ancora; occorre rompere le incrostazioni burocratiche e spazzare via i reiterati esempi di incapacità di spesa che negli anni ci hanno regalato un infelice primato, quello di vedere l'Italia nella classifica dei Paesi che non hanno saputo spendere i fondi europei assegnati.

Parafrasando quello che Cavour ebbe ad affermare rispetto alla Corte dei conti quando fu costituita, vogliamo un'azione di controllo e di monitoraggio forte e indipendente del Piano, che garantisca il Parlamento e gli italiani rispetto al successo e all'azione degli investimenti messi in campo, in maniera determinata. Prima abbiamo raccolto anche qualche dichiarazione che cercava di provocarci, ma non ci facciamo caso, facciamo caso, perché siamo al Governo per spirito di servizio nei confronti del Paese. Se qualcuno pensa di poterci provocare in questo senso, gli diciamo in maniera simpatica di stare sereni, al Governo ci siamo e ci restiamo per l'interesse degli italiani, non ci interessa altro! signor presidente Draghi, invece diciamo di andare avanti con passo determinato, a partire dalle riforme. Indietro non si torna, ma non possiamo neppure permetterci di rimanere fermi nel dubbio su quello che va fatto. Siamo passati velocemente dal «ce lo chiede l'Europa» alla volontà di essere protagonisti e tenere ben saldamente in mano le redini del nostro futuro. Su queste basi, signor Presidente, ci accingiamo a votare a favore della proposta e ad augurarci che questo PNRR abbia il suo futuro e abbia la ripresa dell'Italia saldamente nelle nostre mani.

di questo Piano lei ha parlato come di: «un lavoro che ha grandemente beneficiato dell'azione già svolta dal precedente Governo». Sono parole, queste, che non possiamo non ascoltare con soddisfazione in un mondo come quello della politica, che spesso ignora il valore della riconoscenza, della gratitudine e del rispetto. Lei poi, personalmente, si è anche scusato per i tempi ristretti - li ha chiamati così - con i quali il PNRR è arrivato in Parlamento. Scuse non necessarie per chi come noi ha vissuto quella crisi di Governo del mese di gennaio che ancora oggi resta inspiegabile anche alla luce delle sue stesse parole. Sono scuse non necessarie per un ritardo che ha un padre, un nome e un cognome, un modo di intendere la politica come fatto personale, sopra un palcoscenico di cinismo e di vanità. *(Applausi)*. Un tipo di politica, un modo di fare politica che ci auguriamo sia definitivamente tramontato. Le sue parole di gratitudine ci fanno piacere, Presidente, perché dietro questo *recovery plan* c'è la storia recente del nostro Movimento, c'è la sfida accettata e vinta di Giuseppe Conte, che in quel lontano 25 marzo del 2020, come capofila di un gruppo di otto Governi, dentro il quale si trovavano anche la Francia e la Spagna, scrisse una lettera al commissario europeo chiedendo più risorse europee e un debito comune europeo per finanziare quelle risorse. *(Applausi)*. Sembra tutto facile oggi, sembra tutto scontato,

nessuno all'inizio. Una scommessa come tutte le scommesse del MoVimento 5 Stelle: difficili, difficilissime, quasi impossibili, se non per sognatori, concreti e generosi, che in questi mesi stanno portando avanti un processo globale per un'economia capace di prendersi cura della gente e del pianeta.

ha avuto in consegna, simbolica e virtuale, questo capitale di reputazione e di credibilità, che noi ci siamo guadagnati con il Governo precedente e che affonda le sue radici nel disinteresse e nel bene comune. A proposito però di disinteresse e di bene comune siamo sempre stati molto chiari; noi siamo entrati in questo Governo, raccogliendo l'invito del Presidente della Repubblica per un duplice scopo. per difendere i soldi della rinascita degli italiani dagli artigli di alcune *lobby* e dagli appetiti delle note consorterie italiane. per realizzare un grande piano europeo per una stagione nuova e diversa che porti verso uno sviluppo finalmente equo e solidale. Da questo punto di vista, presidente Draghi, non tutto ci convince di questo Piano; non ci convincono le politiche del mare, non ci convincono le politiche sulla qualità dell'aria e sull'abbattimento delle polveri sottili, non ci convincono le deboli politiche verso la mobilità sostenibile, di cui parlava anche il nostro presidente Pesco, non ci convincono le politiche sulla transizione energetica delle nostre aziende e delle nostre industrie,

Lo so, è un tema molto dibattuto e noi non vogliamo salire sulla giostra o dentro il balletto dei numeri e delle cifre.

A noi importa, Presidente, che lei oggi abbia parlato di indifferibili riforme e di potenziate capacità Vede, Presidente, lei ha detto che in questo *recovery plan* sono in gioco i valori sociali e la vita delle persone, una bella frase. Noi aggiungiamo che è in gioco soprattutto la vita dei cittadini più deboli, delle donne, dei giovani, di chi ha scelto coraggiosamente di continuare a vivere nel Mezzogiorno, di chi non è scappato dal Mezzogiorno. allora, non come un fatto di divisione politica, ma riconosciamo apertamente il ruolo che il Mezzogiorno ha avuto nella determinazione delle quote di risorse europee che sono andate all'Italia. all'Italia. *(Applausi)*. Abbiamo molto apprezzato l'indicazione sulla essenzialità delle riforme e da questo punto di vista ci permettiamo di darle un'indicazione, Presidente: faccia attenzione ai bandi del *recovery plan*, perché laddove sarà assente una quota garantita al Mezzogiorno, i soldi finiranno dove ci sono maggiori capacità progettuali, cioè al Nord e sarà la fine di tutto. *(Applausi)*. Sarà un treno perso per sempre, perché il Sud merita di più, diciamolo senza tono polemico,

attraverso una quota garantita nei bandi e negli investimenti. *(Applausi)*. Solo così il Sud potrà tornare a crescere e rilanciarsi, perché altrimenti dalle parole non riusciremo a passare ai fatti. Infine, da un impegno che vogliamo che oggi lei prendesse sul Sud, passo ad un impegno che invece in queste ore lei si è preso in Aula: la proroga al 2023 del superbonus 110 affinché questa misura possa sprigionare tutte le sue potenzialità, non si può prescindere dalla proroga al 2023. Glielo ha chiesto il Parlamento, glielo hanno chiesto le associazioni di categoria, i sindacati, ANCE, Confedilizia, gliel'ha chiesto e glielo sta chiedendo tutto il Paese e lei si è impegnato e per noi il suo impegno personale in quest'Aula resta agli atti e diventa legge. *(Applausi)*. Il superbonus

questo Governo ha abbracciato la svolta della transizione ecologica e su questo corrono continuamente segnali politici forti e chiari. La nostra proposta, già fatta alla Camera, è che si istituisca una Commissione bicamerale speciale per il *recovery plan*, perché il *recovery plan* sia un treno sul quale possano salire tutti, ma soprattutto possano salire i nostri figli, che non chiedono altro se non una certezza del domani. *(Applausi)*.

Caro presidente Draghi, lei ha calato in Parlamento questo PNRR, lo ha imposto con una modalità tecnocratica vecchia e fallimentare. Le criticità rilevate sono tante, i soldi alle imprese e all'Alta velocità impegnano un quarto delle risorse, mentre alla sanità territoriale solo il 3,7 per cento, sette miliardi in sei anni. La pandemia non ha insegnato nulla. Mi chiedo dove sono finiti coloro che invocavano il MES per la sanità e hanno fatto cadere un Governo per questo. Il Piano archivia l'economia circolare, prevedendo ancora investimenti in energia da combustione, biogas e biometano, archiviando la valutazione di impatto ambientale.

Il Sud, ancora una volta, è umiliato e dimenticato, nonostante le indicazioni europee. Quanto alla scuola, vi è praticamente una riproposizione della pessima buona scuola, con scuole di serie A e scuole di serie B. Infatti, scegliere maestri migliori vorrà dire che a qualcuno arriveranno i maestri peggiori e quindi la disuguaglianza - e lo dico proprio ai campioni dell'uguaglianza sociale - verrà insegnata sui banchi delle scuole elementari.

Il 30 aprile questo Governo presenterà in Europa un Piano mai sottoposto al dibattito pubblico e - ripeto - trasmesso al Senato solo ieri. Poteva essere la grande ultima occasione per una vera rinascita del nostro Paese, un cambio di paradigma; invece, di nuovo, come il suo Governo, si tratta della restaurazione di un sistema di lobbisti e interessi antichi, senza coraggio e visione. Presidente Draghi, fiumi di soldi per domani non basteranno se le idee restano quelle di ieri o addirittura di un secolo fa.

il Governo stima che gli investimenti previsti nel piano avranno un impatto significativo sulle principali variabili macroeconomiche nel 2026, anno di conclusione del piano. Il prodotto interno lordo sarà di 3,6 punti percentuali più alto rispetto all'andamento tendenziale e l'occupazione sarà più alta di 3,2 punti percentuali; gli investimenti previsti nel Piano potranno inoltre apportare miglioramenti negli indicatori che misurano i divari regionali e l'occupazione femminile e giovanile; certamente - e ci mancherebbe che non fosse così - anche se nel 2020 abbiamo perso 8,9 punti percentuali. Si tratta di un'iniezione di capitali mai vista nell'economia del Paese, pari a due piani Marshall della ricostruzione. Eppure nel 2026 non saremo neanche a metà del cammino per tornare alla situazione precedente. Quindi, noi stiamo faticosamente puntando a tornare indietro ed è questo lo sbaglio. Avremmo avuto la possibilità di imparare dagli errori e modificare il modello e la stiamo sprecando. La nostra meta è sola quella di tornare al *day before* la pandemia,

i rischi che la criminalità possa approfittare sono enormi, perché sta passando l'idea che bisogna spendere senza porsi troppi problemi, considerando le regole come sempre di intralcio. La *deregulation* è la situazione che le mafie preferiscono perché possono mettere in campo le loro capacità di convincere, cioè l'intimidazione e la corruzione. Bisogna avere il coraggio di dirlo con chiarezza: il *recovery* è una grande occasione per il Paese, ma può diventare un rischio enorme e non può essere l'occasione che le mafie attendono per prendersi la loro rivincita contro le istituzioni. La cosa che più mi preoccupa è la capacità delle nuove mafie di mimetizzarsi, non più con la coppola e la lupara, ma con la cravatta e la grisaglia. Una mafia che preoccupa meno anche un'opinione pubblica...

Aggiungo alcune osservazioni ancora. Avrei voluto dire che il Piano non è una risposta adeguata alla pandemia, che non si occupa in modo efficace delle cause che l'hanno generata, riconducibili al degrado dell'ambiente. Faccio solo

si parla nel Piano di una profonda semplificazione. Dobbiamo intenderci. Tutti vogliamo raggiungere gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile, ma a scapito di cosa? Della devastazione del nostro territorio? Lo trovo inaccettabile. La VIA è un presidio che va migliorato, responsabilizzando le aziende e non eliminando passaggi procedimentali necessari. Secondo alcune stime riportate nel Piano (quindi leggo esattamente quello che dice il Piano), considerando l'attuale tasso di rilascio dei titoli autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte eolica, sarebbero necessari ventiquattro anni per raggiungere il *target* Paese; mentre, con riferimento al *target* del fotovoltaico, ci vorrebbero cento anni, senza la modifica dell'attuale quadro normativo sulla VIA. E secondo voi la semplificazione dovrebbe essere sui tempi? Invece no! Questo potrebbe comportare un'accelerazione del consumo degli *habitat* terrestri e marini, tale da non consentire più la loro rigenerazione e, quindi, a discapito del capitale naturale. voi lo sapete bene. Si stanziano risorse a favore del Po: va benissimo. E gli altri fiumi? Solo il 43 per cento dei corpi idrici italiani e solo il 20 per cento lacustri raggiunge lo stato di qualità buono. Perciò serve un programma nazionale di rinaturazione e manutenzione di fiumi, laghi, lagune e zone umide. Sull'agrovoltaico, mi chiedo come sia possibile, in un Paese come il nostro, con un consumo di suolo altissimo e un settore agricolo che è un'eccellenza, decidere di destinare terreni agricoli alla produzione di energia rinnovabile. Così si sottrae terreno a cibo di qualità a cibo di qualità e si degradano i servizi ecosistemici del nostro straordinario suolo italiano. *(Applausi)*. Da ultimo, un altro aspetto che mi preoccupa molto è quello della abrogazione e revisione delle norme che alimentano la corruzione. Con la quantità di finanziamenti che arriveranno bisogna tenere alta l'attenzione e non introdurre semplificazioni normative in relazione...

l'impianto culturale del suo *Premier*. Respingevo la sua formazione e la sua azione da perfetto banchiere centrale. la sua spietata bravura non si allinea con il dolore di una società che sta piangendo con dignità e a cui imporrete altre riforme sociali distruttive. L'Italia non sarà più la stessa, perché la state smontando delle sue caratteristiche virtuose. Quando il Governatore dell'Italia chiede di mettere dentro il Piano di ripresa e di resilienza le vite degli italiani, dice il vero. Le vite degli italiani, i risparmi degli italiani, in cambio di prestiti avvelenati. State svendendo un'altra volta le piccole e medie imprese. Le vite degli italiani sono invisibili al suo freddo sguardo. Sono vite sospese tra bollette vergognosamente care e rate di mutuo da pagare con la paura di perdere la casa, il negozio, il capannone. Le vite degli italiani arrancano nella sfida generazionale tra genitori e figli per un contratto di lavoro vero, dove i diritti sono appesi a un filo. Il presidente Draghi si pone come figura garante presso l'Europa perché il suo *curriculum* offre abbondanti garanzie mercatiste e neoliberiste. Glielo dissi già una volta: lei incarna quella cultura che ha sostituito le vite delle donne e degli uomini con i numeri, i diritti con gli equilibri contabili. Il suo mondo di riferimento non può intercettare le spaccature sociali, perché il suo campo visivo è finanziario e non politico; il *recovery* *fund* è un pessimo affare; è un tradimento. Il *green* è un imbroglio semantico, altro che ecosostenibilità! La vita degli italiani, che lei infila in questo piano, non ha pieni diritti; è piuttosto mera esistenza infilata in un mondo disegnato con il compasso dall'*élite*. Volete più mercato nell'energia e nelle concessioni autostradali? Ma non vi bastano i bidoni che avete venduto dal Britannia in avanti? Ai Benetton e agli altri soci di Atlantia darete adesso 400 milioni di ristori, in barba alle frustrazioni dei ristoratori e degli altri operatori economici al collasso, che per lei, però, sono aziende *zombie*. L'*ex* capo di Vodafone, Colao, si è preso McKinsey per scrivere un'agenda digitale che progressivamente spingerà i lavoratori e i professionisti fuori dal mercato del lavoro e sarà il mondo dell'automazione e dell'algoritmo. Questo piano è la rete perfetta dopo impigliare le vite e il futuro degli italiani. Lei potrà garantire anche presso l'Europa, ma si metta nel taschino una pagina memorabile del romanzo «Furore»: «Le strade pullulavano di gente assettata di lavoro, pronta a tutto per il lavoro. E le grandi imprese e le banche stavano scavando la fossa con le loro stesse mani, ma non se ne rendevano conto. E la rabbia cominciò a fermentare». Non abusate della pazienza degli italiani; potreste pentirvene amaramente.

Signor Presidente, presidente Draghi, durante la lunga discussione di oggi sono state molte le critiche nei suoi confronti riguardo la ripartizione dei fondi fra Regioni del Nord e Regioni del Sud. Nella sua replica, dopo un lungo passaggio dedicato a snocciolare i numeri e a cercare di smentire la narrazione fatta dai tanti Gruppi presenti, c'è stato un passaggio in cui lei, quasi *en passant*, rimproverava la classe dirigente delle Regioni del Sud per l'incapacità del passato e anche dell'immediato presente di saper gestire i fondi avuti a disposizione finora. È stata un'affermazione senza dubbio legittima, anche se, a mio avviso, leggermente populista oppure - se vogliamo - leghista alla vecchia maniera. ciò che mi ha fatto, però, sorridere amaramente è stato che, a seguito di questa affermazione, si sono levati una serie di applausi da una parte dell'emiciclo, soprattutto quello alla sua destra, e da tanti colleghi, che forse, avendo perso la memoria nell'immediato, hanno scordato che diverse Regioni del Sud italiano, a partire dall'Abruzzo, dal Molise, dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Sicilia e passando per la Sardegna, sono amministrate attualmente dal Centrodestra. Presidente, lei ha una grandissima occasione. Visto che l'impegno che le viene chiesto dai Gruppi di maggioranza è di trasmettere il Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione europea, di assicurare il pieno svolgimento del Parlamento, nonché la leale collaborazione con le Regioni, le Province e gli enti locali, la pregherei di allegare allegare al Piano anche una raccomandazione ai Presidenti di quelle Regioni ad agire meglio rispetto al passato e, quindi, a garantire ai cittadini di quelle Regioni e di quei Comuni il giusto riversamento del denaro dovuto. Lei ha fatto anche un altro passaggio a proposito

Presidente, annuncio il mio voto di astensione, che non è completamente di opposizione in quanto vorrei che questi soldi, grazie alla collaborazione di tanti colleghi perbene, anche se non tutti, arrivassero finalmente ai cittadini italiani. il Piano che ci ha presentato è insufficiente o addirittura controproducente in materia ambientale. Prefigura il depotenziamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, si disinteressa sostanzialmente dell'economia circolare, non coglie l'occasione di un complessivo piano di bonifica e messa in sicurezza del territorio, stanzia pochi fondi per potenziare il trasporto pubblico e far diminuire lo smog nelle città. Il suo Piano è poi pericoloso nelle prospettive di riforma: prevede assunzioni nella pubblica amministrazione senza concorsi, fa prevalere le consulenze e le *task force*, depotenzia i presidi anticorruzione e antimafia

deresponsabilizza gli amministratori pubblici mediante scudi in caso di colpa grave. Il Piano annuncia nuove privatizzazioni, meno controlli e un'ancora più marcata concorrenza; prevede aiuti alle imprese medio-grandi, ma si disinteressa dei piccoli produttori: degli artigiani, dei commercianti, dei lavoratori, dei disoccupati e non destina che pochissimi fondi alla ricerca e alla lotta alle disuguaglianze. È poi caratterizzato da genericità e mancanza di chiarezza. Il Parlamento è stato preso in giro con il deposito di un Piano modificato ieri, a poche ore dalla presentazione alla Camera. lei sta eseguendo il compito che le hanno assegnato in Europa; sta gettando le basi infrastrutturali, economiche, normative e financo culturali favorevoli alle poche grandi imprese del Nord Italia a discapito di tutto il resto. Siccome lei non ha avuto rispetto del Parlamento, io non ne avrò per lei e le dirò quel che tutti qui pensano ma non hanno il coraggio di dirle. Presidente Draghi, il suo Piano è come la corazzata Potëmkin di fantozziana memoria *(Applausi)*, e lei sta ipotecando il nostro futuro su mandato straniero. L'Alternativa C'è non la perde d'occhio e resisterà a questo progetto. Per questo, a differenza di altre forze, che blaterano ma poi si allineano, voteremo contro la risoluzione di maggioranza e a favore di quella alternativa da noi depositata.

giorni fa, il «Financial Times», tra i più liberisti dei quotidiani europei, fautore del mercato senza regole e del primato della finanza sull'economia, classificando il *crack* Lehman Brothers e le cicliche crisi sistemica globali che hanno falcidiato milioni di posti di lavoro, la distruzione dei risparmi depositati o investiti in banca come incidenti della storia, non distinguendo la realtà dai luoghi comuni, ha appellato l'Italia come delinquente d'Europa, arrecando gravissima offesa all'Italia e agli italiani. Per omaggiare lei che, da Presidente della BCE, ordinò la chiusura degli sportelli bancari causando indicibili privazioni, aumento della mortalità infantile e terribile sofferenza della popolazione più debole (vecchi, donne e bambini greci), il «Financial Times» si è permesso di marchiare l'Italia con l'epiteto di delinquente. Come riportato dal quotidiano nei titoli, l'Italia, che è sempre stata vista come il giovane delinquente d'Europa, è ora diventato il modello europeo, tra il disinteresse della politica e il masochismo dei partiti che hanno governato dal 2018 il Paese. Si aggiunge che Draghi presenterà il suo Piano all'Europa, fatto di riforme strutturali, considerate fondamentali e così via, e che e che l'Italia gestirà il suo più grande *deficit* di bilancio dall'inizio degli anni Novanta e per ora i mercati finanziari, preoccupati spesso per il debito pubblico, restano indifferenti, segno di fiducia nel nuovo *Premier.* Tra luoghi comuni e mistificazione, omettete di ricordare che il duro negoziato per ottenere il *recovery* *fund* venne portato avanti dal Governo Conte, defenestrato da una congiura di Palazzo; che lo *spread* sui titoli di Stato, oggi attestato a 107, col precedente Governo era sceso sotto i 100 punti; la quotazione media di alcuni BTP decennali deprezzati tra i 10 e i 18 punti (ad esempio il BTP al tasso del 2,80). Nei giochi di prestigio da mago Silvan, il Governo che rappresenta il modello europeo ha fatto sparire la versione del PNRR, come già ricordato, per non parlare del superbonus, formidabile strumento di ripresa dell'economia assieme ai crediti fiscali, che, invece di essere finanziato fino al 2023, è stato sostituito dalle solite promesse scritte sulla sabbia, dell'assenza del salario minimo e di quota 100, della consueta razzia dei fondi destinati al Sud e alla ricerca. Insomma, la propaganda sovrasta la realtà e la penuria di finanziamenti per il sociale. ricordando ai pavidi smemorati la massima di Don Abbondio, per cui se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare, e annuncio il mio voto di astensione. Grazie, signor Presidente, e buona fortuna.